del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,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

oggi, novembre 2023, intende attivare una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pregressa gestione dell'emergenza Covid-19. Ricordo a tutti qui che il 31 dicembre 2019, quattro anni fa, la commissione sanitaria di Wuhan in Cina segnalò all'Organizzazione mondiale della sanità un *cluster* di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan. Quattro anni fa quindi cominciò, per il mondo intero e per il nostro Paese, uno dei periodi più incerti del dopoguerra. Ben presto i sentimenti dominanti furono la paura, l'angoscia e la morte. Ci trovammo tutti a lottare contro qualcosa di sfuggente ed invisibile, un virus nuovo, di cento nanometri, che si diffondeva per via aerea ed era pericoloso e letale.

ci fanno comprendere l'estrema gravità di questa epidemia. Oggi, a distanza di quattro anni da questi tragici giorni, con una finalità che io

ha rinunciato alle cure, dal sottofinanziamento del Sistema sanitario nazionale, dalla mancanza di medici e infermieri, dalla medicina territoriale delle cure primarie e dalla privatizzazione sempre più spinta del bene salute, bene salute, questa maggioranza e questo Governo trovano la volontà di istruire un processo, un'inchiesta sulla gestione della pandemia, mentre secondo noi ci vorrebbe un'inchiesta su come è stato smantellato pezzo per pezzo il sistema sanitario nazionale. *(Applausi)*. Altro che Commissione Covid! È evidente che il motivo per cui il Governo intende istruire questa Commissione d'inchiesta annida le proprie radici nella volontà di sputare veleno contro Giuseppe Conte, che invece ha messo in sicurezza questo Paese nel momento più delicato della propria storia repubblicana.

perché forse vale la pena di farlo: aver messo in campo misure rapide e tempestive per contenere la diffusione del virus, aver collaborato senza sosta con gli altri Stati del mondo e ancora aver messo in campo ingenti finanziamenti per potenziare il sistema sanitario (11 miliardi), aver adottato una comunicazione chiara e trasparente con la popolazione, aver messo in sicurezza le fasce deboli della popolazione e ancora aver implementato in misura significativa il piano di ripresa economica europea con il PNRR. PNRR. Onorevoli colleghi, anziché concentrare le proprie forze per trovare risposte alla galoppante crisi economica, all'acuirsi della guerra in Ucraina, al conflitto in Israele, questa maggioranza questa maggioranza ha la faccia tosta di distogliere energie dal Parlamento per canalizzarle lungo il solco di un'arena politica. Di questo si tratta; abbiate il coraggio di dirlo agli italiani. Desiderate ardentemente solo ed esclusivamente lo scontro politico e non ve ne frega nulla di far luce sulle eventuali criticità gestionali verificatesi durante la pandemia. Perché diciamo questo? Perché non ve ne frega nulla di verificare la verità fattuale. Se infatti così fosse, tra le funzioni di questa Commissione avreste previsto anche quella di far luce sulle responsabilità delle Regioni, che durante i mesi della pandemia hanno ovviamente contribuito alla realizzazione delle ordinanze che provenivano dal Governo. Quindi è vergognoso che si istituisca una Commissione senza avere la possibilità di chiamare in causa gli assessorati, i Presidenti delle Regioni, le Aziende sanitarie, sanitarie, le RSA. È veramente vergognoso. *(Applausi)*. Tutti ricordiamo il ritardo nella risposta iniziale delle Regioni. Ricordiamo il ritardo della Lombardia e del Piemonte, che erano rette da Governi di centrodestra. Forse non vogliamo chiamare in causa questi Presidenti e non vogliamo chiamare in causa chi oggi governa la barca? Quindi vi chiediamo di essere trasparenti su questo. La trasparenza per noi è chiamare in causa tutti gli attori che hanno concorso effettivamente a generare la gestione della pandemia. Vorrei anche dire che questo atteggiamento di scarsa trasparenza probabilmente è stato dettato da una volontà di nascondere sotto il tappeto la scarsa disponibilità - lo abbiamo visto all'inizio - dei letti ospedalieri, dell'offerta ospedaliera

ricordo che era compito delle Regioni distribuirli, quindi non potremo indagare effettivamente anche su questa assenza di dispositivi

della maggioranza, perché non avete deciso di estendere l'attività di inchiesta anche all'operato delle Regioni? Perché avete impedito al popolo e a noi di fare luce su quello che è successo nelle varie Regioni italiane? Avevano piani di emergenza adeguati, pronti ad affrontare questa emergenza sanitaria? Hanno fornito informazioni tempestive accurate sullo sviluppo della pandemia, coinvolgendo esperti scientifici e contrastando la diffusione e la disinformazione? Hanno garantito la trasparenza e l'accessibilità ai dati epidemiologici? Oggi tutte queste cose, compresa la possibilità di capire cosa è successo nelle RSA, non le potremo sapere. Non sapremo mai che cosa veramente è successo, nonostante il fatto che potremmo istruire una Commissione bicamerale sulla pandemia. pandemia. Quindi dobbiamo riconoscere con onestà intellettuale che non saremo in grado di addivenire ad una verità. Dunque, ci resta da dire che formalmente

cosa effettivamente le Regioni potranno fare successivamente, perché non avremo indagato dove è avvenuto il corto circuito. Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle chiede in realtà una riforma del sistema sanitario nazionale, con l'obiettivo - vi ricordo - di conferire maggiori poteri allo Stato e rivedere il Titolo V della Costituzione. Vogliamo deframmentare la *governance* della sanità invece di frammentarla ulteriormente con autonomie che provocheranno ulteriori asimmetrie regionali? Lo dico più chiaramente possibile: fa specie che, innanzi a questo quadro nefasto, anziché avocare a sé la materia sanitaria, questo Esecutivo stia accelerando la concessione di ulteriori forme di autonomia che condurranno a morte la sanità pubblica a favore di quella privata. Onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle ritiene che sia compito delle istituzioni concentrare i propri sforzi per garantire cure adeguate, per promuovere per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca scientifica. Ma per farlo occorre avere un approccio maturo e costruttivo, promuovendo la collaborazione e concentrando i propri sforzi sulla tutela della salute e delle persone. Infatti solo attraverso una risposta unitaria e coordinata potremo superare questa e altre crisi e prepararci alle sfide che ci aspettano. Tutto il resto, compresa questa Commissione, non interessa; è solo propaganda, è solo una lotta contro il nostro *leader* politico Giuseppe Conte, e noi ci sottraiamo a questa propaganda e a questo tipo di lotta politica *(Applausi)*; non interessa neanche ai 60 milioni di italiani.

7 milioni di morti al mondo, 770 milioni di contagi, 13 miliardi di vaccini somministrati sono solo tre numeri che ci dicono con chiarezza cosa sia stata la diffusione pandemica del Covid, la sua dimensione e l'impatto sui sistemi sanitari. Una catastrofe che dovrebbe imporre ad ogni Governo di mettere a punto strumenti e programmi per contrastare efficacemente il possibile ripetersi di un fenomeno di questa portata. La proposta di questa Commissione non nasce però con l'intento di affrontare i fatti avvenuti durante il periodo pandemico in connessione col funzionamento del sistema sanitario italiano. Non intende mettere in discussione il sistema che non ha funzionato per migliorarlo. Drammaticamente, si pone soltanto altre questioni: mettere in discussione chi in quel momento drammatico ha assunto decisioni. Sin dall'inizio il Partito Democratico ha chiesto che fosse istituita una Commissione indipendente tecnica che avesse il compito di comprendere il funzionamento del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza e individuare, di conseguenza, i necessari miglioramenti per il presente. Mentre si discute, non si ferma il contagio; purtroppo sta andando ancora avanti, anche se con aspetti molto meno drammatici di quello che abbiamo vissuto. Abbiamo chiesto che la Commissione avesse il compito di verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei piani pandemici nazionale e regionali, con l'attuazione di quanto previsto, in particolare nelle fasi inter-pandemiche. Era necessario che la Commissione avesse il compito di verificare lo stato di attuazione da parte delle Regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, lo *standard* delle condizioni di accesso in relazione ai livelli essenziali di assistenza, nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, il numero dei posti letto per pazienti acuti o subacuti nei reparti di terapia intensiva, allo scopo di migliorarne l'offerta dei servizi ai cittadini su tutto il territorio nazionale. individuare soluzioni per un maggior controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private. Siamo convinti che fosse questo il giusto lavoro da portare avanti: una Commissione che aiutasse a prevenire le problematiche emerse durante la pandemia Covid, che aiutasse il sistema sanitario nazionale a farsi trovare pronto in un'altra drammatica eventualità. Ognuno ha il suo vissuto di quel periodo, non è stato uguale per tutti. Il mio vissuto è stato il vissuto di una sindacalista che, insieme ad altri, insieme a altre organizzazioni datoriali e categoriali, insieme al Governo, insieme alle Regioni, ha dovuto affrontare in quel momento scelte non facili. Decidere quali aziende si dovevano tenere aperte, quali dovevano essere momentaneamente chiuse, non sapendo nemmeno per quanto, quali servizi, anche con un rischio alto dei lavoratori e delle lavoratrici addette a quei servizi, dovevano comunque essere garantiti. Bene, sembra che quel momento ce lo siamo scordato. Ci siamo scordati i treni di Bergamo, ci siamo scordati i morti nelle RSA *(Applausi)*, ci siamo scordati che, se non si fossero chiuse le scuole (altra scelta

Abbiamo avuto testimonianze di un coraggio estremo, quello degli infermieri e delle infermiere, dei medici *(Applausi)*, di chi lavorava nella sanità, che per mesi non è andato a casa, per paura di contagiare i propri familiari; quello dei medici e dei sanitari che sono morti contagiati, ma anche quello delle commesse, dei magazzinieri e dei commessi, che hanno lavorato in quel periodo nei supermercati per garantire i servizi ai cittadini e alle cittadine. Ci siamo dimenticati quel vissuto. Abbiamo archiviato nella nostra testa quelli che in quel momento abbiamo definito i nostri eroi e a cui la finanziaria non destina risorse anzi penalizza, a partire dalla loro pensione. Ci sono state inchieste della magistratura e ci sono state archiviazioni molto serie. Perché aprire nuove fratture istituzionali, cercando di orientare l'interpretazione dei fatti come un vero processo di allora, ai politici e a tutti noi? Il Paese non ha bisogno di questo, ma ha bisogno che ci siano investimenti, perché, in una tragica prossima volta, non si rimanga senza mascherine e non ci sia la mancanza totale dei respiratori, perché gli ospedali e le strutture sanitarie siano dotate di strumenti, a partire dal personale, per non combattere a mani nude come per tanto tempo prima del vaccino è successo nel nostro Paese. Non producevamo più mascherine, non producevamo più respiratori: troppo poco valore aggiunto. E abbiamo visto, davanti al contagio e davanti alle morti, quanto sarebbe stato prezioso da subito, immediatamente, avere almeno quegli strumenti a tutela dei sanitari, a tutela di tutti coloro che hanno continuato a lavorare senza mai saltare un giorno e a tutela dei cittadini e delle cittadine tutte. Non abbiamo imparato niente Io ho lavorato, in quel momento, avendo a fianco un Governo attento e governi regionali attenti. Si è fatto di tutto in quel momento, in ogni parte dell'Italia, con quel poco che c'era. Altro che strizzare l'occhio ai no vax! Quante morti si sarebbero potute evitare, se nessuno avesse strizzato l'occhio ai no vax, così interpreti e protagonisti in tanti *talk show* e in tanti momenti informativi anche di questo Paese. C'è stata davvero una noncuranza di questi aspetti, su cui dovremmo riflettere. C'è un punto politico, che non ha avuto finora alcuna risposta. Se vogliamo vedere come ha funzionato quel sistema e porvi rimedio, perché non affrontarlo anche rispetto alle scelte e alle gestioni delle Regioni? Io non riesco a capire perché, in un sistema sanitario che è di competenza delle Regioni, abbiamo escluso anche questa analisi; è dunque evidente che il tema è un altro. Questo tema non si affronta con il rancore, ma con la generosità e la coscienza di lavorare tutti insieme per il Paese.

rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, gli ultimi tre anni hanno rappresentato un momento di particolare rilevanza sociale e sanitaria per il nostro Paese e per il mondo intero. Abbiamo dovuto affrontare un'emergenza che ci ha messo alla prova sotto ogni punto di vista e ha segnato profondamente la nostra storia; è quindi indiscutibile che la complessità e l'urgenza abbiano richiesto risposte straordinarie da parte dei Governi e delle istituzioni; è altrettanto fondamentale riconoscere se queste decisioni siano state eque e improntate alla risoluzione del problema e non piuttosto figlie della fretta o dell'approssimazione, quando non di scelte squisitamente ideologiche e troppe volte prive di basi scientifiche. In quei giorni io e tanti, tra noi, abbiamo perso persone care, abbiamo rinunciato ad abbracciarle nell'ultimo saluto, abbiamo sacrificato con responsabilità la nostra libertà e la nostra socialità. Abbiamo dovuto stringere i denti abbassando le serrande dei nostri negozi in nome della sicurezza e della salute comuni. Eppure i dati ci mostrano chiaramente che l'Italia, pur essendo la nazione ad aver adottato tra le misure più restrittive, è anche quella che ha avuto il maggior numero di decessi. Colleghi, poiché parliamo innanzitutto di salute, di diritto al lavoro, di libertà personali, diciamo chiaramente che non è cinismo voler istituire una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria; cinismo è ignorare che parliamo di diritti umani fondamentali e di diritti sanciti anche dalla nostra Costituzione, che qualcuno ha preteso di nascondere sotto il tappeto di una mal definita sicurezza sociale. Pensate che questo non interessi agli italiani? Credo che innanzitutto non si debba dimenticare e che occorra far chiarezza, in primo luogo per dare risposta al dolore di tutti i familiari delle vittime che non hanno potuto avere neanche la dignità delle autopsie. Iniziamo col ricordare proprio la circolare del Ministero della salute del maggio 2020,

non ha permesso una definizione della causa esatta del decesso, che invece sarebbe stata utile per determinare le cure in tempi più brevi e quindi salvare molte vite. Questo non interessa agli italiani? Indagare su questo per voi è un tribunale politico o piuttosto tutelare il diritto alla salute? *(Applausi)*. Come non ricordare, poi, l'introduzione *sui generis* del *green pass,* immaginato in Europa per semplificare gli spostamenti all'interno dell'Unione ma diventato in Italia uno strumento di selezione delle persone e dei loro diritti, distinguendo tra chi poteva lavorare e chi non poteva, tra chi poteva pretendere un treno e chi non poteva, tra chi poteva accedere agli uffici pubblici e chi non senza tenere conto del fatto che il *green pass* ha prodotto danni economici enormi, danneggiando il turismo e la ristorazione, abbattendosi come la scure del triste mietitore sulle piccole aziende italiane, che da sempre hanno costituito i muri portanti della nostra economia. Siamo arrivati ad assurdi, come quello di equiparare i contagi sul posto di lavoro agli infortuni sul lavoro. Ancora più incomprensibile fu introdurre l'obbligo per i treni a lunga percorrenza e non per quelli locali o fermare un treno a metà corsa perché il macchinista aveva esaurito le quarantott'ore di validità del suo *green pass*. Chi governava allora disse di no all'esenzione dal *green pass* per i lavori all'aperto, dove non c'è pericolo di contagio, no all'esenzione dal *green pass* per chi lavorava da solo, isolato, no all'equiparazione dei bus turistici agli altri autobus, con un criterio ancora da spiegare. E infine disse i no più gravi: quello all'esenzione dal *green pass* per chi aveva avuto un'infezione da Covid rilevabile con i *test* anticorpali; il no a portarne a dodici mesi la validità per i guariti, nonostante tantissimi studi scientifici in tutto il mondo, anche molto dettagliati, evidenziassero come la guarigione da Covid desse una resistenza al contagio molto più affidabile e molto più lunga. Di contro, fu possibile per più di 4.000 persone partecipare a un *rave party* a Valentano, svolgere quindi una manifestazione non autorizzata, occupare abusivamente proprietà private, trasgredire tutte le norme di restrizione, oltre a quelle della legalità e del buonsenso, e, a chiosa di tutto questo, restituirci un ragazzo morto annegato nel laghetto antistante. Insomma, si controllavano tutti gli onesti cittadini, ma nessuno si era accorto dell'arrivo di questa folla a Viterbo e in compenso qualcuno pretendeva di controllare con i droni se persone per bene camminavano in spiaggia. Indagare su questo è per voi cinismo o piuttosto tutelare il diritto alla verità degli italiani? Tra le decisioni politiche errate, come non ricordare l'affare Azzolina, con migliaia di banchi a rotelle acquistati

lei prosegua, ma ovviamente anche il tono delle sue dichiarazioni può suscitare qualche reazione, immagino che sia anche previsto. La Presidenza prova a garantire ovviamente lo svolgimento del suo intervento, come

utili solo per giocare all'autoscontro, dismessi per la poca funzionalità, buttati in discarica in barba ad ogni regola ambientalista. Senza contare la poca trasparenza dell'acquisto di questi banchi *(Applausi)*, visto che ad un certo punto dal sito del Governo scomparvero 63 pagamenti per un totale di 137 milioni relativi a bandi connessi all'emergenza Covid. E allora indagare su questo è per voi cinismo o piuttosto tutelare il diritto degli italiani alla trasparenza e sapere come vengono utilizzati i soldi pubblici, i loro soldi? Ora, secondo le opposizioni, la risposta a tutte queste decisioni politiche errate e prese dai Governi sarebbe indagare le Regioni. Ma se davvero vi era una qualche responsabilità da parte delle Regioni, ci spiegate perché bocciaste, ad esempio, l'istituzione della Commissione Covid in Emilia-Romagna? *(Applausi)*. O forse l'Emilia-Romagna non è una Regione? Ci spiegate perché non avete proposto voi e prima di verificare l'operato della Giunta Zingaretti, Presidente - all'epoca - della Regione Lazio, vostro compagno di partito, per l'acquisto di mascherine acquistate e mai consegnate con un danno erariale di 11 milioni? Abbiamo visto le opposizioni scaldarsi in Aula durante il dibattito, ma vedete, la vostra agitazione è inspiegabile. Ve ne dà l'esempio ancora una volta il Parlamento europeo, che già nel marzo 2022, con responsabilità e senza paura, ha istituito una sua Commissione speciale sulla pandemia da Covid-19 con lo scopo di ragionare sugli insegnamenti tratti e sulle raccomandazioni per il futuro. Quindi, non andiamo fuori tema, cari colleghi, questo è anche lo scopo della Commissione italiana. E non capiamo il vostro vittimismo. O non può, secondo voi, essere utile analizzare quali sono state le falle e le scelte errate, farne esperienza per evitare di commettere gli stessi errori ed essere veramente prontissimi, come diceva qualcuno, in caso di un'altra emergenza? Davvero pensate che tutto questo non interessi agli italiani? Quindi dal *lockdown* della scienza al *lockdown* della politica, passando per i *lockdown* senza criterio a volte imposti agli italiani, sono molti i perché ai quali dare risposte. Il compito di questa Commissione sarà dare quelle risposte e il compito di questo Parlamento sarà impegnarsi affinché la verità e la trasparenza vincano sempre sulla faziosità e sulla manipolazione della salute con dogmi inaccettabili. Chi tra noi, colleghi, non porterà avanti questo impegno non risulterà più credibile agli occhi degli italiani.

Signor Presidente, vorrei provare a ristabilire un po' di verità dopo le cose ascoltate. Non so dove fosse la collega che mi ha preceduto nel 2020, ma io ero qui, ero senatrice ed ero in Commissione sanità, quella che ha affrontato realmente i problemi. *(Applausi)*. Ero tra quei colleghi che si sono trovati a dover rispondere ai cittadini italiani delle loro scelte.

cose dette, ma partiamo dai famigerati banchi a rotelle. Vorrei ricordare a tutti - come è stato ripetuto innumerevoli volte, ma evidentemente abbiamo un analfabetismo funzionale dilagante tra i membri della maggioranza i banchi a rotelle non sono stati acquistati dalla ministra Azzolina, che - poverina - ancora viene additata per questo. Il Ministero dell'istruzione ha messo a disposizione diversi tipi di sedute per le scuole e i dirigenti scolastici, in totale autonomia, quella stabilita dalle nostre leggi, hanno deciso quali erano quelle più opportune per le loro scuole. *(Applausi)*. Mi auguro quindi che sia l'ultima volta che dobbiamo ripetere questa spiegazione e che anche nelle menti poco aperte della maggioranza entri questo concetto elementare. contrario, a scuola, anche sui banchi a rotelle, ci dovreste tornare voi. *(Applausi)*. Per non parlare del fatto che della scuola vi ricordate solo per i banchi a rotelle, ma non quando si tratta di tirare fuori i soldi. Noi ci abbiamo messo 10 miliardi di euro e voi bruscolini, come si dice in alcune Regioni. E parliamo invece dei banchi a rotelle, solo perché non avete altri argomenti più solidi da trattare. Vorrei ricordare a tutti quanto sono stati drammatici quei primi mesi del 2020,

dei cittadini di questo Paese, e non per giocare a guardie e ladri. Il Governo di allora e quelli che sono seguiti dopo - il Governo Draghi che ha seguito il Conte 2 - hanno dovuto affrontare scelte difficili anche sulla limitazione delle libertà delle persone. Ma, al di là di quello che può scoprire una Commissione di inchiesta parlamentare, sulla limitazione delle libertà si è già pronunciata la Corte costituzionale diverse volte, stabilendo che la tutela della salute viene prima di qualsiasi altra cosa, in base a quello che è scritto nella nostra Costituzione. Ma voi la Costituzione la volete usare come carta straccia e non rispettarla. E questo è solo uno dei tanti esempi in cui pensate di rigirarla a vostro uso e consumo, senza nessuna base. Ne stiamo sentendo tante sulla Commissione d'inchiesta. Nessuno ha mai voluto opporsi a una seria, totale e globale Commissione d'inchiesta. L'abbiamo detto in tutte le sedi. È stato detto alla Camera, l'abbiamo ripetuto qui in Commissione sanità e lo stiamo ripetendo in quest'Aula. Il problema è che voi non volete scoprire che cosa non ha funzionato per dare verità e trasparenza ai cittadini italiani. Voi volete fare solo un processo politico a chi c'era prima di voi, perché volete strizzare l'occhio ai no vax e ai tanti complottisti che stanno lì fuori. *(Applausi)*. Di che cosa non ha funzionato realmente nella sanità e di che cosa andrebbe migliorato ce ne siamo già occupati nella scorsa legislatura, con un affare assegnato in Commissione, proprio per capire quali erano state le falle, soprattutto della medicina territoriale, e come riorganizzarla. Scienza: una questa sconosciuta nei vostri lidi. lo sapevamo tutti che cosa andava fatto e che cosa andrebbe fatto e che cosa andrà fatto per tutelare la salute dei cittadini italiani da qui in avanti. Anzi: da ieri in avanti, perché con qualsiasi interlocutore detto tutti la stessa cosa. E li abbiamo ascoltati in sedute pubbliche, e non segrete. La trasparenza, dunque, c'è: basta voler credere alla scienza e non agli untori, come al tempo dei Promessi Sposi. È inconcepibile quello che state facendo. Non si può indagare su quello che non ha funzionato o su quali possano essere stati i problemi della sanità o del Paese a causa del Covid-19, se non guardiamo a quello che è successo all'interno delle Regioni. Lo sapete benissimo che la sanità è regionale. Lo stabilisce l'articolo 117, sempre di quella Carta costituzionale che voi evidentemente non conoscete per questo come per tanti altri argomenti. E ritorniamo al problema di tornare a scuola, che vi farebbe molto bene.

altra competenza. Va bene: insomma, bisognerebbe imparare dai propri errori, ma evidentemente anche su questo avete qualche difficoltà. Vogliamo fare una seria Commissione d'inchiesta sul Covid-19? Allora non poniamo paletti, perché non si può pensare di puntare il dito solo contro il Governo, quando i problemi della sanità risiedono, se non solo, ma soprattutto all'interno delle varie gestioni regionali. E soprattutto risiedono anche nelle carenze di personale, nel *burn out*, in tutti quei problemi che abbiamo visto fino ad oggi, di cui parliamo continuamente e che voi invece, in questo caso, volete tranquillamente ignorare. I problemi stanno nelle differenze, nei LEA che vengono erogati in qualche Regione e in qualche altra no: da una parte il 90 per cento, da una parte il 70, da una parte il 60, con Regioni che non sanno gestire nel migliore dei modi e con altre Regioni che hanno privatizzato troppo. Ma allora diciamocelo che voi non volete inserire le Regioni all'interno di questa Commissione d'inchiesta, perché non volete che venga fuori quello che, in realtà, in parte,

È questo che voi non volete far venire fuori dalla Commissione: quella che dovremmo commissariare è la sanità lombarda, non il Governo che c'era nel 2020. Quando ammetterete che tutto quello che volete fare è solo distruggere o quantomeno indebolire ulteriormente il Sistema sanitario pubblico? Si vede anche dalla legge di bilancio che ci avete presentato, che è questo quello che volete fare. Perché non lo dite? Volete fare un attacco politico al presidente Conte. Non citate mai il fatto che il *green pass* e tutte le restrizioni sul lavoro le ha messe Draghi e non Conte. Sottolineiamolo questo, perché voi puntate sempre e solo il dito contro Giuseppe Conte. Dopo di lui, però, c'è stato il presidente Draghi e voi lo omettete continuamente. Oltretutto, nel Governo Draghi, quello contro cui state puntando particolarmente il dito, come nell'intervento precedente, sedevano due dei partiti che fanno parte di questa maggioranza. La Lega e Forza Italia erano parte del Governo Draghi e allora perché non ne discutete anche con loro? *(Applausi)*. State puntando il dito contro Conte, ma anche contro voi stessi. Avete dei problemi al vostro interno, dei problemi grossi che cercate di oscurare con bagarre e polveroni mediatici. Questa è la verità. Questo è quello che dovreste raccontare ai cittadini italiani e non il fatto che volete fare trasparenza. Dite che state strizzando l'occhio ai no *green pass*, ai no vax e volete fare un tribunale contro Giuseppe Conte e il ministro Speranza. Tutto questo vi si ritorcerà

Signor Presidente, intanto mi lasci ringraziare anche la collega Pirro che ha davvero riassunto molto bene quella che è la realtà. Tra ieri e oggi in quest'Aula ho ascoltato tante belle parole, degli interventi - devo dire - anche apprezzabili dal punto di vista dello sforzo retorico che alcuni esponenti della maggioranza hanno sostenuto nel cercare di dare delle motivazioni che fossero quanto meno decenti per l'istituzione in questo modo della Commissione d'inchiesta in esame. I problemi però sono perlomeno due:

chiunque si sarebbe aspettato un minimo di responsabilità da persone che siedono all'interno delle istituzioni, gridavano alle riaperture nei giorni dispari e alle chiusure nei giorni pari hanno dato uno spettacolo di se stesse assolutamente inconcepibile, da ghiacciare il sangue nelle vene. Chi propone l'istituzione di questa Commissione di inchiesta non è credibile. Qualcuno Qualcuno si illude che le persone abbiano la memoria corta, ma non è così. Purtroppo questa epidemia ha lasciato delle ha lasciato delle cicatrici profonde nella coscienza degli italiani e delle italiane e voi potete provare a dire e a fare qualunque cosa, ma non c'è nulla che potrà nascondere la falsa coscienza con cui voi state utilizzando uno strumento istituzionale per fini politici. questo disegno di legge di istituzione della Commissione d'inchiesta, che era già stato discusso alla Camera,

Provate a fare cassa - come si è detto - strizzando l'occhio a uno sparuto numero di persone - io credo che non siano in alcun modo la maggioranza, ma d'altra parte nemmeno i voti che vi hanno portato al Governo sono la maggioranza del Paese *(Applausi)* - che parla di siero invece di parlare di vaccino, che parla di pozioni magiche invece di basarsi sulla scienza. State avallando questa linea

è questo. Se l'avessimo fatta a trecentosessanta gradi, magari avremmo scoperto che Fontana non ha fatto proprio il massimo per la propria Regione dal punto di vista della sanità.

alla doppiezza anche del senatore Renzi, che ieri è intervenuto e ha detto sì, e infatti il suo partito ha votato contro la pregiudiziale

Lui parla del sindaco d'Italia ed è costretto per sopravvivere ad andare a fare convegni dallo sceicco d'Arabia.

Eravamo ancora in pandemia quando colui che oggi inneggia al sindaco d'Italia e fa capire che intende spalleggiare questo Governo e la sua maggioranza nel suo progetto di premierato, un *unicum* al mondo,

Voglio chiudere ricordando un altro tassello che vi toglie credibilità. Il prossimo

politico dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta, c'è un uso punitivo addirittura della legge di bilancio. Lasciatemi chiudere con una notazione. Visto che le forze di maggioranza hanno un'ossessione per i banchi a rotelle, io dico che questa è solo la vostra ennesima dimostrazione di ignoranza crassa. Ma non avete mai messo piede fuori dall'Italia, evidentemente? Io sì. Ho insegnato in Germania e sono stata in Finlandia, dove i banchi a rotelle, le postazioni mobili, sono uno strumento principe

Noi avremmo voluto che le istituzioni si impegnassero in una laica, sana, seria ricerca di come affrontare pandemie, di come affrontare situazioni emergenziali, come purtroppo è successo nel 2020. Ci troviamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione e all'ennesimo utilizzo degli stivali nelle istituzioni. E, quindi, ovviamente non può esserci l'avallo di queste modalità e finalità da parte del MoVimento 5 Stelle.

Signor Presidente, colleghi, Governo, vorrei prima di tutto fare una premessa, prima di entrare nel merito delle questioni che stiamo affrontando in questo provvedimento, e sottolineare un aspetto: credo fermamente nel valore delle idee politiche, che tra l'altro sono portate avanti in quest'Aula da ogni Gruppo e credo anche fermamente nel valore della diversità delle idee, che di solito genera ricchezza, che è il sale della nostra democrazia. Ma, quando si arriva a rappresentare il Paese, a essere istituzione, bisognerebbe farlo con serietà e rispetto. Questa premessa la trovo doverosa, perché mi preme sia chiaro un punto: nessuno, tra chi è seduto in questi banchi, ha qualcosa da nascondere rispetto al grande lavoro che è stato fatto in uno dei periodi più complessi e delicati della storia del nostro Paese. *(Applausi)*. Al contrario, lo rivendichiamo con forza. Rivendichiamo il coraggio delle scelte fatte. Rivendichiamo la serietà delle scelte prese. Rivendichiamo la linearità dei nostri atti. Mentre qualcuno aizzava e usava la piazza e strizzava l'occhio al mondo no vax, noi ascoltavamo e rispettavamo le indicazioni della scienza. Mai - e dico mai - abbiamo dato seguito alla pancia del Paese o, peggio ancora, alla ricerca del consenso. *(Applausi)*. Decidere di chiudere un Paese intero, mentre migliaia di persone, giorno dopo giorno, perdevano la vita, non è stato semplice e credo che non lo sarebbe stato per nessuno, a prescindere dall'appartenenza politica. Ho letto qualche giorno fa dei dati diffusi dalla Fondazione Veronesi, elaborati da un *team* di epidemiologi dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità; dati che da scienziata, prima ancora che da senatrice, mi hanno davvero colpito: con le vaccinazioni contro il Covid e con riferimento all'arco temporale che va dalla fine del 2020 ad oggi abbiamo salvato un milione di vite umane in Europa. in Europa. *(Applausi)*. Parto da qui, perché credo sia utile ricordare cosa abbia significato la gestione di uno dei periodi più difficili della nostra storia: due milioni di morti e conseguenze enormi dal punto di vista economico, sociale e sanitario. Lo voglio ricordare, perché oggi sembra quasi scontato, ma una buona fetta di chi oggi chiede di istituire una Commissione sul Covid è la stessa che in quel periodo strizzava l'occhio ai no vax, giocava con le aperture le chiusure, soffiava sulle difficoltà. *(Applausi)*. Con quale credibilità queste forze politiche sentono di poter analizzare e verificare il lavoro svolto in quella fase così difficile? Mi chiedo davvero quale credibilità possano avere quelle forze politiche che passavano dall'apriamo al chiudiamo tutto, che hanno messo in discussione l'utilità dei piani vaccinali e la loro obbligatorietà. La butto lì: nessuna credibilità. Se ci fosse stato un tentativo diverso, se avessimo fatto lo sforzo di seguire quello che hanno fatto altri Paesi europei, forse avremmo avremmo svolto un servizio utile per la Nazione e ovviamente da questi banchi sarebbe arrivato un plauso. La differenza è netta: a livello internazionale dopo la pandemia di Covid-19 sono stati commissionati molti rapporti, con la finalità di analizzare quanto le decisioni politiche, scientifiche e di gestione siano state in grado di contrastare il disagio, prevenire le infezioni e salvare milioni di vite; un tentativo costruito non per per colpire chi si è assunto la responsabilità di gestire quella fase complicata, ma per capire cosa migliorare per permettere al proprio Paese di essere maggiormente attrezzato e pronto a prevenire e fronteggiare eventuali fenomeni simili in futuro. Il primo c'è stato nel maggio del 2021: è il rapporto del *panel* indipendente presieduto dall'ex primo ministro neozelandese Helen Clark, intitolato «Covid-19, far sì che sia l'ultima pandemia». A questo è seguito il rapporto della commissione paneuropea sulla salute e lo sviluppo sostenibile dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, intitolato «Trarre luce dalla pandemia». Poi ci sono stati i due rapporti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: «Costruire una ripresa resiliente, emergere più forti dalla pandemia di Covid-19», e poi ancora «Pronti per la prossima crisi? Investire in sistemi sanitari resilienti». Non leggo questi titoli a caso: li leggo perché rappresentano e sottolineano la profonda diversità di quelle commissioni rispetto a quella che volete istituire voi. Un tentativo simile è stato fatto e portato a termine dal Regno Unito; l'indagine è stata varata con un approccio terzo e con le forze politiche pronte a comprendere gli errori e le enormi falle. Lo stesso è accaduto in Svezia e uno sforzo simile l'ha fatto la Francia, la cui commissione ha individuato in maniera puntuale diversi impegni da rispettare, come ad esempio il coordinamento tra gli enti regionali territoriali e quelli sovraordinati. Per capirci, è ciò che da noi non ha funzionato, e penso chiaramente alla Lombardia. Non so se è chiara la differenza: da un lato, c'è la serietà delle istituzioni, che commissionano analisi e rapporti basati sul rigore scientifico, sulla terzietà dell'approccio metodologico, sulla multidisciplinarietà e multiprofessionalità dei partecipanti, con la volontà di comprendere gli errori e far sì che non si ripetano. C'è uno sguardo al futuro, all'esigenza di arrivare preparati in futuro. Dall'altro lato, c'è questo provvedimento, che sembra quasi un vestito cucito per indagare su questioni che oltretutto sono già state sollevate e chiuse dalla magistratura, che - come un abito su misura - tengono fuori dall'ambito di analisi alcune questioni; la più rilevante è quella delle Regioni, di cui hanno parlato già i miei colleghi. Mentre in Europa questa discussione diventa lo strumento per non commettere gli stessi errori, noi decidiamo ad esempio di ignorare gli errori commessi, che hanno determinato il decesso di tantissimi anziani nelle RSA. In pratica, mentre gli altri Paesi fanno un'indagine a tutto tondo, noi circoscriviamo circoscriviamo il nostro lavoro solo ad alcuni aspetti, lasciando fuori quelli che potrebbero essere scomodi per alcuni pezzi di questa maggioranza, ma che magari potrebbero farci capire che trascurare la sanità pubblica e la medicina territoriale per molte Regioni è stata una scelta sbagliata. E lo facciamo fare oltretutto a una Commissione con una maggioranza politica, come se

Mi dispiace doverlo dire anche ai colleghi di Italia Viva, che purtroppo non ci sono, ma che sentiranno sicuramente, i quali pure hanno condiviso, con profondo senso di responsabilità, le scelte assunte durante quella fase così complicata. Questa Commissione, così come è stata istituita, con le finalità che si si è data e con gli strumenti che intende darsi, assume un altro significato: essa è del tutto inutile, se non addirittura dannosa. Vede, Presidente, le ragioni per cui si decide di utilizzare strumentalmente lo strumento delle Commissioni di inchiesta rappresentano anche un pericoloso precedente. Temo che, se continueremo così, l'unica commissione che dovremo costituire sarà quella che indagherà per capire le ragioni che hanno portato al fallimento del Sistema sanitario pubblico italiano. Nei nostri ospedali mancano medici e infermieri; gli stipendi dei nostri operatori sanitari e le condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti non rendono giustizia al sacrificio quotidiano di tante donne e tanti uomini che esercitano queste professioni. Colleghi, se proprio dobbiamo usare il nostro tempo in una Commissione, vi faccio un accorato appello: usiamolo per salvare il nostro Sistema sanitario nazionale. Usiamo questo tempo per capire cosa non ha funzionato, cosa non sta funzionando e cosa potrebbe non funzionare nel caso in cui dovessimo essere nuovamente chiamati ad affrontare una pandemia. Usiamolo per evitare a milioni di cittadini di vedersi negata la tutela di un diritto fondamentale come il come il diritto alla salute. Dato che purtroppo non state facendo niente di tutto questo, concludo con le parole usate dal ministro Speranza, a cui sento di rivolgere un pensiero affettuoso: continuate pure su questa strada. Noi continueremo a servire il Paese nel rispetto della Costituzione e della scienza, con disciplina e onore.

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,

ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sanitario e soprattutto ha sconvolto tutte le nuove generazioni, colpendole nel cuore della loro vita, nel momento più importante di crescita. Una Commissione parlamentare d'inchiesta su questo tema potrebbe essere veramente lo strumento più utile e valido solo - e ripeto solo - laddove ricostruisse la storia nell'ottica di evitare in futuro eventuali criticità, e formulare raccomandazioni e prevenzione per il futuro. In particolare, dovrebbe indagare su due temi specifici:

Questi dovrebbero essere gli obiettivi principali di questa Commissione, che non dovrebbe utilizzata come uno strumento per individuare delle responsabilità, come clava contro le opposizioni, ma soprattutto come strumento per prevenire una futura emergenza. Io ho sentito tanti discorsi alla Camera e oggi ne sentirò tanti qui in Senato.

Io li invidio perché non hanno la minima idea del sacrificio umano, del peso di un legislatore durante una pandemia. Eppure si permettono di dire delle banalità atroci. Io li invidio perché non hanno dovuto cambiare la vita delle persone, delle nuove generazioni e non hanno dovuto incidere su quello che è successo in questo Paese. Io li invidio perché non hanno dovuto affrontare una pandemia con un Sistema sanitario che ha rischiato il collasso per quello che hanno causato i loro Governi precedenti. Io li invidio perché non hanno dovuto aiutare

tutte le Commissioni che hanno lavorato a creare il superbonus, uno strumento fondamentale che ha protetto e creato economia in un momento in cui il Paese era assolutamente chiuso. Ma qualcuno di voi era presente nella scorsa legislatura e, davanti all'appello del capo dello Stato Mattarella a un Governo di unità per salvare il Paese

«Criminale!». E adesso ce la troviamo in quest'Aula a chiedere toni pacati. In Romagna si dice «Mo sta bon, va

che hanno condiviso con noi la stessa responsabilità di quei giorni, una responsabilità gravissima, che abbiamo pagato tutti quanti insieme nelle urne. Quelle scelte difficili, per il bene del Paese, quelle scelte coraggiose andavano fatte e sappiamo in cuor nostro che andavano fatte, in larga parte, a tutela dei cittadini. È a voi che chiedo cosa state cercando e cosa state creando insieme agli altri in questa patetica caccia alle streghe, viste tutte le responsabilità che ci siamo assunti insieme. Questa Commissione ha soprattutto un perimetro ben specifico: ha evitato di toccare le Regioni e mi chiedo per quale motivo volete evitare di toccare le Regioni. Forse lo sappiamo: perché la maggior parte delle Regioni è amministrata da voi e quindi volete evitare di toccarle in questo momento. Dall'altra parte c'è un'ossessione, in questo Parlamento, che si chiama Giuseppe Conte e volete continuamente costruire dei perimetri intorno a lui per poterlo massacrare comunicativamente.

sulla pandemia e vi volete sostituire alla magistratura, perché quello che decide la magistratura non vi va bene, ma in magistrati vi volete trasformare. E allora buona caccia alle streghe, colleghi ratificatori. Mi piacerebbe chiamarvi così e non legislatori, perché avete trasformato questo Parlamento, in maniera vergognosa, in un mero posto di ratifiche. Si sta ratificando e basta. La gente fuori purtroppo non si rende conto di quello che state costruendo qua dentro, ma qui siamo diventati dei passacarte. Non vi va bene la magistratura e volete fare la magistratura e quello che dovreste fare - i legislatori - non lo fate. Questo Parlamento è diventato un posto di ratifiche, ne avete addirittura fatte due in un giorno, una doppia fiducia, nemmeno Van Basten faceva delle doppiette del genere. E allora buona caccia alle streghe a tutti i nemici che vi state costruendo e adesso ne avete trovato un altro, l'ennesimo.

Con questa Commissione avete creato l'ennesima caccia alle streghe in un Governo passato, quello Conte, mentre la Commissione avrebbe dovuto avere dei *focus* ben definiti e precisi, analizzare delle criticità che hanno portato all'emergenza Covid-19 al fine di individuare i punti deboli di questo Paese e del nostro sistema di prevenzione e dare delle risposte a un'eventuale emergenza sanitaria. Dall'altra parte, sarebbe stato necessario formulare delle raccomandazioni per implementare la preparazione nel nostro Paese, con un sistema sanitario che avrebbe potuto avere avere migliorie, soprattutto nel percorso intrapreso nelle emergenze. L'istituzione di una Commissione d'inchiesta è una cosa seria: questo Parlamento la chiede spesso,

Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, vorrei svolgere una riflessione sul tema che oggi discutiamo, cercando di spiegare come mai ritengo estremamente discutibile questo provvedimento. L'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Covid-19 su com'è stato affrontato nel nostro Paese non è di per sé una cosa sbagliata; lo è se si porta avanti questo progetto con intenti strumentali, a scopi di propaganda e - vorrei dirlo con molta chiarezza - anche con evidenti finalità di ripicca, se non di rappresaglia politica. Trovo che ciò sia estremamente sbagliato e non contribuirà a farci capire come possiamo rafforzare i nostri sistemi sanitari per essere più resilienti e resistenti, dovesse in futuro capitare una cosa simile a quella che è capitata tra il 2020 e il 2021. Non ci aiuterà nemmeno a capire bene l'origine delle singole mancanze che possono esserci state. Creerà soltanto un polverone, che non credo contribuirà a legittimare l'attività del Parlamento. Ho ascoltato ieri anche il dibattito che si è svolto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e l'ho ascoltato con un certo stupore, perché è stato fatto l'elenco delle tante Commissioni di inchiesta che in Parlamento si sono succedute, ma, a mio avviso, senza fare una precisazione. La precisazione da fare è la seguente e vorrei che i colleghi ponessero mente a questo: ci sono state, nella storia della nostra Repubblica, Commissioni di inchiesta che si sono rivelate utili, che sono servite a farci a farci capire meglio le origini e le modalità con cui certi fenomeni perversi si sono prodotti nel nostro Paese. Ci hanno aiutato per questa via, anche con gli interventi legislativi che a quelle Commissioni sono seguiti, contribuendo così a rafforzare gli anticorpi del Paese contro questi pericoli: penso, ad esempio, alla Commissione stragi, alla Commissione sulla P2 e a tante altre Commissioni che hanno avuto questa natura. Ci sono state, invece, Commissioni d'inchiesta che, come questa, sono nate su basi di propaganda e di strumentalizzazione e che non hanno reso, né ai cittadini, né al Parlamento, alcun servizio. Io sono fermamente convinto che questa Commissione d'inchiesta, per come la maggioranza, con l'aiuto di pezzi di opposizione,

Un'altra caratteristica di questo disegno di legge, che mi lascia estremamente perplesso, è che trovo sia un regalo,

strizza l'occhio ai ni vax, che sono portatori di colpe altrettanto gravi di quelle dei no vax. *(Applausi)*. Questo provvedimento strizza l'occhio a chi ha alimentato una narrazione complottista. Questo provvedimento va incontro a chi, se fosse stato ascoltato in quei momenti drammatici, avrebbe condotto il Paese in un vicolo cieco e in una situazione terrificante.

mentre si cercava di convincere la popolazione a vaccinarsi e a fare l'unica cosa possibile per sconfiggere la pandemia, alimentavano la narrazione ni vax, no vax e complottista. La vera Commissione d'inchiesta andrebbe fatta su questi aspetti. *(Applausi)*. Vi è poi un ulteriore elemento che mi lascia gravemente perplesso e sconcertato. Posso capire che un'iniziativa come questa se la intesti e la porti avanti chi, in quelle fasi, sedeva all'opposizione a demolire il lavoro di chi cercava di salvare gli italiani dalla pandemia. Non lo capisco molto, perché, quando si hanno responsabilità di Governo, si dovrebbero acquisire un altro modo di fare e un'altra cultura e si dovrebbe anche cercare di dimenticare i momenti più irresponsabili di quando si è stati all'opposizione. Se però questo tipo di

ma può essere politicamente comprensibile. Che si associno però a un'iniziativa del genere una serie di forze politiche che in quel momento stavano al Governo

io credo che l'Italia abbia attraversato quella fase in maniera seria, perché serio è stato il comportamento delle istituzioni e seria è stata la risposta dei cittadini. Mi domando, però, se così stanno le cose: una Commissione di inchiesta che nasce con scopi di infangamento così plateali quale servizio rende al Paese? Quale alta finalità realizza? Quale scopo giustificabile si prefigge? Nessuno. Servirà soltanto a spaccare l'opinione pubblica, ad avvelenare il dibattito tra le forze politiche e soprattutto a farci capire, ancora una volta, che una Commissione d'inchiesta pensata e attuata come un plotone d'esecuzione contro gli avversari politici è un'iniziativa politicamente malsana, sbagliata e da condannare con grande fermezza.

Non userò giri di parole, Presidente, per definire questo provvedimento un vero e proprio schiaffo dato in pieno volto non solo alla verità dei fatti - prima di tutto ai

anche all'intero sistema Paese che in quel periodo ha sofferto una pandemia mai vista prima. Dovremmo tutti ricordarci quali sono stati gli stenti di tutti gli italiani in quel periodo. La pandemia è stata contrastata dal Governo a guida Giuseppe Conte nel migliore dei modi possibili, lasciatemelo dire e confermare in questa seduta. È proprio questo che a voi, signori della maggioranza, non sta bene e non sta bene nemmeno a qualche altro vostro spasimante politico. Come noto, solo invidia e gelosia innaffiano un ormai appassito giglio magico e la frase «ho fatto fuori Giuseppe Conte da Palazzo Chigi»

ha le prove di qualcosa andato storto, tanto da gridare al complotto messo in atto da Giuseppe Conte con i russi o a favore addirittura dei russi, le tiri fuori, altrimenti non si può che constatare che alcune persone vengono qui a parlare di fuffa, di aria fritta.

Questa maggioranza e questo Governo impegnano il Parlamento con il testo in esame in una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica e sulle misure adottate in quel periodo. Perfetto. Il problema sono il modo e la maniera singolare con cui lo fa. Lo fa a proprio esclusivo uso e consumo. La cosa non stupisce, visto che, di fatto, questa maggioranza e questo Governo hanno eletto a prassi e metodo la mortificazione delle due Camere. È una questione per per me fondante. Lo so, lo ripeto spesse volte in Aula e lo faccio anche in Commissione, ma è chiaro che per me è un elemento fondante. Per voi la rappresentanza parlamentare ha senso solo se espressione della vostra volontà; in caso contrario, è un mero fastidio e certamente non tenete in considerazione che la rappresentanza parlamentare è uno dei punti fondanti della nostra democrazia *(Applausi)*, cosa che dovreste invece ben tenere a mente nel caso in cui lo faceste, smetterei di ripetere queste cose). Queste mie affermazioni trovano conferma nell'indegno e pericoloso disegno di riforma che avete approvato di recente. Certo, perché non vi bastava più una madre cristiana, avevate bisogno di una madre delle riforme per continuare la vostra opera di distrazione e gettare le basi di una inquietante dittatura democratica. Non è però un caso il mio accenno alla Carta costituzionale, e questo perché è proprio la nostra Carta a definire la competenza concorrente in materia di di sanità, ovvero lo Stato detta i princìpi generali e le Regioni poi sono chiamate a legiferare sulla sanità. È proprio in questo contesto che vi siete sinceramente superati, mettendo in luce tutti i vostri volti diversi e gli evidenti contrasti, che sono la sintesi del vostro modo di stare insieme e della vostra coalizione, che poi estrinsecano l'idea del Paese che avete. Da un lato, rincorrete un'irrinunciabile legge sull'autonomia e, nello stesso tempo, lì dove a legislazione vigente vi è una seppur minima autonomia in in ambito regionale, considerate bene l'idea di tenere fuori le Regioni da questo testo di legge. Anche questo è normale, anche perché mi sembra di intendere che i partiti di destra non sbagliano mai e la colpa è sempre degli altri. E se qualcuno vi fa notare le vostre tantissime mancanze, allora è il momento che parte l'urlo al complotto, calate il guscio sul capo e vi impegnate in un improbabile coro di esaltazione della politica di Calimero, cioè la vostra. Proprio voi, i forti, potenti, competenti e pronti combattenti sovranisti, con questo testo impegnate le risorse dei contribuenti in una Commissione che parte già monca e che, come dicevo, a poco servirà nell'accertamento della realtà, della verità dei fatti e delle responsabilità. Altra perla che viene riportata nel testo - la cito testualmente - è quella che dice di indagare e verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia. Signori, che mancanza di fantasia. Potevate proporre - magari qualcuno di voi lo ha anche pensato - l'eliminazione della *pochette* da taschino come inutile orpello di eleganza, per sostituirla con una comoda felpa da comizio. Ma è è proprio l'abbinamento tra voi e i reali bisogni del Paese che non riuscite a fare, e questo provvedimento ne è l'ennesima prova. La verità è che questa Commissione nasce con un unico, malcelato e pertanto palese obiettivo, obiettivo, ossia colpire Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio che in quel periodo si è permesso non solo di contrastare la pandemia nel modo migliore, ma anche di mettervi di fronte alle vostre responsabilità. *(Applausi)*. Colleghi, chi chi è che l'ha dimenticato? Di certo non noi, di certo non il popolo; la gente fuori da queste Aule non dimentica come vi siete comportati in quei mesi: aprite; no, chiudete; bisogna aprire; chiudiamo un po', lasciamo un po' accostato. Un gran caos avete generato. *(Applausi)*. E poi non avete dimenticato di strizzare l'occhio ai no vax, certo, perché anche quelli votano. E perché no, visto che non governavate voi, promesso 1.000 euro a ognuno. Quello è stato un periodo veramente dannato, anche per le vostre sconsideratezze. Evidentemente, quelle figure ancora oggi pesano sulle vostre teste. Signor Presidente, concludo questo mio intervento con un briciolo di speranza e cioè con l'auspicio che in futuro non si debba più assistere alla trascrizione nei disegni di legge della voglia di rivalsa di una maggioranza politica nei confronti di un'altra maggioranza che li ha preceduti alla guida del Paese. Colleghi della maggioranza, non avete fatto nulla, se non urlare e straparlare in quel brutto periodo. Oggi invece chiedete conto dell'operato di chi ha guidato il Paese in uno dei suoi momenti più bui. Giuseppe Conte non ha nulla da temere; il MoVimento 5 Stelle non ha nulla da temere davanti a voi. A quei tempi la vostra a voi. A quei tempi la vostra irresponsabilità generò sgomento e preoccupazione. Oggi le vostre scelte destano tristezza e confermano la siderale distanza che c'è tra voi, le che c'è tra voi, le vostre azioni, il vostro modo di intendere la politica, il vostro modo di intendere il potere decisionale e tutto il resto del Paese. *(Applausi)*.

a parlare. Rimango un po' perplesso quando sento interventi come quelli di alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto. che mi hanno preceduto. Non voglio risalire come un salmone a tutte le cose che sono state dette, ma rimango alle ultime parole della senatrice Di Girolamo,

moralmente obbligati a non votare gli obblighi vaccinali, perché era inserito nel loro programma elettorale e questo era il MoVimento 5 Stelle. Eppure erano lì in prima fila a votare ogni tipo di obbligo, anche quello più strano, e noi cercavamo in qualche maniera di ragionare, forse qualcuno si ricorda, abbiamo anche votato contro in Commissione con grande fatica e ci è costato anche molto in termini elettorali questo voler voler rimanere in ogni caso fedeli alla maggioranza. Che sia però il MoVimento 5 Stelle a dirci che strizzavano l'occhio ai no vax, quando erano tutti eletti con un programma che diceva «nessun obbligo vaccinale», mi sembra veramente curioso. Anche in questo caso

sono interessato a vedere che cosa c'è. Sono interessato anche a vedere quali siano state le motivazioni di certe scelte, perché sembra di sentire che le scelte del Governo italiano, segnatamente quello guidato inizialmente da Giuseppe Conte, abbiano salvato l'Italia. Non mi risulta di vedere alcun tipo di metrica tale per cui l'Italia ha fatto meglio di qualsiasi altro Paese al mondo, da nessuna parte. In compenso, sono state prese decisioni senza precedenti e a me interesserebbe capire cosa le abbia originate o le abbia spinte. Perché prendere e chiudere di botto tutto un Paese, senza precedenti di altri Paesi, che non fossero la Cina? Anche in tal caso, forse qualche ispirazione da parte dei cinesi è arrivata, ma allora lo voglio sapere. Invece, è stato fatto con la massima leggerezza. Come e perché, quando altri prendevano decisioni differenti, mi interessa saperlo, mi interessa saperlo, perché da quelle decisioni è cominciato a discendere ogni tipo di cosa. Quando i nostri nipoti sapranno cosa è successo in quegli anni si metteranno abbastanza a ridere: gli inseguimenti dei *runner* sulla spiaggia, i droni per evitare le grigliate di Pasqua, i vecchietti che dovevano prendere il cane finto

Poi uno dice: sì, parli *ex post*. Magari parlo *ex post*, senza dubbio; ma io ho un'abitudine tale per cui, quando uno ha una responsabilità, dopo, se certe cose erano sbagliate, le responsabilità forse vanno mantenute. È comodo dire: vabbè, ma non si sapeva. Non si sapeva, ma c'erano dei dati. Volete sapere un motivo, uno solo, tale per cui questa Commissione d'inchiesta va fatta? Molto semplice: il ministro Speranza all'epoca aveva un solo obbligo nei confronti del Parlamento, che tanto era un'apposizione in quel periodo. Per chi parla di dittatura democratica, il Parlamento all'epoca era un'apposizione. Il ministro Speranza aveva un solo obbligo: quello di rispondere alle interrogazioni dei deputati. Io ne ho fatte quattordici. Risposte del ministro Speranza: zero. Non ha risposto a niente, neanche a una. Io avevo detto: bene, se il Ministro non mi risponde con le buone, mi risponderà per altri modi. E sarò molto lieto di avere di fronte a me, davanti a una Commissione di inchiesta con i poteri della magistratura, l'ex ministro Speranza, per chiedergli tutto quello che non ha voluto dirmi

e anche come la collaborazione tra le forze politiche sia stata fondamentale per affrontare uno dei periodi più bui della storia repubblicana. È indubbio che la pandemia abbia rappresentato una delle sfide più difficili che abbiamo dovuto affrontare come Nazione, richiedendo una risposta rapida, efficace e coordinata da parte delle istituzioni. Ebbene, però, spiace constatare e leggere nei pilastri fondativi che sorreggono l'istituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2 un'unica e chiara intenzione, quella di delegittimare l'operato e le misure messe in campo dal Governo Conte per affrontare un'emergenza che ha profondamente lacerato il nostro Paese. La verità è che questa maggioranza sta portando avanti una becera propaganda, che infanga la memoria di chi, per colpa di questo maledetto virus, non è più tra noi. La verità è anche un'altra, Presidente: quell'Esecutivo ha adottato in tempi *record*, cogliendo il plauso dei principali Stati mondiali, una serie di provvedimenti che di fatto hanno messo in sicurezza il nostro Paese, tutelando la salute dei nostri concittadini, preservando la sicurezza del sistema sanitario e mitigando l'impatto economico che in altre parti del mondo ha incrementato come non mai la sperequazione economica tra le diverse classi sociali. Non spetta certo a me ricordare che siamo stati i primi sul pianeta Terra a disporre la chiusura delle scuole, a istituire una quarantena nazionale per limitare la diffusione del virus, a monitorare attentamente la situazione epidemiologica e a prendere decisioni basate sulle evidenze scientifiche e sulle raccomandazioni degli esperti sanitari riuniti in seno a un comitato tecnico-scientifico. Queste decisioni non sono state facili, ma si sono rivelate necessarie per prevenire un'ulteriore *escalation* dei contagi e proteggere i più vulnerabili. Non spetta certo a me ricordare che il Governo Conte ha potenziato il sistema sanitario, incrementando il numero dei posti letto nelle terapie intensive, fornendo dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari e aumentando la capacità di effettuare tamponi e test diagnostici. E non spetta certo a me ricordare l'impegno del Governo Conte per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, amplificate dalla pandemia, attraverso politiche di inclusione sociale e assistenza adeguata ai più vulnerabili. modo, Presidente, non spetta certo a me ricordare le ingenti misure di sostegno per il reddito di cittadinanza, che il Governo Meloni ha smantellato. Erano più che probabili forti tensioni e disordini sociali. Onorevoli colleghi della maggioranza, vi siete chiesti perché il nostro capo politico istituì un coordinamento tra le Regioni e il Governo centrale per garantire un'allocazione equa delle risorse e gestire efficacemente l'emergenza in tutto il territorio nazionale? Ve lo spiego io: questa decisione fu dovuta per correre ai ripari dalla scellerata riforma del Titolo V della Costituzione, che ha frammentato la gestione della materia sanitaria in tanti centri decisionali quante sono le Regioni italiane e ciò dimostra il pericolo del progetto autonomista che inconsciamente state portando avanti. Tuttavia, la decisione di coordinare l'emergenza è stata anche la diretta conseguenza dell'incapacità politica e amministrativa di alcune Regioni. Presidente, è stato già detto, ma mi riferisco a due Regioni in particolare, la Lombardia e il Piemonte, tra le più colpite dalla diffusione del virus. Pertanto chiedo ai colleghi della maggioranza perché tra i compiti di questa Commissione d'inchiesta non abbiano previsto anche la valutazione dell'operato gestionale di queste due Regioni. facile e ve la dico io: perché queste Regioni erano e sono governate dal centrodestra. Onorevoli colleghi, la pandemia è stata un duro colpo per il nostro Paese, ma abbiamo dimostrato resilienza e capacità di adattamento. Il Governo Conte ha messo in campo misure importanti per affrontare questa emergenza, ma la sfida non è ancora terminata. Ebbene, dobbiamo essere consapevoli che l'emergenza da Covid-19 non è ancora completamente risolta e che dobbiamo rimanere vigili e pronti a far fronte ad eventuali nuove sfide. Per questo, signora Presidente, più che dedicare tempo, risorse ed energie per finalità propagandistiche, da questo Esecutivo mi sarei aspettato un impegno rapido e concreto per rafforzare il sistema sanitario, migliorare la pianificazione e la prevenzione delle future emergenze e promuovere una maggiore cooperazione internazionale. Evidentemente, però, il vostro unico obiettivo era e rimane solo quello di alimentare quotidianamente la vostra macchina della propaganda, insultando la dignità di 60 milioni di italiani, ma noi non ve lo consentiremo. *(Applausi)*.

potremmo renderci conto che in realtà il Covid ha profondamente mutato molte delle convinzioni che avevamo e forse bisognerebbe proprio provare a ragionare di questo. Provo a raccontarvelo dal punto di vista del lavoro, a partire dalla data del 25 marzo del 2020, quando in Lombardia le aziende metalmeccaniche e chimiche scioperarono per chiedere norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quella Regione, nonostante Codogno, nonostante si avesse la certezza che si stava diffondendo il virus, continuava a dire che bisognava correre, essere sui luoghi di lavoro e non avere paura della malattia.

che una delle cose che avrebbe fatto dannosamente il Governo in quel periodo era stato sancire che il contagio da Covid era infortunio, vi pregherei, colleghi, di non tornare indietro di secoli, perché contagiarsi sul luogo di lavoro è infortunio, non è vero che non lo è ed anzi è norma di civiltà riconoscerlo. *(Applausi)*. Allora avevamo un problema e bisogna interrogarsi anche su questo: quelli che non potevano andare a casa e trasferire lì la loro postazione di lavoro. Anche di questo dovremmo parlare molto, perché le evoluzioni del lavoro e il cambiamento tecnologico inducono possibilità infinite che non si possono non affrontare provando a ragionare su quali conseguenze hanno avuto, su cosa hanno determinato diversamente per uomini e donne e su quello che hanno proposto, anche in termini di protocolli sulla salute, che magari sono facili da fare in un grande luogo e molto più complessi nei piccoli luoghi di lavoro o negli ambienti più ristretti.

Pensate davvero che bastino un processo o un'inquisizione per sapere come si determina la sicurezza delle persone? Oppure proviamo a domandarci come mai abbiamo scoperto, perché eravamo chiusi nelle case o con le norme - per fortuna - di sicurezza nei luoghi di lavoro, che esiste di lavoro, che esiste un grande mondo del lavoro del tutto ignoto: le lavoratrici delle imprese di pulizia, i lavoratori che andavano fuori dai supermercati per prendere la spesa e per portarla nelle case, quelli che si occupavano della logistica, quelli che si occupavano delle disinfezioni o quelli che si occupavano della nostra sicurezza e che noi non avevamo mai visto. Quelle persone sono spesso precarie per condizioni di lavoro, in appalto, con poche ore di lavoro e con basse retribuzioni, e sono quelle che nel nostro sentire collettivo e in quella strana gerarchia del valore dei lavori che utilizziamo valgono poco e stanno in fondo alla scala, perché prima ci sono coloro che generano profitto rapido e distribuzione di risultati importanti per le imprese. Eppure è a loro che dobbiamo la nostra vita, a quella commessa del mio supermercato che ben conosco da tanti anni, che mi diceva di avere paura, perché le persone andavano lì senza mascherina, senza stare dietro al vetro, pretendendo di toccare

e l'idea che tutto sia dovuto è invece la dimensione della cura. Dove sta tutto questo nella nostra scala di valori? Vogliamo provare a ragionarne? Come ragioniamo su quale sia il *welfare* di prossimità, se non ci domandiamo com'è l'organizzazione sociosanitaria nel territorio e che effetto ha il lavoro collettivo rispetto a tutto questo? Potremmo domandarci - lo hanno già detto altri colleghi e colleghe - cos'è successo nelle residenze sanitarie per gli anziani

E allora possiamo ricordare una cosa che sarebbe essenziale, che abbiamo scoperto in quei mesi: la malattia non è un fatto individuale, ma drammaticamente collettivo e i comportamenti intorno sono quelli che decidono anche della nostra possibilità di essere sani e di andare avanti. avanti. Discutere di tutto questo vuol dire pensare alla nostra struttura del lavoro, alla nostra struttura del *welfare*, a quali risposte abbiamo, al fatto che la sanità non è solo cura della malattia, dai comportamenti che abbiamo e da come si determinano. *(Applausi)*. Di tutto questo sarebbe straordinariamente importante parlare e invece siamo di fronte a una proposta che è una Commissione, come ci ha appena detto il senatore Claudio la Commissione d'inchiesta, per sostituirsi alla magistratura, a quella nazionale e anche a quella internazionale, visto che vogliamo fare il processo anche all'Organizzazione proposta. Vorrei dire che non è vigliaccheria non volere una Commissione fatta così, ma è rispetto del Parlamento e della sua funzione; è alzare l'ambizione che dobbiamo dare alle Commissioni di inchiesta, che hanno il valore di pensare al futuro e a che cosa dobbiamo fare. Questo perché noi - badate bene - una responsabilità ce l'abbiamo ed è quella di dare la necessaria fiducia al Paese di fronte ai grandi cambiamenti, da quelli climatici a quelli che riguardano la salute. Come Parlamento lavoriamo per attrezzarci per riconoscere il loro lavoro, per valorizzare in positivo le cose che abbiamo imparato durante la pandemia, situazioni non si ripetano e per provare a far avanzare complessivamente la società. Invece, non vogliamo dare questo al Paese; non vogliamo dare un elemento di speranza e di futuro rispetto alle lacerazioni che ci sono state e alla paura che c'era. Vogliamo continuare ad agitare quella paura. Vogliamo continuare a dire che, anziché anziché una straordinaria fatica per sperimentare e provare a curare le persone e a salvare vite umane, abbiamo fatto chissà quali nefandezze. Ma chi voleva rivolgersi alla magistratura ci si è già rivolto e io penso che la magistratura giustamente debba indagare. Ciò che credo sia, invece, un grande svilimento della politica è pensare che noi siamo una magistratura dopo la magistratura e che, invece di domandarci come far funzionare il sistema sanitario nazionale e come far funzionare il *welfare* di prossimità, ci domandiamo come diventare tutti giudici incompetenti e non laureati. E come si fa a fare tutto questo senza parlare delle Regioni? Io non ho denunciato il Presidente della regione Lombardia. Non penso che sarebbe giusto, ma non dimentico:

vorrei parlare del perché, nel rapporto tra pubblico e privato, in Lombardia noi non abbiamo più la sanità pubblica e non siamo in grado di curarci. Lo abbiamo visto durante il Covid-19. Io vorrei sapere perché i miei coetanei, coetanei, i miei colleghi di lavoro, della stessa fascia d'anzianità, quelli che avevano diritto al vaccino fin dall'inizio, in Lombardia hanno potuto vaccinarsi quattro mesi prima di me; e perché è dovuto arrivare il generale Figliuolo in Lombardia perché le vaccinazioni tornassero nelle regole nazionali e si determinassero. Io penso, però, che non serva fare questo processo lo dico anche contro il mio interesse e contro l'interesse della mia parte politica. Non mi interessa fare la classifica di quelli che hanno fatto bene o hanno fatto male, perché penso che tutti abbiamo in qualche modo fatto gli apprendisti di una situazione di grande difficoltà. In conclusione, signor Presidente, vorrei dire

che ventuno sistemi sanitari non funzionano, che il rapporto col privato va ripensato, che curare chi è in difficoltà è un onere che il Paese deve sempre sostenere. Questa servirebbe come risposta, perché altrimenti

Possiamo fare tutto questo, laddove vorrei ricordassimo che, invece, la grande lezione del Covid-19 è che la malattia non è solo una questione individuale, ma collettiva e sociale.

con i suoi sette milioni di morti, l'economia in ginocchio, gli ingenti danni sociali, la pandemia è stata la più grande catastrofe che il mondo ha vissuto dalla Seconda guerra mondiale. Da eventi così radicali, non si esce mai uguali a prima. La pandemia ci ha insegnato ad avere più rispetto della scienza e del metodo scientifico, ci ha ricordato il valore inestimabile della sanità pubblica e della medicina territoriale di base, della necessità di modificare il modello di sviluppo avendo più rispetto degli equilibri naturali, dell'importanza di combattere la disinformazione e le false notizie. Oggi una Commissione d'inchiesta sul Covid-19 dovrebbe occuparsi di queste cose. Dovrebbe, cioè, aiutare il decisore politico a costruire politiche più efficaci nella gestione delle emergenze e per rimuovere le cause che possono portare all'insorgenza di nuove pandemie. Una Commissione, cioè, che voglia valorizzare la lezione di questi anni, proiettandola a beneficio dell'interesse generale. Invece, questa Commissione, per come si prefigura, per i compiti che si attribuisce e per quelli che non si attribuisce, a tutto risponde tranne che a questa finalità. È una Commissione che guarda indietro, alla ricerca di chissà quali negligenze e responsabilità, rimuovendo completamente dal tappeto la gravità di quei giorni, il fatto che si fosse davanti ad un evento senza precedenti e che non esistevano strumenti concreti per fronteggiarlo. Quegli strumenti sono stati costruiti strada facendo in parallelo alle indicazioni che via via venivano dalla scienza, impegnata nello studio della malattia. L'idea di chiudere, ad esempio, fu consequenziale alla scoperta della facilità di propagazione del virus. Il ricorso alle mascherine e la differenziazione tra luoghi chiusi e aperti fu legata alla scoperta che il virus in determinate condizioni aveva meno facilità di attecchire. Si potrebbe continuare ancora dal *green* *pass* al ruolo svolto dai vaccini, il tema della loro efficacia, le soglie critiche rispetto al numero di posti delle terapie intensive, l'andamento della campagna vaccinale e così via. Fare un processo a tutto questo, a chi ha avuto compiti di responsabilità è un atto ingeneroso anche nei confronti dell'unità nazionale di quelle settimane che tutti invece dovremmo conservare come una delle pagine più preziose della storia d'Italia. Utilizzare una Commissione parlamentare per riscrivere *ex post* la storia o peggio ancora per usarla come arma di rappresaglia verso gli avversari politici è qualcosa di inaccettabile. Questa riscrittura della storia, si tratti di quella lontana o anche di quella più recente, è soltanto funzionale ad una destra smaniosa di affrancare il Paese dalla presunta egemonia culturale della sinistra. Peccato che nel farlo si compiono due errori madornali. Il primo è nell'attribuire al pensiero di sinistra qualsiasi convinzione sia maturata in questo Paese negli ultimi dieci anni, come se fosse stata possibile una versione alternativa di gestione della pandemia a quella gradualmente costruita attorno alla scienza, al principio di massima precauzione per la salute pubblica e alla tutela dell'interesse generale. Il secondo è nel piegare le Istituzioni, nella fattispecie lo strumento della Commissione parlamentare d'inchiesta, al servizio di un bisogno tutto politico. Questa Commissione crea un pericoloso precedente e determina un potere parallelo, un contropotere giudiziario su decisioni politiche, come lo ha chiamato il Presidente della Repubblica, al di fuori dei precetti e delle funzioni costituzionali. Allora quella di oggi potrebbe essere una cattiva giornata per questo Senato e per tutte le Istituzioni, per tutti i lavoratori che durante la pandemia hanno continuato a lavorare - io sono uno di questi - per far funzionare il Paese e purtroppo anche per i lavoratori, soprattutto della sanità o delle case di riposo, che sono morti nell'adempimento del dovere, anche e soprattutto per salvare la vita degli altri.

Signor Presidente, non dovevo intervenire oggi, mi sono fatta aggiungere, come potete vedere dall'elenco, e vi devo dire che mi è arrivato un pugno nello stomaco. Per voi infatti questo è un provvedimento forse come tanti altri, per me no. Ricordo che vengo da Bergamo, che faccio il sindaco e che ero sindaco durante il Covid. Ascoltare oggi gli interventi, alcuni molto profondi, altri meno, alcuni forse troppo politici parlando di una pandemia, altri un po' più umani, ho rivissuto i periodi più tragici della mia vita e di quella di tante persone della mia zona, di Bergamo, ma non solo. Qua non siamo a me contro te, stiamo parlando di migliaia e migliaia di morti e di persone, tra cui anche la

da dove è partita l'idea e lo *slogan* «chiudere tutto»? Qualcuno in quest'Aula che allora aveva anche ruoli di Governo lo sa. Da noi sindaci di Bergamo. «Chiudere tutto» ce lo siamo inventato noi: siamo noi che abbiamo cercato di convincere il Governo a chiudere tutto.

ne sono passati due o forse anche meno, se contiamo tutti i *lockdown* che ci sono stati. Non so, ho perso anche un po' la cognizione del tempo dal Covid in poi. Ma è bene che se ne parli e grazie a questa Commissione si potrà far luce su tante cose che non hanno funzionato. Ciò deve servire non per fare un processo a quello che ormai è successo, perché i morti sono morti e la gente che piange ancora i propri cari l'abbiamo sparsa su tutto il territorio nazionale (un po' più da noi forse). Quindi su quello non possiamo farci assolutamente niente, ma noi siamo politici, siamo responsabilità di fare in modo che, se dovesse accadere qualcosa di simile in futuro, non si svolga più nello stesso modo, non ci siano più così tante carenze, così tanti errori e tanto pressappochismo. Sì, era una cosa inaspettata, però vi assicuro come sapete ormai - che da noi non abbiamo aspettato i DPCM per chiudere tutto. È la gente che da sola ha chiuso fabbriche, negozi, attività, qualsiasi cosa. Quindi non abbiamo aspettato nessuno per chiudere. Di certo si faceva fatica si faceva fatica a interpretare alcuni provvedimenti sul territorio; c'erano le FAQ, c'era l'interpretazione autentica di testi di legge: delle cose folli; vi assicuro che è stata una follia. Quindi sì, gli errori sono stati fatti. Sicuramente ci sarà qualcuno sul territorio nazionale che magari ci ha anche guadagnato. Non parlo del Governo, di chi è qui presente o di chi c'era prima. Parlo in generale, perché quando ci sono queste tragedie sicuramente c'è qualcuno che specula; succede sempre, succede con le guerre e sta succedendo adesso con le guerre più o meno più o meno lontane nel mondo. Quindi figuriamoci se nessuno ha guadagnato con una pandemia. Però questa Commissione è sicuramente utile per dipanare alcuni dubbi e anche per rassicurare chi non ha creduto fino in fondo che fosse la strada giusta da seguire. Non è stata giusta per ogni aspetto, ma secondo me qualcosa di buono è stato fatto a diversi livelli di governo. Io sono lombarda, come sapete, e anche lì c'è un me contro te oggi, perché vogliamo la Commissione per far luce sulle carenze solo del Governo, ma ricordo anche quando c'erano degli attacchi folli contro le nostre Regioni, che in quei momenti stavano vivendo un dramma. Quindi credo che le colpe ci siano state, nei vari passaggi fra maggioranze e minoranze, un po' dappertutto, chi più chi meno. Vorrei solo dirvi che serve rispetto soprattutto per la gente di Bergamo, ma non solo, per tutte le vittime, per chi ha visto la propria vita stravolta, per chi continua a vivere senza più grande entusiasmo perché non riesce a uscire da questo vortice di disperazione e di tristezza.

prossimo sabato sono invitata ad Alzano Lombardo perché verrà inaugurata la fontana della comunità, un monumento che celebra la virtù della fortezza e la centralità dell'impegno civico nella comunità alzanese, che è la cosa più importante

è nato un comitato, sono stati coinvolti gli alpini, la protezione civile, la proloco e sono state coinvolte altre 23 associazioni e fondazioni. La fontana è stata pagata completamente da privati, aziende, società, associazioni, da tutto il mondo del volontariato che si è riunito dopo il grande lavoro che avevano fatto assieme durante l'emergenza. Questa fontana ha un suo significato perché rappresenta tre temi principali: la vulnerabilità della vita, riconducibile all'anziano; la fortezza, la tenacia e il vigore rappresentate dall'età adulta (virtù delle quali dovremmo dare esempio al popolo italiano visto che siamo tutti adulti) e la speranza, il futuro, la generazione di vita propria dell'età giovanile. I tre temi

una fontana è una cosa, ma racchiude tutto un mondo e penso che questa Commissione debba servirci anche per un altro obiettivo: ricordarci, ogni volta che parliamo del Covid, con tutti gli errori che sono stati fatti da tutte le parti, che abbiamo una risorsa fondamentale in questo Paese che stiamo tornando a dimenticare: le nostre comunità locali, i nostri piccoli Comuni, le nostre associazioni e tutto il mondo incredibile del volontariato. L'unico modo per far funzionare questo Paese, sia nelle difficoltà che in tempi di pace, è quello di ricordarci di valorizzare i territori, perché da soli, abbandonati a loro stessi, grazie all'aiuto dei cittadini hanno saputo andare avanti e sopravvivere. che questa Commissione venga affrontata con grande rispetto da tutte le parti, perché parliamo della gente e soprattutto della mia gente. Auguro buon lavoro a chi ne farà parte e ricordo anche che le rinunce non sono tutte uguali: rinunciare a un affetto, rinunciare a un amore, rinunciare a un pezzo di vita non è di certo come dover rinunciare a un corso sportivo.

Italia Viva, com'è stato detto anche nella giornata di ieri dal senatore Renzi, è stato il primo partito a chiedere l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul Covid già nel 2020, nel 2021 e nel 2022 abbiamo anche lanciato una petizione. Oggi devo dire che mi dispiace ascoltare alcuni interventi e apprendere dalle agenzie il dietrofront di alcuni colleghi di Azione, che hanno cambiato idea sull'istituzione della Commissione Covid dopo averla sostenuta fortemente con noi anche qualche settimana fa alla Camera. Per carità, si può anche cambiare idea, ma c'è un un discorso di coerenza politica che forse dovrebbe essere portato avanti, almeno nelle Aule parlamentari. Questa Commissione - lo ha detto bene il senatore Renzi anche nella giornata di ieri non vuole essere un tribunale politico nella maniera più assoluta, perché noi rispettiamo il lavoro che faranno la magistratura e la procura e quello per noi è un percorso che non riguarda il lavoro parlamentare. Oggi invece vogliamo parlare del merito di questa Commissione, di cosa si dovrà occupare questa Commissione. Ricordo anche che il testo è stato modificato nel passaggio dalla Camera al Senato noi come Italia Viva avevamo presentato un emendamento che chiedeva di estendere la Commissione di inchiesta anche alle Regioni, com'è giusto che sia, ma questo emendamento purtroppo è stato bocciato dalla maggioranza nelle Commissioni competenti. Ovviamente noi oggi questo emendamento lo ripresentiamo in Aula, insieme a tutti gli altri emendamenti che saranno discussi. Ciò non toglie il valore di questa Commissione, che avremmo preferito sicuramente migliore rispetto al testo attuale, ma questo non significa non affrontare il tema. Significa per noi invece parlare di ciò che non ha funzionato; su questo vogliamo fare chiarezza. Non cadiamo nella provocazione facile e mediatica della propaganda, perché non vogliamo generare confusione, come si sta cercando di fare in questi giorni, anche dalle agenzie di questa mattina. Ma allora, se restiamo nel merito e vogliamo parlare di ciò che non ha funzionato, perché avete paura, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle? Perché dovete avere paura della verità? Questo è quello che noi non comprendiamo. Questa è la differenza tra il populismo, la propaganda e il riformismo: i riformisti sono quelli che hanno il coraggio di portare avanti la verità. E noi vogliamo parlare di questo, soltanto della verità, perché saremo sempre dalla parte della scienza e dei vaccini, come abbiamo sempre fatto, e non strizzeremo mai l'occhio ai no vax, come invece è stato fatto

da colleghi della maggioranza, che hanno strizzato l'occhio ai no vax. Noi, come Italia Viva, siamo stati sempre molto chiari, perché la serietà della politica è anche questa. Riguardo poi

Ne approfitto per ringraziare questa mattina in Aula gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, le Forze dell'ordine, tutti gli operatori e tutti i volontari che hanno cercato di evitare un'ulteriore catastrofe, che in quei giorni erano definiti eroi e che poi da alcuni sono stati completamente abbandonati. Vogliamo parlare di questo, dei banchi a rotelle, vogliamo parlare delle cosiddette primule, vogliamo parlare di tutto quello che non ha funzionato e vorremmo capire perché chiudere in quel periodo le scuole, per esempio, e quali criteri sono stati utilizzati, soprattutto a danno dei più deboli e dei più fragili. Penso alle persone con disabilità, ma penso anche ai bambini, ai ragazzi - lo dico da genitore e da madre - e agli anziani.

in termini sociali e sanitari. Guardate all'aumento che c'è stato, dopo il Covid, del disagio giovanile, del disagio mentale, della solitudine degli anziani e delle persone fragili. quindi verificare i pro e contro e cosa era giusto fare. Nessuno ha la verità in tasca e nessuno vuole fare un processo politico alle singole persone (questo lo voglio ribadire). Ma vogliamo fare chiarezza, perché gli errori che sono stati fatti in quella fase non si debbano più ripetere. Questo è il punto e questo è anche il senso che vogliamo dare oggi all'istituzione della Commissione;

non diamo un segnale di fronte al Paese di quello che è accaduto? Guardiamolo anche dal punto di vista economico e sociale e pensiamo a cosa ha voluto dire chiudere un intero Paese. È possibile che non riusciamo a vedere i lati negativi e positivi di quello che è stato fatto e di quello che forse andava a fatto? Signor Presidente, desidero concludere il mio intervento aggiungendo un argomento che a noi sta molto a cuore, proprio perché parliamo di sanità, di sociale, di persone e di famiglie che non ci sono più e di persone che si sono ammalate di Covid. I temi della sanità rimangono tutti qui e purtroppo non li risolverà la manovra finanziaria, che darà soltanto delle briciole, solo tre miliardi di euro alla sanità. Su questo mi appello al Sottosegretario, al Governo, ai colleghi di maggioranza, per fare in modo di trovare maggiori risorse per la sanità,

tempo a prendere le risorse del MES sanitario, quei 37 miliardi che avrebbero davvero cambiato il sistema sanitario in questo Paese, permettendo l'assunzione di personale medico e infermieristico, programmazione nel sistema sanitario, di cui abbiamo urgente bisogno e l'azzeramento delle liste d'attesa. Cerchiamo di impostare un lavoro con la Commissione d'inchiesta non solo sugli errori fatti,

voteremo a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta e daremo il nostro apporto affinché sia davvero utile a fare chiarezza

ogni volta che la memoria ci riporta, anche per questioni di attualità, al periodo Covid, non posso non non aver chiaro quello che abbiamo passato e quello che ha passato chi aveva delle responsabilità di Governo. Questo vale per i sindaci, come ricordava prima la senatrice

Da uomini abbiamo dovuto prendere decisioni con dei confronti interminabili, con con la consapevolezza che tutto poteva essere giusto e tutto poteva essere sbagliato, perché non avevamo un libretto delle istruzioni che ci spiegasse come si affronta una realtà che non era mai stata affrontata prima nel mondo. Ricordo il giorno delle prime zone rosse; ricordo come ci siamo confrontati per capire qual era la decisione più giusta, qual era lo spazio di intervento che avevamo. Ricordo perfettamente ciò che ci arrivava dal territorio e ricordo perfettamente i dubbi che ciascuno di noi aveva quando

possono fare errori e che stavamo decidendo della vita delle persone. *(Applausi)*. Abbiamo cercato di farlo ascoltando in primo luogo la scienza, il comitato tecnico-scientifico, chi aveva le competenze per aiutarci a prendere quelle decisioni.

in un modo serio, cercando di capire come si può rendere più resiliente il sistema sanitario di questo Paese per affrontare eventuali nuove ondate pandemiche, oppure lo si poteva fare in modo strumentale. Ma anche ove si fosse scelta la prima strada - e così non è - ho dei dubbi e cerco di rispondere a chi, oggi, come il senatore Borghi, dice di poter dire, con il senno di poi, chi ha sbagliato, perché quelle condizioni in cui noi prendevamo le decisioni non sono indifferenti alle decisioni stesse e la valutazione va fatta in quel momento, in quelle condizioni, con quelle conoscenze, non con il senno di poi. *(Applausi).*È troppo facile, con il senno di poi. Avrei voluto vedere voi in quel posto, con Salvini che il 21 febbraio diceva: ascoltiamo la comunità scientifica, blindiamo, sigilliamo i nostri confini, ne va della salute di decine di milioni di persone e sei giorni dopo diceva di riaprire tutto quello che si poteva riaprire, di rilanciare,

«L'opposizione ha tutto il diritto di criticare l'Esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato». *(Applausi)*. Lo dice quella che dava del criminale a Conte.

che introducono una valutazione anche a livello regionale di ciò che non ha funzionato come avrebbe dovuto, noi siamo disposti a votare a favore dell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Basta un emendamento, perché non abbiamo nulla da nascondere, senatrice Sbrollini. *(Applausi)*. E quando mi si viene a dire che uno dei problemi su cui investigare sono i banchi a rotelle, allora chiamate i dirigenti scolastici che hanno voluto i banchi a rotelle, perché non c'è un Ministro che abbia preso quella scelta, esclusivamente una scelta dei dirigenti scolastici. Chiamiamo allora i Presidenti di Regione, non per accusarli, ma perché vogliamo dotarci di qualche strumento in più per affrontare eventuali nuove ondate pandemiche. E che nessuno abbia nulla da nascondere riguarda anche l'altro grande elemento che sta alla base di questa Commissione, almeno per una forza politica come Italia Viva, che ha evidentemente l'ossessione del presidente Conte, perché non fa altro che parlare di lui.

«da quanto si è appreso, la missione russa si sarebbe svolta esclusivamente in ambito sanitario, con il compito di sanificare ospedali e residenze sanitarie assistenziali (RSA) e il convoglio si è mosso sempre scortato dai mezzi militari italiani». È scritto nella relazione dell'attuale ministro Urso, che era a capo del Copasir in quel momento, dopo aver ascoltato il presidente Conte,

La senatrice Pirovano ha detto una cosa giusta: di errori sicuramente ne sono stati fatti, non può non essere così, a tutti i livelli. Tutti possono aver commesso degli errori che, valutati oggi, si manifestano come tali. Quello che però non può, a mio avviso, passare come messaggio è che è che ci siano state delle scelte scientificamente fatte per creare danno al Paese, perché questo è il presupposto di questa maggioranza allargata, anzi non tanto allargata, d'altra parte ho sempre definito il presidente Renzi il peggior Presidente di centrodestra di questo Paese non mi stupisce questo avvicinamento alla maggioranza. Comunque non può passare questo messaggio, perché lo dobbiamo alle persone che non ci sono più, ai loro familiari, ai sanitari che ci hanno rimesso la vita, che si sono adoperati per salvare vite, vite, umiliati da chi prima e poi non vuole capire quali siano le loro esigenze e cerca di mandarli in pensione con il 50 per cento dello stipendio in meno. Il messaggio che passa è questo. C'è stata una gestione politica dell'emergenza. Non c'è stata alcuna gestione politica. C'è stata la gestione di uomini e donne, comprese due persone davvero perbene, come Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che hanno con noi condiviso tutte le scelte che abbiamo fatto in Consiglio dei ministri. Quegli uomini e quelle donne hanno cercato di dare il massimo, nelle loro limitate capacità, per affrontare un disastro che ha colpito l'intero pianeta. Ecco, da questa Commissione emerge, invece, che c'è solo un chiacchiericcio politico. E io credo che non valga la pena soffermarsi oltre. Si manifesta una evidenza. Voi cercate di fare questa Commissione per colpirci, per colpire chi ha gestito il Paese in quella fase, ma vi ritornerà totalmente indietro, come un *boomerang.*

dovrebbe essere la norma che contraddistingue ogni singolo operato della pubblica amministrazione. In sintesi: verificare, in ogni settore, tutti gli impieghi e gli esiti delle risorse messe a disposizione e la coerenza rispetto alle finalità volute, non tanto in una chiave inquisitoria, ma in una visione programmatoria, a garanzia di crescita e sviluppo, del benessere collettivo ed individuale. Semplifico ulteriormente, istituire il *rating* per ogni attività di Governo, perché noi siamo chiamati ad una nuova visione, dove prima dobbiamo valutare, sulla base di dati oggettivi, per orientare le decisioni. Non è più possibile generare debito senza avere prima percorso convintamente la strada della razionalizzazione gestionale e misurate le effettive necessità. Abbiamo sin qui fatto debito per pagare debito - il superbonus ne è controprova - e non per creare PIL in modo strutturale, in un contesto di interessi particolarmente favorevole per chi, come il nostro Paese, era ed è fortemente indebitato. Ma negli ultimi dieci anni il debito pubblico è aumentato di mille miliardi, senza andare a sostenere quei settori di eccellenza che generano prodotto interno lordo strutturale. Scusate se lo ripeto, ma è l'unico fattore in grado di farci uscire dalle secche delle limitate disponibilità di risorse incrementali. Mi auguro che la Commissione, con compiti così vasti, sappia identificare le sacche di inefficienza e le incongruenze, che sicuramente si sono verificate, senza necessariamente andare a prefigurare fattispecie illecite, nella responsabilità dei singoli, che pure ci saranno state. La Commissione, però, dovrà saperci indicare la strada per chiudere quelle maglie larghe che le hanno permesse e, quindi, stupisce che alcuni ne osteggino la costituzione. Il compito, veramente ultimo e meritorio della Commissione, sarà quello di generare una piccola unità che sappia riscrivere procedure per valutare effettivamente tutti gli impieghi, ancor prima degli esiti. E tutto questo in una logica che possa, quindi, consentire di appostare, per ogni singola voce di bilancio, le giuste risorse rispetto ai bisogni. l'ambito di indagine di cui avrà mandato ha la finalità strategica di contribuire, imparando dagli errori del passato, al processo di revisione del nostro Servizio sanitario nazionale in epoca post-Covid, concretamente bilanciato in prevenzione, medicina territoriale e ospedaliera, mediante la finalizzazione mirata e controllata delle risorse disponibili, che consentano in futuro di avere maggiori prestazioni con minore spesa a salvaguardia di tutti i livelli essenziali delle prestazioni a cui devono tendere i nuovi LEA, per evitare, anche nell'eventualità - speriamo remota - di una nuova ondata pandemica, il ripetersi di situazioni emergenziali ad elevata criticità. Riflettere sugli sprechi, anche in emergenza, ci dovrebbe far ragionare sul mancato riconoscimento del giusto ristoro ai medici vittime del Covid, ponendovi finalmente rimedio, non lasciando trascorrere invano un altro 18 marzo, Giornata nazionale della memoria. Ricordare non è sufficiente: bisogna fare. Potrebbe sembrare che non sia il momento di dire chi doveva fare di più e chi di meno, ma sicuramente è il momento di fare emergere le norme che lo hanno permesso. E certamente andare a vedere chi non ha fatto quanto andava fatto negli anni precedenti in termini di prevenzione predittiva e reale contrasto delle malattie infettive è cruciale per non ripetere gli errori del passato, per chiudere le maglie larghe che hanno permesso le criticità e le distorsioni che si devono combattere con un governo dei rischi endemici e pandemici tutta la filiera della sanità umana e animale, implementando efficaci sistemi di sorveglianza, effettivamente predittivi ed integrati, dove l'epidemiologia applicata è fondamentale. Ignorare sarebbe un grave errore storico, etico ed istituzionale, che non renderebbe neppure onore alla memoria di chi non ce l'ha fatta lo dobbiamo anche a loro - andando a percorrere strade diverse da quelle che i problemi li hanno generati. Ed è per questo che abbiamo elaborato il riordino del sistema di emergenza-urgenza e il potenziamento della medicina territoriale di prevenzione assistenza primaria. Questi esempi sono per dire che il mio Gruppo ritiene che il compito più alto della Commissione, in sede di analisi e di approfondimento delle criticità e delle incongruenze che emergeranno, si traduca in un contributo qualificato per la costruzione della sanità del futuro; quella sanità cui siamo chiamati in un orizzonte più ampio, data la complessità e la rilevanza degli interventi necessari in questa legislatura, facendo sì che i risultati degli accertamenti in tempi definiti assurgano a linee guida di indirizzo per la rimodulazione della spesa e per il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale a vocazione universalistica, agendo in prevenzione rinforzata, e governo dei rischi delle zoonosi, atteso che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti rinviene causa diretta o comunque trae origine dal serbatoio animale. E dunque dobbiamo potenziare la sanità veterinaria e la sicurezza alimentare in un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, così come abbiamo previsto nel nostro disegno di legge ordinamentale n. 225, nel quadro di un rafforzamento delle strategie di prevenzione e protezione del benessere delle persone, delle famiglie e della comunità, con un patto di reciprocità fra salute umana, animale ed ambientale che dobbiamo saper promuovere e sviluppare. Non mi resta che confermare convintamente la nostra intenzione di sostenere la Commissione ed augurare buon lavoro.

usare due verbi: ringraziare e ricordare, ricordare e ringraziare. Ricordare, ricostruendo davvero con onestà intellettuale come sono andate le cose, altrimenti si corre il rischio di fare altro male a questo Paese e altro male alla politica, che sarebbe meno importante del primo. è un Paese che ha già sofferto sufficientemente per la pandemia. Ricordare anche perché, senza la correttezza della ricostruzione, non c'è la possibilità di comprendere ciò che è accaduto.

coloro che nei momenti in cui tutti avevano paura di quello che stava accadendo, avevano paura per se stessi e per i propri familiari, non si sono sottratti al proprio dovere e hanno fatto ovunque ciò che dovevano, mostrando anche uno straordinario senso di servizio e responsabilità nei confronti delle proprie comunità. Lo ha ricordato la collega

ringraziare anche tutti coloro che si sono sacrificati nelle corsie degli ospedali facendo straordinari, non risparmiandosi la fatica e regalandoci persino il sorriso. Nel ricordo, credo che oggi in testa a tutti vada chi è stato vittima, chi ha perso la vita per malattia da Covid; ai loro familiari va anche un commosso ricordo di tutti noi che siamo qui, in particolare di coloro che si sono trovati a esercitare responsabilità. Per quanto mi riguarda, ci sono alcune date che sono stampate nella mia memoria. Il 21 febbraio si decise che Codogno doveva chiudere.

primo per modo di dire, perché era chissà che numero, visto che non siamo mai stati in grado di ricostruire dove e chi fosse il paziente zero o il paziente Io ero a Torino, stavo facendo una visita all'ospedale pediatrico, perché avevo in corso una sorta di missione: avevo la delega alla medicina per l'infanzia e avevo deciso di visitare gli ospedali. Ero a Torino, scrissi un messaggio sms al ministro Speranza,

Avevamo tutti tirato un sospiro di sollievo dopo che per un mese non c'era stata più apparentemente alcuna traccia. Nessuna Regione aveva capito, compreso, rintracciato casi che probabilmente invece si andavano uno dopo l'altro preparando ad esplodere tutti insieme. Ebbene, scrissi al ministro Speranza chiedendogli se fosse utile che anch'io fossi presente all'incontro a Milano che il Ministro, insieme al vice ministro Sileri, si accingeva a fare con il presidente Fontana. Andai anch'io a Milano. Di lì in poi è cominciata un'altra vita per tutti, per tutti noi che abbiamo esercitato quelle responsabilità e poi, di mano in mano, per il Paese.

Io pensavo che fosse quasi crudele quest'idea, tant'è che c'era all'epoca un collega - ero stata sua collega come deputata leghista ricorderete sicuramente, l'onorevole Guidesi, che era cittadino di Codogno e rimase chiuso insieme a tutti i suoi concittadini. Ci scrivemmo più volte in quel periodo. La seconda data, il 26 febbraio 2020, è quella della prima informativa del Governo: credo che difficilmente si possa dire che il Governo non fu pronto a riferire immediatamente al Parlamento la gravità della situazione. Poi c'è una terza data che resta incancellabile nella mia memoria: il 27 marzo 2020, Papa Francesco solo in quella piazza che tutti gli italiani videro. Si comprese da quel gesto, dalle sue poche parole - abbiamo però dimenticato - che ci poteva essere solo una cosa più grave della pandemia ed era sprecare quella pandemia, sprecare quel dolore, sprecare quella sofferenza. Oggi è la dimostrazione che quelle parole non sono state comprese. È una dimostrazione molto grave che quelle parole non sono state comprese, perché tutt'altro avremmo dovuto fare in Parlamento che prendere questa strada.

decidemmo di accompagnare a Bergamo medici e infermieri volontari, a cui davvero va una profondissima gratitudine, non solo nostra e di quelli che sono qui, ma di tutti gli italiani che hanno saputo riconoscere quanto generoso sia stato il loro gesto. *(Applausi)*. Mi chiamò il ministro Boccia e mi chiese di accompagnare il gruppo che andava a Bergamo: ci andai insieme al professor Franco Locatelli. Un gruppo andava a Brescia e un altro gruppo andò a Bergamo.

di ricordare come si sentiva, quali erano le impressioni, le sensazioni, i sentimenti, chiusi nelle proprie case, circondati tutti tutti da quel grande e incredibile silenzio che è diventato sacrale in un certo modo, perché accompagnava, giorno dopo giorno, il trasformarsi di un'epidemia che faceva sempre più paura per la sua incapacità di essere conosciuta e impossibilità di trasformarsi in provvedimenti clinici, in terapie e in cure. Non c'erano gli strumenti. un silenzio che però accompagnava una comunità che aspettava col fiato sospeso le decisioni, ma che al tempo stesso noi sentivamo vicina. Vi devo dire che quel 2 aprile a Bergamo, quando andai a visitare l'ospedale che gli alpini regalarono alla città - e li trovai incredibilmente pieni di vita, di voglia di fare e di rispondere - ho avuto la certezza che questo Paese si sarebbe rialzato e avrebbe trovato la forza di ricostruire, passo dopo passo, ciò che la pandemia gli stava portando via. Ebbene, queste date le porto con me, le porterò con me e ancora mi accompagnano. Userò per questo mio intervento un testo, che ho consegnato ed è stato pubblicato, di uno dei tantissimi confronti a distanza che si sono tenuti, quando ancora ero Sottosegretaria alla salute nel Governo Conte II e quando la via di uscita dalla pandemia, individuata poi essenzialmente e principalmente nella vaccinazione di massa, era ancora tutta da percorrere. È per questo che è così grave che oggi in realtà ci si appresti, con l'istituzione di questa Commissione, a riaprire di nuovo i dubbi tra i cittadini italiani sul valore della vaccinazione. Se oggi ci si può ammalare di Covid, e sta avvenendo ancora tanto - sono sicura che ognuno di voi ha un parente o un amico che in questi giorni, in queste ore o nei giorni scorsi è stato ammalato di Covid - se oggi lo possiamo raccontare con più serenità è proprio dovuto al fatto che ci siamo vaccinati. E noi sapevamo che quella era l'unica strada. Invece continuare a insinuare il dubbio che il vaccino sia appunto un siero, che forse produrrà dolore, sofferenze e danno, credo sia di una gravità estrema. Ma anche a questo servirà quella Commissione ed è per questo che mi ha sorpreso molto

destinata e finalizzata a conoscere e a comprendere davvero quali sono i percorsi migliori dal punto di vista organizzativo e amministrativo e soprattutto quale servizio sanitario serve a questo Paese, dove sono state le falle (perché c'erano) e come sono andate le cose, avremmo dovuto fare come hanno fatto gli inglesi e tanti altri Paesi, con una commissione indipendente dalla politica.

Fratelli d'Italia, c'era la Lega e c'erano i colleghi o esponenti di Forza Italia. Così come c'erano, nell'agosto successivo, quelli che dicevano che un giorno bisognava chiudere e un giorno bisognava aprire, un giorno non chiudete abbastanza in fretta e un giorno chiudete troppo, e che andavano a ballare o rivendicavano l'assoluto diritto di aprire le discoteche durante l'estate. Poi - guarda che strano caso - è tornato fortemente il Covid. Dicevo che userò questo testo perché riporta sentimenti e impressioni di ore molto vicine a quei fatti. Dicevo che appunto non si disponeva della vaccinazione. La strada era chiara, ma in quel momento non c'erano le dosi indispensabili per intraprenderla. Di fronte all'idea che ci si potesse impiegare così poco - ricordo quando il ministro Speranza annunciò che si contava di riuscire ad avere il vaccino in un anno,

poco prima che poi, nel 2021, davvero cominciasse invece a funzionare - c'erano anche molti scetticismi, persino nel mondo della scienza, che si interrogava su come questo fosse possibile. Questa è un'altra cosa che ci siamo dimenticati. Come è stato possibile? È stato possibile perché, una volta tanto, abbiamo capito che quella cosa era la più importante. Ma c'era proprio bisogno di avere questa lezione, questo schiaffo in faccia, per capire che bisogna potenziare la ricerca quando parliamo di salute, che bisogna studiare, bisogna impegnarsi e bisogna metterci le risorse che servono? Dobbiamo aspettare che accada per scoprire che non abbiamo numero sufficiente di posti letto e che tra noi e la Germania - dato che oggi parliamo di decessi - c'era una differenza abissale in numero di posti letto e di macchine per la respirazione? C'erano Paesi che avevano già molto di più di noi, mentre noi avevamo coltivato l'idea che la resilienza del Servizio sanitario nazionale, la sua straordinaria capacità di rispondere nonostante i tagli, fosse ancora così importante. Invece non era così: i tagli hanno pesato La strada - come dicevo - era chiara e con l'arrivo dei vaccini in Italia e in Europa e l'avanzare della campagna c'è stata la svolta che avevamo sperato. Tuttavia, fino a quel momento si è dovuto combattere facendo ricorso al distanziamento sociale - parola che abbiamo, anche questa, dimenticato - all'isolamento vero e proprio, ai dispositivi di sicurezza, al potenziamento delle terapie intensive, alla messa a punto di protocolli terapeutici. Ancora oggi, a grande distanza da allora, dall'individuazione del cosiddetto paziente uno, sono in corso studi e ricerche che stanno approfondendo e cominciano davvero a darci risposte, a chiarire dinamiche degli eventi, a interrogarsi sui fatti, sulle risposte del sistema immunitario. Tuttavia, sono ancora molti i dubbi e le domande che la scienza si sta ponendo. Tutto questo non ha interrogato e non interroga solo la scienza, ma chiama in causa la politica, a cominciare da coloro che hanno avuto l'onore - io lo considero tale - e la responsabilità di governare in quanto componenti di Esecutivi nazionali, ma anche di amministratori regionali, a cominciare dai Presidenti delle Regioni, che oggi voi volete lasciare fuori a qualunque costo - guarda che strano caso - ma anche in quanto eletti. In questo io mi rivolgo a chi era in Parlamento: sottosegretario Gemmato, ci incontravamo in Commissione, dove io andavo spessissimo, abbiamo vissuto in Commissione. erano tanti, e oggi ne rivedo ancora molti qui, e si sono trovati a svolgere il loro lavoro parlamentare. Mi domando se vi siete fatti anche voi una domanda. I primi tempi io ricordo una grande unanimità nelle decisioni e nelle scelte. Ma questo vale in riferimento non solo all'attualità e ai suoi protagonisti, ma anche a chi ha governato in passato e ha progressivamente ridotto le risorse e le forze del Servizio sanitario

dove tutto ha avuto inizio, l'Europa e tutti i continenti. La differenza, nella gravità e nella severità dell'impatto, è stata determinata dal tempo, una variabile che ad ogni analisi si rivela centrale, e non solo perché il Covid corre e correva e ha costretto a correre sperabilmente più forte chi doveva contrastarne la diffusione, una macchia d'olio che si espandeva e debordava per ogni dove.

Non per caso si dice che l'Italia ha pagato un prezzo gigantesco, perché è stato il primo Paese occidentale ad essere colpito. Anche per queste ragioni, la prima riflessione che spetta alla politica riguarda il ruolo dell'Europa e delle organizzazioni europee, come lo (OMS). L'Italia si è trovata sola, forse persino pagando, in una fase iniziale e in termini di immagine internazionale, il prezzo di questa sua condizione di solitudine. Anche in faccio appello alla memoria, ai ricordi: all'inizio sembrava quasi una vergogna che questo Paese fosse così fortemente colpito dal Covid, come se fosse una colpa. L'Europa, però, in quel momento non ha saputo fare fronte comune nel momento in cui a Roma il ministro Speranza decideva di bloccare gli arrivi dalla Cina. Guardate che è stato ovunque criticato, aggredito, preso in giro per questa decisione. Eppure, se l'Europa avesse seguito quella decisione, probabilmente avremmo frenato molto di più la pandemia che stava arrivando. Lanciavamo una richiesta di attenzione collettiva rispetto a un pericolo sconosciuto. A Bruxelles in una prima fase si è trascurato questo problema, come se fosse una vicenda destinata a non riguardare l'intera Comunità europea e non è stata colta l'enormità della sfida che avrebbe di lì a poco messo a dura prova tutti i sistemi sanitari di tutti i Paesi. L'OMS, dal canto suo, ha impiegato un tempo eccessivo a dichiarare che il mondo era di fronte a un'emergenza sanitaria globale. Guardate che l'emergenza sanitaria globale entra nelle parole dell'OMS il 30 gennaio 2020, un tempo davvero troppo lungo per mettere nero su bianco che quella da SARS-CoV-2 era pandemia, 11 marzo 2020.

Guai, però, se cercassimo oggi e ci ricordassimo solo questa responsabilità. Sarebbe un errore, l'ennesimo della politica. Ciò non toglie che dobbiamo sapere come sono andate le cose, se davvero siamo intenzionati ad agire perché non accada mai più. E, quindi, certamente occorre fare una grande pressione sull'Europa perché costruisca una risposta a future pandemie a fatti, perché vicende come queste trovino non solo i Paesi singolarmente e individualmente indicati, ma tutta l'Europa pronta a dare una risposta. Dopo gli errori, per fortuna l'Europa ha saputo fare ha saputo fare molto bene, come in occasione delle trattative per la produzione del vaccino e degli altri strumenti come i dispositivi e le terapie che si sono rivelati essenziali e indispensabili. Ma voglio ricordare anche come l'Europa, in qualche modo nella persona di Ursula von der Leyen, volle dare un segno a questo Paese, che era anche un modo per dire a questo Paese che si erano anche loro E lo ha fatto quando è venuta fisicamente a salutare e ha voluto esprimere venendo qui in Italia la sua vicinanza europea a un Paese profondamente sofferente come il nostro era in quei giorni. Così come la dichiarazione di Roma siglata al termine del Global health summit - altra cosa che abbiamo dimenticato - del maggio 2021 ha davvero saputo esprimere. Soprattutto, ha saputo dimostrare il proprio valore e il proprio ruolo per i destini individuali e collettivi quando ha varato il piano di ricostruzione europeo che ci accompagna e che ci dovrebbe accompagnare e che purtroppo questo Governo, soprattutto nella parte della salute, sta secondo me davvero trascurando eccessivamente. Invece da quel PNRR dovevano venire fuori risposte importanti, a cominciare da quella della medicina del territorio su cui questo Governo oggi è ancora al caro amico. sono un piano, un progetto, una parola. Quella era la prima risposta di un Paese che non vuole sprecare, come ci aveva detto il Papa. Più grave ancora di questa sofferenza, c'è solo sprecare tutto questo e noi lo stiamo facendo, voi lo state facendo. Sul Piano nazionale non possiamo che indicare la progressiva riduzione di risorse destinate alla sanità, ma persino nell'affievolirsi del senso del valore del Servizio sanitario pubblico, perché è venuto lentamente meno il senso del valore di uno straordinario patrimonio di questo Paese che è il Servizio sanitario nazionale. E poi c'è lo smantellamento dei distretti, dei dipartimenti di prevenzione, perché eravamo impreparati e il paziente di Codogno sembrava il paziente 0 o 1. Peccato però se andate a prendere la rassegna stampa del dicembre 2019 della Lombardia, troverete un grande numero di articoli in cui si denuncia la presenza di una strana diffusione di polmoniti,

prigionieri nei condomini in cui vivevano e li guardavamo come fosse una cosa così lontana e distante da noi che non avrebbe mai potuto toccarci (succede in Cina, pensavamo; come se si sapesse non abbia alcuna possibilità di competere con noi). Eppure noi intanto avevamo strane pandemie di polmonite a cui nessuno ha poi

tecnico scientifico, il CTS. Mi riferisco a uno pneumologo di chiara fama, il professor Richeldi. Nella sua straordinaria onestà, il professor Richeldi ha pubblicato un libro che vi vi invito a leggere, perché già in esso, secondo me, trovereste tutte le risposte che dite di voler cercare con questa Commissione d'inchiesta sul Covid. Egli racconta

A quel punto, decise di scrivere a un amico e collega che aveva conosciuto e con cui aveva lavorato a Londra (poi è rientrato in Italia, per fortuna, il professor Richeldi).

(venne chiamato con la richiesta di andarlo a sdoganare, poiché arrivava dalla Cina). Quel pacchetto conteneva decine e decine di mascherine: era un segnale evidente che il professore dalla Cina voleva mandare al suo collega, a cui aveva dovuto mandare una comunicazione ufficiale - non essendogli possibile fare altro, evidentemente

in una stanza della sede operativa della Protezione civile in via Vitorchiano (dove abbiamo vissuto il ministro Boccia, io e tanti altri, anche molto più meritevoli di noi di essere ricordati qui oggi)

epidemia ignota, senza precedenti oltre alla Cina, nessun protocollo per affrontare il virus, nessuna cura. Un vero *shock* per uno scienziato, che però oggi spiega tanto di ciò che da quel momento in poi abbiamo fatto e della tanta straordinaria strada che abbiamo percorso. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che questo Paese ha saputo fare, perché ha dato un esempio che è stato poi ripreso dagli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito, che hanno adottato, esattamente come noi, l'isolamento

Fate molto male, oggi, a pensare che si possa processare fintamente la storia e fa molto male chi, come ho sentito ieri in quest'Aula, ricorda le buone Commissioni di inchiesta. Peccato che abbia dimenticato, ad esempio, la Commissione Telekom Serbia. Una Commissione che sceglie con una maggioranza politica qual è il risultato di quell'indagine, è una Commissione che tradisce la fiducia degli elettori e tradisce anche i suoi compiti. Noi non abbiamo paura, però vi conosciamo; ed è per questa ragione che pensiamo che questa Commissione non doveva in alcun modo avere corso. In ogni caso, non temiamo e portiamo davvero a testa alta la responsabilità di ciò che è stato fatto. Lo facciamo con disciplina ed onore. Lo faremo fino in fondo. finestra"). Alla luce della convocazione della Giunta per il Regolamento, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14,45.

difficile parlare di quel periodo storico in Italia, anche perché sembra passata un'eternità; sembrano passati davvero tanti anni, più di quelli realmente trascorsi, da quando il Covid ha travolto l'Italia e gli italiani, e da quando da quando oltre 190.000 nostri concittadini sono morti, molti dei quali non sono stati neanche abbracciati dai propri cari poiché morti da soli nelle corsie degli ospedali o nelle case di cura per anziani. Sembra passato tantissimo tempo, ma in realtà ciò che è successo in quel periodo credo che sia rimasto nella memoria di tutti. È stato un periodo nel quale le famiglie italiane hanno vissuto dei drammi, hanno visto i parenti morire, sono visti chiusi in casa. L'Italia ha visto qualcosa che non avrebbe mai pensato di vedere. L'ha già detto qualcuno prima di me:

italiani. Qualcuno ha detto che questa Commissione d'inchiesta è un atto di vigliaccheria; qualcuno ci ha dato dei vigliacchi.

che questa maggioranza sia scappata dalla Camera quando è stata votata la Commissione Covid; non mi sembra che fosse questa maggioranza o Fratelli d'Italia a scappare dopo le conferenze stampa a reti unificate per non dare risposte agli italiani. Non mi sembra che sia questa maggioranza a scappare per non dare le risposte che verranno date dalla Commissione d'inchiesta. Mi sembra che sia qualcun altro che stia scappando e che sia vigliacco. Lo dico perché molti hanno detto: noi ci siamo assunti le responsabilità di quello che abbiamo fatto. A me hanno anche insegnato che chi si assume le responsabilità lo fa fino in fondo: se le assume prima, se le assume dopo e se le assume durante quello che accade. Oggi noi vi chiediamo: vi volete assumere quelle responsabilità? Avete il coraggio di spiegare perché avete fatto determinate scelte? Avete il coraggio di dare le risposte che in quel periodo non avete dato? *(Applausi)*. Questo è quello che vi chiediamo e quello che bisogna dire in quella Commissione. Questo vuol dire assumersi le responsabilità.

Allora, assumetevi le responsabilità di quello che è successo e delle scelte che avete fatto in quel periodo. Assumetevi le responsabilità di quelle scelte

*(FdI)*. Assumetevi la responsabilità di spiegarci perché non avete ritenuto di adottare il piano pandemico, perché non avete ritenuto di utilizzare quello esistente e non l'avete aggiornato. Spiegateci la responsabilità e spiegateci a che cosa dovevano servire i centri "primule", l'app Immuni, i soldi spesi per roba che non è mai arrivata. Spiegateci perché partivano milioni di mascherine verso la Cina quando servivano in Italia. *(Applausi)*. Spiegateci perché avete nascosto le carte e non rispondevate alle interrogazioni né alla Camera, né al Senato, e non rispondevate neanche agli accessi agli atti. Fratelli d'Italia ha dovuto fare dei ricorsi al Consiglio di Stato - che ha vinto - per avere gli atti. *(Applausi)*. Spiegate perché avete voluto nascondere tutto in quel periodo e lo volete nascondere oggi. Spiegate - e spiegherete - il rapporto ritirato che doveva essere pubblicato dall'OMS, che diceva che l'Italia non era pronta, perché qualcuno si è adoperato perché non venisse pubblicato. Spiegate agli italiani perché

Degli effetti avversi non si può parlare, perché sennò si demolisce il vaccino. Eppure, anche nel bugiardino dell'aspirina sono descritti gli effetti avversi, ma il vaccino non ha effetti avversi. Spiegate e spiegherete il *green pass*, spiegherete perché ci avete chiuso in casa quando non ce n'era bisogno e quando invece c'era bisogno di chiudere non avete chiuso. Avete detto: ci avete chiesto di chiudere e di aprire, non siete stati coerenti. Qualcuno ha ricordato delle date; forse la collega Zampa si è scordata nell'elenco delle date che mentre

Per favore lasciamo intervenire il collega, come i colleghi hanno lasciato intervenire voi. LISEI *(FdI)*. Però siamo felici se

avete imparato che bisogna difendere i medici e noi ne siamo strafelici, perché i medici sono diventati eroi, ma durante quel periodo i medici erano da soli nelle corsie, senza le mascherine, senza i dispositivi di protezione e senza gli strumenti. *(Applausi)*. All'inizio della pandemia a coloro che avevano le mascherine era impedito di utilizzarle. Sono state date delle direttive negli ospedali: non mettete le mascherine, perché spaventate la gente. *(Applausi)*. Questo veniva detto negli ospedali e questo veniva detto in tanti luoghi d'Italia: non mettete le mascherine, perché spaventate le persone. *(Commenti)*. Per favore, lasciamo intervenire il collega, come i colleghi hanno lasciato intervenire voi. E due. da questo tragico periodo abbiate imparato qualcosa. Sono contento di aver sentito la senatrice Zampa ricredersi sui tagli alla sanità e parlare di tagli alla sanità, seduta a fianco di Beatrice Lorenzin, che ha fatto quei tagli alla sanità prima di lei.

Era molto semplice evitare questa Commissione d'inchiesta, perché tutti fanno degli errori; io per primo faccio tantissimi errori. Il problema è prendere contezza dei propri errori, ammettere di aver fatto quegli errori, spiegare perché qualcuno ha fatto quegli errori. Ma voi ci avete raccontato fino ad oggi che siete stati bravissimi, che qualsiasi errore è sanato perché era una situazione di emergenza, che qualsiasi cavolata sia stata fatta era inevitabile. Però i dati dell'Italia, rispetto agli altri Paesi, ci dicono che l'Italia, nonostante sia stato il Paese con le maggiori restrizioni al mondo, è anche il Paese che ha i dati peggiori per quanto Quando l'Italia chiudeva e altri Paesi aprivano, come la Svezia, qua venivano criticati e venivano guardati come dei marziani. Venivano Venivano inseguite le persone con i droni sulle spiagge; ci sono state delle scene surreali durante la pandemia. Io credo che, se non si ha niente da nascondere e se non si è vigliacchi, si affronta la Commissione d'inchiesta con la massima serenità, con la serenità di chi anche in quel periodo o in parte di quel periodo governava *(Commenti)*. Invece c'è qualcuno che evidentemente ha paura della Commissione di inchiesta, c'è qualcuno che pensa c'è qualcuno che pensa e ha paura che la Commissione d'inchiesta sia un plotone di esecuzione. Si è parlato di plotone di esecuzione. Qualcuno ha paura che questa Commissione d'inchiesta sia un plotone di esecuzione. Qualcuno ha paura che useremo questa Commissione d'inchiesta per sostituirci alla magistratura. Qualcuno ha paura che questa Commissione d'inchiesta venga utilizzata come uno strumento per condannare l'operato di chi c'era allora. Guardate, vi dico una cosa: forse non ve ne siete accorti, ma l'amico Conte e l'amico Speranza sono già stati condannati dagli italiani. Quella maggioranza è già stata condannata dagli italiani il 25 settembre. È già stata punita per le scelte che ha fatto; noi non dobbiamo condannare nessuno e non dobbiamo sostituirci alla magistratura, anche perché, se il timore fosse quello, non bisognerebbe fare neanche una Commissione d'inchiesta, visto che le Commissioni d'inchiesta hanno un'altra funzionalità, come ha detto molto meglio di me il collega Renzi. Per carità, abbiamo fatto Commissioni d'inchiesta su qualsiasi cosa; magari qualcuno può ritenere che fare una Commissione d'inchiesta su un evento come questo sia inutile. Noi riteniamo di no riteniamo che la Commissione abbia uno e un solo scopo, quello di perseguire la verità. Ha uno e un solo scopo, quello di spiegare a milioni di italiani perché sono successe determinate cose. Ha uno e un solo scopo, quello di scoprire, anche all'interno dei procedimenti giudiziari che ci sono, chi ha detto cosa e cosa è accaduto veramente. Credo che, quando si persegue e si insegue la verità e la trasparenza, saranno poi gli italiani a giudicare se la Commissione d'inchiesta Covid era utile o meno. Noi non abbiamo paura; qualcun altro evidentemente ne ha molta.

Signor Presidente, è difficile replicare dopo un dibattito che ha anticipato molti dei temi,

senatori intervenuti e la loro consapevolezza di aver fatto tutto il possibile sulla base delle conoscenze e, come ha detto qualcuno, sulla base condizioni nel momento in cui bisognava prendere le decisioni, non avrei nessuna paura, perché sarei certo che da questa Commissione uscirà la verità e sarei certo che la verità sarà quella che non poteva essere fatto

all'esito dei suoi lavori, quando sarà costituita, avremo finalmente una verità basata sui fatti e quella Commissione metterà a tacere tutte le polemiche che in questi anni, esattamente dal marzo 2020, si sono succedute e moltiplicate nel Paese.

quindi in cosa può far paura una Commissione che deve dare queste risposte, perché non si vuole questa Commissione che deve dare queste risposte nel pieno delle conoscenze scientifiche che potrà avere leggendo tutti gli atti? Non solo i colleghi che oggi siedono all'opposizione e che hanno avuto ruoli di Governo hanno dovuto gestire la pandemia. Io ero assessore presso la Regione Liguria e, sebbene all'epoca fossi all'opposizione in Parlamento, ero in maggioranza in Regione, dove abbiamo dovuto fare moltissime scelte, alcune anche antecedenti a quelle del Governo: il 24 febbraio 2020 la Liguria ha emanato un'ordinanza molto restrittiva rispetto a ciò che i cittadini liguri potevano fare. Anche lo abbiamo fatto con le conoscenze che avevamo in quel momento e io non avrei nessuna paura se in Regione Liguria fosse

Ci sarà poi anche una parte di ricerca per valutare se ci sono stati degli sprechi, se ci sono stati comportamenti al limite del lecito o dell'illecito, come si fa in tutte le Commissioni. Mi dispiace che un'altra ossessione che colpisce soprattutto un Gruppo politico sia quella dei banchi a rotelle, perché non c'è bisogno di far rientrare le Regioni nelle

Quindi, basta chiedere al Ministero dell'istruzione cosa è successo nel 2021, senza dimenticare che la Ministra dell'istruzione, nel libro che ha scritto, ha ribadito e ha

ci sono aspetti che sono incomprensibili e che è bene capire anche in prospettiva futura, come quando si è deciso che sui *pullman* di trasporto pubblico non si potesse salire prima oltre il 30 e poi il 50 per cento della loro capienza, unico caso in Europa che ha esposto l'Italia a un un caos nei trasporti e a spese incredibili per portare, ad esempio, i ragazzi a scuola, con i treni che viaggiavano mezzi vuoti per comando quando non ce n'era alcuna necessità, quando nessun altro Paese ha adottato questa misura. quando si stabilì che sulle macchine si potesse stare in due, uno seduto davanti, uno seduto dietro, come se nell'abitacolo di una macchina il virus non circolasse da davanti a dietro. tutte cose che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Era giusto, era sbagliato? A mio parere era sbagliato, ma ci sarà nella Commissione il modo, anche scientifico, di capire perché certe scelte sono state prese e per capire se o cinquant'anni, se ci sarà ancora questa condizione e con queste stesse macchine, dovremo viaggiare sui *pullman* e sulle macchine nella medesima situazione.

portare un contributo che auspico sia di serenità al dibattito di questa sera, nella misura nella misura in cui vorrei condividere un sentimento che è quello che sottende all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, che non è punitivo, ma collaborativo e di emersione della verità. Faccio un esempio. Come la collega Cinzia Pellegrino, anche il relatore senatore Berrino richiamava il tema dei banchi a rotelle. In maniera appassionata, una collega del MoVimento 5 Stelle rappresentava le giustissime, a

l'istituzione di una Commissione d'inchiesta è un atto puramente parlamentare, quindi non è stato il Governo a volere l'istituzione della Commissione, ma si tratta di un organo parlamentare che nasce in Parlamento, che non vede rappresentanti del Governo al suo interno e quindi e quindi ha una genesi parlamentare e per questo, rappresentando il Parlamento il popolo italiano, ha un'enorme valenza. I temi da sottolineare sono tanti. Nel dibattito, su uno in

nella banale propaganda politica. Mi sto convincendo che, a furia di ripeterlo, vi stiate convincendo veramente del fatto che il Governo Meloni abbia tagliato il Fondo sanitario nazionale. *(Applausi)*. E questo mi porta a citarvi qualche dato e numero, e lo farò in maniera incidentale: me ne scuso con la Presidenza e con l'Assemblea, ma l'argomento è stato introdotto durante la discussione e non posso non lasciare traccia di una verità rappresentata dal Governo. Nel 2019 il Fondo sanitario nazionale si dotava di 115 miliardi di euro.

2024, 136 miliardi di euro; sono 21 miliardi di euro in poco più di quattro anni alla sanità pubblica. Se ci fossero sempre tagli così, direi evviva i tagli alla sanità pubblica, se un Governo li facesse sempre tanto puntuali. Ora, se nel 2019 con 115 miliardi di euro non si gridava allo scandalo e non si parlava di una sanità complessa e in difficoltà - cosa che in realtà è, evidentemente, così come ha detto il presidente Meloni - insieme a una maggiore dotazione del Fondo sanitario nazionale che abbiamo dato alla Nazione con questa legge di bilancio, servono nuovi modelli organizzativi ai quali siamo chiamati tutti quanti insieme a concorrere. Peraltro, pur non volendo scendere troppo nel tecnico, lo faccio perché sono nel Senato della Repubblica: se confrontiamo i dati, anche quelli prodotti dal vostro Governo nel 2023 (specificatamente ad aprile, nel DEF), prevedevate

e il 6,1 di percentuale rispetto al PIL del Fondo sanitario nazionale; noi in fase previsionale abbiamo appostato il 6,2 (e il 6,2

quindi, ai 2,3 miliardi di euro in più che avevamo messo nel DEF abbiamo aggiunto 3,3 miliardi, dunque 5,6 miliardi di euro in più solo per quest'anno. *(Applausi)*. Vi prego: non dite più che stiamo tagliando il Fondo sanitario nazionale oppure continuate a dirlo, ma evidentemente i risultati elettorali non vi arriveranno, perché il popolo italiano non è un popolo di stupidi *(Applausi)* e in generale, ma soprattutto quando si parla di numeri, sa discernere fra chi dice fesserie e chi dice verità.

È del tutto evidente - e l'intervento del Sottosegretario lo dimostra - che vi manca la cultura del Governo. *(Applausi)*. Vi mancano la cultura di Governo e il rispetto istituzionale.

Quindi, avendo io avuto un ruolo all'interno del Governo Conte II, quando, in piena pandemia, ero Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, penso di avere non il diritto, ma il dovere di spiegare alcune questioni. Le spiego perché. Credendo io profondamente nei valori delle Commissioni d'inchiesta, così come sono e come dovrebbero essere le Commissioni di inchiesta,

che si è trovato a gestire la pandemia, mi sono sentita e mi sto sentendo sotto processo. In una Roma deserta per il *lockdown*, risuonavano sui sanpietrini i passi dei pochi che potevano uscire e che uscivano, come per esempio chi aveva dei ruoli di Governo, per provare a trovare delle soluzioni dopo le lunghe riunioni.

eravamo il primo Paese europeo ad affrontare la pandemia; eravamo anche il primo Paese in Occidente ad affrontarla.

perché non c'erano un ricettario, una regola o un manuale per la sopravvivenza. C'era da capire che cosa fare andando per tentativi, tentativi che poi sono stati utilizzati dai Paesi entrati in pandemia dopo di noi e che hanno guardato quello che l'Italia ha fatto per provare a farlo. Tra quelle cose lo dico cercando di riportare un po' di onestà intellettuale nel dibattito - siamo stati costretti nostro malgrado a chiudere le scuole. ricordo a tutti che le parole con cui abbiamo chiuso le scuole sono state «quei danni li rivedremo dopo», perché noi dovevamo salvare

Colleghi, per favore, lasciamo parlare la collega.

di risorse che servivano per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; per potenziare la didattica digitale e, poi, ancora per riaprire le scuole, per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti, per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo è quello che è stato stanziato e per le finalità Concludo perché vorrei evitare di sentirmi sotto processo per aver provato a lavorare a mani nude per salvare vite umane, per garantire ai nostri ragazzi di rientrare a scuola in presenza, sperimentando ciò che non era ancora stato sperimentato. Per il resto, complimenti, perché invece per voi la politica sta da tutta un'altra parte. Noi proveremo ad aspettarvi là quando ci arriveremo.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento, sulla base delle comunicazioni del Sottosegretario e quindi del Governo, chiedo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare immediatamente una discussione su quanto comunicato dal Sottosegretario.

tra il mantenimento della correttezza negli scontri politici anche duri tra maggioranza e opposizione e la scorrettezza nel far valere invece solo la logica dei numeri con arroganza e con prepotenza? *(Applausi)*. Potrei dirvi che ho vissuto passo dopo passo il trauma della gestione della pandemia, piombata all'improvviso nella vita del Governo e nella vita degli italiani. Potrei dirvi che sono passati mesi in cui abbiamo operato senza alcun punto di riferimento: non arrivavano notizie da nessuna parte del mondo perché eravamo il primo Paese occidentale a gestire la pandemia. Potrei dirvi del trauma di una gestione ignota, inaspettata nella vita di un Governo e degli italiani. Potrei dirvi che abbiamo operato sempre secondo il criterio di maggior prudenza e, quando molto spesso si è trattato di dover decidere tra salute e economia, abbiamo scelto prioritariamente di tutelare la salute. Potrei ricordarvi il dramma dell'assenza di mascherine, delle terapie intensive che non bastavano, dei pronto soccorso invasi dalle persone, del numero dei contagi che si prevedeva crescente sempre di più e che andava affrontato. Avevamo il dovere di tentarle tutte, anche a costo di sbagliare perché, quando si governa, si sbaglia anche. Potrei dirvi in coscienza che abbiamo fatto tutto il possibile e che personalmente trovo ingiusto trovarmi in stato di accusa, pur non temendo per niente l'esito di questa Commissione d'inchiesta che lavorerà soltanto secondo criteri di maggioranza. Lo trovo comunque profondamente ingiusto e guardo con un certo

Governo precedente. Non è mai successo e nella vostra superficialità non vi rendete conto che state creando un precedente, in base al quale ogni Governo successivo potrebbe creare una Commissione d'inchiesta sulle scelte politiche del Governo precedente: un *boomerang* per voi. Non vi fermerete, lo sappiamo. Non ci saranno casi di coscienza, ma mi basterebbe questo: quando voterete pensate che state sbagliando, che state commettendo un errore, perché le regole della democrazia e dell'alternanza devono restare e devono essere fatte di rispetto reciproco e non di abuso della forza dei numeri e del potere.

le ha spiegate adesso il senatore Franceschini, seppur facendo un intervento non nel merito dell'emendamento, ma più generale rispetto al dibattito politico che si è sviluppato anche nella giornata di oggi e alle cose che abbiamo sentito dire dal Sottosegretario. Altre cose abbiamo avuto modo di dirle ieri durante l'illustrazione delle questioni pregiudiziali. Ripeto una cosa che ho detto anche ieri e che penso debba entrare in questo dibattito parlamentare. Peraltro se ne era discusso anche alla Camera la scorsa estate, quando

eravamo in una condizione tale - chi fa finta oggi di non ricordarselo, penso agisca con significativi elementi di malafede - per cui qualunque decisione si prendeva, quella decisione inevitabilmente emergevano contrasti, perché questo accade in una situazione inedita. Fu talmente inedita (lo ricordo ai colleghi, perché forse se lo dimenticano) che quell'anno furono spostate le Olimpiadi. Non semplicemente una scuola chiusa, ma le Olimpiadi. *(Applausi)*. Erano duemila anni che non erano mai state toccate, nemmeno durante le guerre. Furono spostate le Olimpiadi, per capire di cosa sto parlando: una cosa un po' più grande della polemica politica

Tenere aperte le scuole significava inevitabilmente rischiare di far precipitare la condizione sanitaria, chiuderle significava, altrettanto difficilmente, mettere in discussione la didattica così come l'avevamo conosciuta fino a quel momento, sperimentare una cosa complessa come la didattica a distanza. Insomma, era la classica situazione in cui qualunque decisione prendi naturalmente te ne assumi le responsabilità fino in fondo e rischi di sbagliare. Ora, francamente,

tre anni dopo, voi che in quei mesi avete raccontato tutto e il contrario di tutto e che per l'appunto non avete avuto la decenza, in una fase così complessa della storia di questo Paese, di farvi fino in fondo carico della complessità della situazione? È la classica situazione in cui Governo e opposizione non dovrebbero esistere, ma dovrebbe esistere semplicemente la salvaguardia dell'interesse di tutti, per gestire la pandemia più complessa con la quale questo Paese e il mondo intero si sono confrontati nel corso degli ultimi decenni. Davvero potete farci questa morale di quart'ordine? Davvero chi ha detto, nel corso di quei giorni, che bisognava prima aprire tutto e poi chiudere tutto oggi può cercare di mettere in campo un processo politico, dal quale però, guarda caso,

pandemia. Io penso che davvero la propaganda, la strumentalizzazione e il cinismo dovrebbero una volta tanto, quando si parla di cose serie come una pandemia, lasciare il passo, cedere il passo. *(Applausi)*. È per questo che abbiamo presentato questo emendamento soppressivo, perché pensiamo che l'istituzione di questa Commissione non sia certo un modo per fare chiarezza sul Covid; non lo vuole essere anche e soprattutto per decisione vostra, visto che avete escluso che questa Commissione potesse occuparsi anche dei livelli di governo territoriale. Essa risponde a una pura scelta politica,

il mio contributo è stato sempre lo stesso, finalizzato a promuovere l'inclusione fra gli elementi di interesse di questa Commissione anche delle Regioni e delle Province autonome. Ritengo che effettivamente adesso, al di là di qualsiasi discussione politica o partitica, aver soppresso dall'inizio la possibilità per tutti noi di conoscere la verità su ciò che è accaduto nelle Regioni, nelle Province autonome, negli enti locali e quindi poi, a catena, anche nelle aziende sanitarie, nelle ASL e nelle RSA significhi effettivamente non avvicinarci neanche un po' alla verità. È chiaro che

si parla di estendere l'analisi della Commissione parlamentare d'inchiesta alle Regioni e alle Province autonome. Se mi sarà concesso, Presidente, in fase di dichiarazione di voto su ogni emendamento, mi alzerò per ricordare a questo Senato della Repubblica che ha voluto oscurare la verità.

anche in un'Aula che solitamente si ascolta poco, di ascoltarci a vicenda. Quando nei mesi scorsi ci furono polemiche che investivano il ruolo del Presidente della Regione Lombardia e del Presidente della Regione Veneto, oltre che del presidente del Consiglio Conte e del ministro Speranza (per altri versi), io intervenni in più di un'occasione per difendere gli uni e gli altri, per dire che ogni strumentalizzazione politica rispetto ad una verità ricostruita *a posteriori* secondo logiche di comodo sul funzionamento delle Regioni Lombardia e Veneto e sul funzionamento del Governo nazionale non poteva che essere una polemica basata solo su intenti politici. questo perché credo che ci sia in quest'Aula chi in qualche modo si sforza di vedere le cose secondo una logica di obiettività. Io sono contrario a questa Commissione d'inchiesta, ma aggiungo, a beneficio dei colleghi della mia parte politica che domani si appresteranno a votare una Commissione d'inchiesta istituita per fatti diversi, che io esprimo una contrarietà di fondo all'uso improprio che questo Parlamento da tempo sta facendo sulla costituzione

Io penso che qualsiasi persona in buona fede in quest'Aula, a partire dai tempi di lavoro che basta confrontare con quelli di vent'anni fa o di trent'anni fa, capisce che è in atto una sorta di espropriazione della competenza del Parlamento. Il Parlamento tutto - anche quello della scorsa legislatura, non mi riferisco solo a quello attuale - registra una drammatica perdita di peso politico e istituzionale a beneficio di altri soggetti *(Applausi)*, che naturalmente sono il soggetto del Governo, ma non solo, perché sappiamo che ci sono stati nella storia recente d'Italia anche appropriazioni indebite rispetto al potere autonomo di legiferare del Parlamento da parte di soggetti che le leggi dovrebbero applicarle e non sindacarle. Dunque, abbiamo un problema serissimo di perdita di identità e di peso del Parlamento. Come reagisce il legislatore a questa perdita di peso legislativo? Cercando di avventurarsi sul terreno di nuove competenze e nella storia d'Italia questa pratica è stata riservata a fatti del tutto particolari - pensiamo alla Commissione d'inchiesta Anselmi sulla P2 - eventi che hanno costituito assolute eccezioni rispetto alla normalità.

in questo Paese come negli altri - perché questa è la democrazia - i Governi passano (il Parlamento dovrebbe rimanere). Quale principio si istituisce se davanti a emergenze drammatiche come il Covid la maggioranza che segue si prende il diritto di sindacare con una Commissione di inchiesta, che è diversa rispetto a una Commissione di indagine parlamentare che dà un giudizio politico, in quanto la prima

a un arrivo anomalo di immigrati - perché mai ne sono arrivati come oggi e certamente nessuno di noi in buona fede attribuisce la colpa individualmente alla presidente Meloni, perché non sarebbe leale, sappiamo che ci sono

Qui il tema non è la paura della verità, perché la paura della verità è un altro film, è un'altra cosa. Tra l'altro, chi dice che c'è paura della verità,

di essere espropriato giornalmente si va a prendere competenze che non gli spettano quando ci sono indagini giudiziarie in corso e il principio dell'autonomia della magistratura e anche della sua indipendenza, ma anche le sue prerogative di avere la responsabilità di un giudizio di questo tipo sono assolutamente insindacabili. Oggi istituiamo la Commissione d'inchiesta sulla vicenda del Covid, che è stato sostanzialmente un cataclisma mondiale. Guardate quali altri Paesi stanno procedendo come stiamo procedendo noi: quasi nessuno. Dico quasi perché nella statistica poi magari spunta fuori un piccolo Paese che ha istituito una Commissione d'inchiesta, ma non mi risulta che ce ne sia un altro. Domani istituiremo una Commissione di inchiesta su un fatto drammatico che ha riguardato una famiglia e la sparizione di una ragazza quarant'anni fa. Ma voi pensate realisticamente che il Parlamento possa apportare delle novità sconvolgenti rispetto ad indagini giudiziarie che durano da anni e che sono state peraltro oggi rilanciate dall'autorità giudiziaria? Noi suppliamo a tutto questo con un errore oggi che si moltiplicherà domani in un altro errore. Voglio dire con chiarezza che voterò contro l'istituzione di queste Commissioni di inchiesta o non parteciperò al voto, perché ritengo che stiamo mettendo un'altra pietra nella delegittimazione dell'istituto parlamentare. Il Parlamento con queste Commissioni d'inchiesta non sarà più forte, ma registrerà solo le sue debolezze, perché sarà permeabile alle strumentalizzazioni politiche. Mi dispiace molto.

allora saremmo di fronte a un elemento positivo che serve alla società. La circostanza non soltanto delle ragioni dette, ma che ci sia un riferimento all'articolo 1, che fa riferimento anche al fine di far fronte a emergenze future, fa capire la natura dell'intervento,

con il senno di poi, per quello che possiamo fare in futuro, da quella che si aveva nel momento in cui si è presa una decisione. Oggi abbiamo un grande vantaggio nel valutare cos'è successo in quei momenti terribili: il fatto di essere sopravvissuti. Non abbiamo un controfattuale

un decreto-legge in Parlamento che viene subito emendato. Gli unici paragoni che abbiamo a livello internazionale sono gli Stati Uniti di Trump il Brasile di Bolsonaro, quei luoghi in cui per moltissimo tempo si è negata l'esistenza del virus. Adesso non voglio fare richiami

procede tutto molto bene; grazie alle strette misure che abbiamo preso, possiamo dire che l'Italia è sicura, anche perché abbiamo isolato il virus per la prima volta nel mondo. Si trasmetteva scambiando evidentemente il fatto che si possa isolare un virus in laboratorio - cosa che può fare qualunque Paese ai fini di studiarne la mutazione e l'evoluzione - col fatto che invece il virus fosse stato isolato e, quindi, non ci fosse più il contagio. A parte questo, è evidente che la conoscenza è un tema fondamentale. A me la cosa che dispiace di più rispetto a questo tipo di attività è che invece non c'è esattamente il rispetto della conoscenza e del rapporto fra politica e scienza, che è fatto di di consapevolezza dell'ignoranza e dei nostri limiti, ma anche del rispetto nei confronti delle persone che lavorano nel mondo sanitario e scientifico e che quindi, attraverso quelle misure, ci raccontano la verità che viene raggiunta in quel momento e che disegna anche le attività politiche. Rispetto al nuovo

dei rischi dei vaccini: a parte che questo è facilmente verificabile che non è vero, ma allora ciò che significa? Significa che stiamo tornando di nuovo ad aprire un tema no vax? Ora, se questo io posso capirlo in un contesto elettorale, quando si è in una posizione di Governo, incoraggiare la disinformazione per una ricerca di consenso, incoraggiare forme del tutto incontrollate di opinionismo su questioni scientifiche, significa veramente far fare un passo indietro indietro al Paese. Noi siamo usciti dalla pandemia e ricordo che siamo stati i primi a entrarci. Quello che sostanzialmente possiamo ricordare di quei giorni erano le ragazze che giocavano a tennis su due tetti, le persone, chiuse in isolamento, che cantavano in una periferia di Napoli, e tutta una serie di meccanismi di solidarietà che ci facevano dire: ne usciremo migliori. Ecco, noi, come parte politica, possiamo dire che ne siamo usciti. Sulla qualificazione di chi ne è uscito meglio o peggio, speriamo che il Paese non debba essere interrogato molto presto.

e non riusciamo a comprendere come mai l'opposizione continui a pensare che si voglia istituire questa Commissione per processare membri del Governo passato. Abbiamo ribadito più volte che l'intento di questa Commissione è cercare di capire gli errori che tutti hanno fatto, che tutti abbiamo fatto; l'intento è cercare di usare questa Commissione per

Il Parlamento, senatore Casini, non può trasformarsi in un contropotere giudiziario rispetto alla magistratura, né tantomeno può decidere se una legge sia conforme o meno alla Costituzione. Esistono degli organismi indipendenti che devono fare questo. Lo dico perché poi qui

Signor Presidente, mi fa piacere, intanto, vedere che i toni di questa discussione si sono un po' placati, perché davvero è questione di rispetto per le tante persone che hanno perso familiari, cari o che semplicemente hanno sofferto molto. Penso, però, che tutti noi abbiamo sofferto molto in quel periodo. Visto che il presidente Romeo ha invitato tutti, appunto, a stare calmi, perché c'è buona fede nell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, allora rivolgo un invito al senatore Romeo, alla Lega e a tutte le forze di maggioranza. Gli emendamenti sono molto pochi. Votino gli emendamenti in cui si istituisce una Commissione d'inchiesta che davvero va ad agire su tutti i livelli decisionali, cioè sul livello nazionale, sul livello regionale, sul livello locale. Ve ne sono tanti di emendamenti di questo tipo. L'unico modo che avete per dimostrare la vostra buona fede è fede è votare a favore di questi emendamenti, perché, altrimenti, le chiacchiere stanno assolutamente a zero.

rispetto alla necessità riconosciuta di individuare nella Commissione di inchiesta lo strumento attraverso il quale riuscire a fare chiarezza rispetto a quanto accaduto nei tragici mesi del Covid. Prima di essere eletto al Senato, ero un consigliere regionale del Veneto e nel giugno 2021 il Partito Democratico, in mille occasioni, chiese con grandissima virulenza che venisse - scusate il termine che magari è poco appropriato, visto che si parlava di Covid - che venisse istituita una commissione d'inchiesta in Veneto per accertare le gravissime responsabilità *(Applausi)* che evidentemente venivano accreditate a chi amministrava la a cominciare dal presidente Zaia, dalla sua Giunta e dalla sua maggioranza. Noi, che eravamo in maggioranza, decidemmo di acconsentire. C'è qui un un testimone che ha partecipato, il nostro collega Crisanti, componente del Partito Democratico, che all'epoca non faceva politica nel Partito Democratico, ma si occupava di virologia negli ospedali e magari talvolta anche in televisione. Il collega Crisanti è stato, almeno una volta, ospite della commissione d'inchiesta proprio per permettere ai colleghi, allora consiglieri regionali, di avere tutti gli elementi utili per comprendere se

una autorevole rappresentante del Partito Democratico. *(Applausi)*. Il Partito Democratico dice che la commissione di inchiesta

molteplici audizioni e alla fine prodotti dei documenti che potranno essere validamente acquisiti dalla Commissione di inchiesta che andiamo a a costituire e che permetteranno di far conoscere al Parlamento italiano e a tutti gli italiani come il Veneto ha saputo gestire la pandemia, ma soprattutto come non si è nascosto e si è assunto le responsabilità rispetto alle decisioni che ha preso in

che quella commissione si fece sulla seconda ondata del Covid e si è conclusa con la votazione della vostra maggioranza e non delle considerazioni che dalla minoranza erano state fatte in una apposita relazione.

che quella commissione ha svolto il suo lavoro, è stata presentata una relazione

avrebbero votato a favore dell'emendamento, e non contro. *(Applausi)*. Se in Veneto non avete avuto paura e avete fatto la Commissione d'indagine, non capisco perché qui avete una paura tremenda. Senatore Lisei, qui gli unici ad avere paura di qualcosa siete voi, perché noi vi stiamo dicendo di allargare il perimetro per poter votare tutti a favore.

escludiamo le Regioni, quelle stesse Regioni che poi invece non hanno avuto paura di provare, con tutti i limiti delle loro competenze, a fare un po' di chiarezza. Quindi toglietevi il velo dell'ipocrisia, ammettete che state solo difendendo i vostri Presidenti di Regione *(Commenti)* e votate a favore di una Commissione che includa le Regioni. senatore Romeo, intervengo su questo emendamento solo per dire, da cittadino lombardo, che quando ci è stato chiesto, come Regione Lombardia, di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid, non solo l'abbiamo fatta, ma abbiamo dato anche la Presidenza all'opposizione. Quindi noi di sicuro non abbiamo avuto paura.

non tanto la non conoscenza del Regolamento, quanto una volontà di sopprimere la nostra parola, la nostra verità. *(Applausi. Commenti)*. tale comportamento. Alzatevi pure ad applaudire nuovamente, perché ancora una volta dobbiamo sostenere questo emendamento che hanno sottoscritto tutte le opposizioni, esclusa Italia Viva,

riteneva opportuno anche allargare il perimetro alle Regioni. Ma evidentemente facendo questo e votando contro, sicuramente otterrebbe la Presidenza di questa Commissione. Sta puntando esclusivamente a questo. Lo dobbiamo dire in quest'Aula, perché altrimenti si falsa tutta la discussione. Voglio complimentarmi apertamente con il ragionamento del senatore Franceschini. Franceschini. Lancio un monito a questa maggioranza: il ragionamento del senatore Franceschini è molto importante, perché ha allargato la nostra riflessione, la riflessione di tutti i parlamentari a un pericolo che potrà sorgere potrà sorgere successivamente, e cioè che qualsiasi partito politico domani vinca le elezioni potrà costituire una Commissione d'inchiesta sull'operato del Governo. Allora io chiedo, a questo punto, di istituire in via preventiva la Commissione d'inchiesta sul Ponte dello Stretto di Messina. *(Applausi)*. *(Applausi)*. A questo punto la istituiremo noi la Commissione d'inchiesta sul Ponte dello Stretto di Messina, perché 14 miliardi - scusatemi - sono troppi e li vorremmo dedicare alla sanità pubblica e non allo Stretto di Messina.

attraverso lei, Presidente, hanno sollevato un'altra volta il caso delle Regioni. Hanno detto che la loro Regione ha approvato una commissione d'inchiesta. Ebbene, lo dimostrino su questo emendamento, che richiama la possibilità di aprire alle singole Regioni e alle Province autonome il perimetro di di indagine: sono le Regioni italiane, e non solo la Regione Lombardia, senatore Romeo, come ho già detto. Voglio sapere se anche il Presidente della mia Regione ha agito giustamente, non solo il suo Presidente. Questo lei ce lo sta negando. Quindi, state occultando preventivamente la verità. Questo deve sapere il popolo italiano: state occultando preventivamente la verità.

apprezzare le parole dei senatori Speranzon e Romeo nel ricordare come la Regione Veneto e la Regione Lombardia abbiano istituito delle commissioni di inchiesta, per quanto di ambito Grazie, chiarezza, di mettere a disposizione alcuni dati sui diversi operati delle Regioni. Stamattina - mi dispiace - nel corso della discussione generale

qualche dubbio sulla volontà di agire nella trasparenza a noi viene. *(Commenti)*. Qualche dubbio nella volontà di voler utilizzare

che questa Commissione voglia essere utilizzata con un'altra finalità, dalle parole di alcuni esponenti della maggioranza, a noi può anche venire. Una buona occasione, però, per dimostrare che invece si vuol lavorare nella trasparenza, in un lavoro collettivo, sarebbe quella, appunto, di estendere l'indagine anche alle Regioni. Presidente, io sono lombarda e, nonostante le commissioni e tutto quello che c'è stato, non ho ancora capito perché la Lombardia abbia adottato delle regole diverse, e non dico tanto dall'Emilia Romagna, perché allora sembrerebbe una questione di parte politica, ma dal Veneto. Rispetto alle RSA per esempio, io non ho ancora capito

protezioni siano stati dati tardivamente al personale delle RSA, a differenza delle altre Regioni. Non ho ancora capito perché la delibera in Lombardia sia stata tardiva rispetto a vietare l'accesso ai visitatori, cosa che per esempio Emilia Romagna

al fatto che tutti i presidi di difesa non dovessero essere dati alle RSA, perché erano strutture private, le quali dovevano reperire quei dispositivi da sole, senza tener conto che invece tutti i servizi delle reti sanitarie sono regolati da convenzioni e contratti. E chi più della Lombardia, che ha appunto una sanità anche privata convenzionata, dovrebbe sapere che avviene così? Per quale motivo tutta questa paura nello stabilirlo in questa Commissione d'inchiesta sul Covid che facciamo a livello nazionale, per poi sventolarci il fatto che nelle singole Regioni le commissioni di inchiesta sono state fatte? Se vogliono davvero avere un quadro comune e complessivo, dovrebbero semplicemente consentire l'approvazione di questi emendamenti e fare in modo che tutti noi possiamo lavorare con una cornice completa di tutto il territorio nazionale. Signora Presidente, vorrei motivare le ragioni per le quali sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 il nostro Gruppo si asterrà. asterrà. Vi è ogni tanto la surreale modalità per la quale il dibattito si innesca, con passioni talvolta molto accese, su questioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto degli emendamenti in questione. La discussione di merito, signora Presidente, non riguarda l'opportunità o meno di istituire una competenza rispetto alla singola Regione, né riguarda l'opportunità di coinvolgere le amministrazioni regionali. Essa riguarda, al punto 1, la definizione del perimetro sulla base del quale si è allargata l'emergenza Covid nel nostro Paese. Ora, è di tutta evidenza, avendo l'emergenza nazionale Covid toccato l'intero Paese, per delibere a suo tempo assunte, che appare piuttosto ultroneo o, se preferite, anche ridondante dover specificare e parole «l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale, le altre «e nelle singole Regioni e Province autonome». Si dà per assunto ed è automatico che le Province autonome e le Regioni facciano parte del territorio nazionale. Il testo dell'articolo 1 non esclude l'applicabilità dell'emergenza sulle Regioni. Altro è la competenza delle singole Regioni. Lo dico al collega del MoVimento 5 Stelle che ha parlato in precedenza e che ha eccepito rispetto al comportamento del nostro Gruppo, come se fosse compito di altri Gruppi sindacare le espressioni dei componenti di questa Camera. Altro è l'esigenza di inserire, all'interno della discussione e del perimetro giuridico, l'attività delle singole amministrazioni regionali. Noi abbiamo presentato un emendamento con cui chiediamo di allargare anche alle singole amministrazioni regionali la pertinenza dell'azione della Commissione. Ma appare abbastanza inutile approvare un emendamento che dice che le singole Regioni fanno parte del territorio nazionale, nel momento in cui si definisce che il territorio nazionale è l'intero oggetto dell'applicazione. Altrimenti dovremmo entrare nel merito e dire che dobbiamo coinvolgere anche le Province e i singoli singoli Comuni. Si dà per assodato che il territorio nazionale è uno.

è prima della Lombardia, in particolare la Provincia di Piacenza. Sembra però sempre che la Regione Emilia Romagna sia l'Eden. Per noi va bene, siamo contenti perché siamo emilianoromagnoli, ma purtroppo la nostra Regione è stata colpita tanto quanto la Lombardia.

d'inchiesta, come ha fatto il PD nelle Regioni dove governava il centrodestra. A differenza di quanto è accaduto in Lombardia e in Veneto, dove il centrodestra ha concesso della commissione d'inchiesta alle opposizioni - quindi il PD dove non governa chiede le commissioni d'inchiesta - in Emilia Romagna, dove il PD governa, ha negato la commissione d'inchiesta. d'inchiesta. Noi in Emilia-Romagna non l'abbiamo fatta la commissione d'inchiesta. Aula).* C'è una ragione di coerenza che probabilmente è estranea al Partito Democratico,

Tra le altre cose, evidenzio che il MoVimento 5 Stelle ha votato contro l'istituzione della commissione d'inchiesta in Emilia Romagna, dove è fintamente all'opposizione, ma poi vota sempre col PD. Pertanto, lì dove poteva indagare su quello che ha fatto la Regione Emilia Romagna non lo ha voluto fare,

è evidente che il livello nazionale giudichi il livello nazionale ed è altrettanto evidente che il livello regionale dovrebbe giudicare il livello regionale. se ci fosse coerenza, molto banalmente le Regioni rosse avrebbero concesso le commissioni d'inchiesta dove le opposizioni di centrodestra le chiedevano. Questo non accade perché la coerenza non sapete dove sta di casa.

non riesco a capire la ragione per cui su questo emendamento sia stato dato un parere negativo da parte della maggioranza. Ricordo a tutti - è stato più volte ricordato durante la discussione

le questioni che attengono alle commissioni d'inchiesta delle singole Regioni con quello che stiamo facendo noi. Ma questo è un inciso che serve a parlare di ciò di cui stiamo discutendo in questo momento. Quello che non capisco, però, è perché si dia parere negativo a un emendamento che precisa che con questa Commissione di inchiesta non si affronteranno temi e argomenti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria. Fra i limiti e i rischi che si corrono sempre con le Commissioni di indagine e di inchiesta vi è quello che vi sia una sovrapposizione indebita, che non è consentita, tra le attività delle Commissioni di inchiesta e le attività dell'autorità giudiziaria. Come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, la Commissione d'inchiesta non può indebitamente o surrettiziamente sostituirsi all'autorità giudiziaria. Con l'emendamento in esame, semplicemente, si precisa che questa Commissione d'inchiesta non può avere a oggetto aspetti che sono oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge. Non capisco per quale motivo si dia parere negativo a circoscrivere in modo migliore l'attività di indagine della Commissione di inchiesta e che evita i rischi, che ci sono sempre, di una sovrapposizione con l'indagine dell'autorità giudiziaria. Aggiungo anche, rispetto al dibattito che c'è stato sul tema delle commissioni di indagine fatte nelle singole Regioni, che quelle commissioni non potevano potevano approfondire uno dei temi che non potranno essere approfonditi neanche da questa Commissione d'inchiesta, che è il tema degli effetti che ha avuto sulla gestione di un tema così rilevante come la pandemia la frammentazione dei servizi sanitari regionali. La frammentazione del nostro Servizio sanitario nazionale in tanti servizi sanitari regionali ha prodotto o non ha prodotto effetti anche sulla gestione della pandemia? Questo le singole Commissioni di indagine regionali ovviamente non possono accertarlo. Non potrà accertarlo neanche questa Commissione se non viene ampliato il perimetro anche alle cose che sono state fatte dalle singole Regioni. Ieri ho fatto un esempio degli effetti della frammentazione della risposta nelle singole Regioni sul servizio sanitario regionale, richiamando quello che è accaduto in Regione Lombardia. Quando la Regione Lombardia era sottoposta a una condizione drammatica

perché la Regione Lombardia non era in grado di farlo. Non lo hanno fatto perché non si è stati in grado di superare quella barriera invisibile che c'era tra i servizi sanitari regionali. Questo è un esempio della necessità di allargare il perimetro come noi stiamo chiedendo per rendere davvero utile questa Commissione di inchiesta.

di nessuna indagine, ma siamo fieri di quello che abbiamo fatto in quel periodo difficilissimo, com'è stato detto dai colleghi senatori e senatrici che

tra i compiti che avevamo pensato di dare alla Commissione c'era anche quello di verificare lo stato di attuazione da parte delle Regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale. che questo compito fosse davvero molto necessario. Dopo aver ascoltato le parole del sottosegretario Gemmato, credo che sia addirittura diventato indispensabile, perché forse lo stesso Governo non comprende lo stato in cui si trova il nostro Servizio sanitario nazionale, che è un malato che definirei grave.

così come aveva fatto il *premier* Meloni quando ha illustrato alla stampa, subito dopo l'approvazione della legge di bilancio in Consiglio dei ministri, quanto questo Governo aveva fatto in favore del nostro sistema sanitario nazionale. ha detto che esso mai è stato finanziato così prima di adesso. In realtà, quando abbiamo potuto leggere il testo, abbiamo potuto verificare che i tre miliardi destinati al sistema sanitario nazionale sono, in realtà,

l'innalzamento degli stipendi per gli operatori sanitari (e meno male che si fa). Poi ci sono tutta una serie di altre misure secondarie, tra cui anche l'innalzamento del fondo per le cliniche private, per l'abbattimento delle liste d'attesa.

questi toni trionfalistici saranno un *boomerang*, perché le persone, i cittadini, gli operatori sanitari non ci metteranno molto a comprendere che i servizi erogati nel 2024 saranno inferiori ai servizi erogati nel 2023. *(Applausi)*. Non ci vorrà tanto a capire che, in realtà, con queste risorse si sono tagliate le risorse al Servizio sanitario nazionale di almeno un miliardo rispetto al 2023, almeno un miliardo! E dobbiamo ancora capire, ad esempio, qual è l'effetto dell'innalzamento della spesa farmaceutica sulla questione del *payback*, che è una risorsa per le Regioni. Tutto questo per dire che, siccome noi non abbiamo paura e siccome a voi è utile conoscere lo stato in cui si trova il nostro sistema sanitario nazionale, vi invitiamo ad approvare questo emendamento, che ridefinisce 3 reca i compiti della Commissione

quanto noi dall'inizio avevamo chiesto, anche nell'altro ramo del Parlamento e che abbiamo ribadito oggi in discussione generale. Noi avremmo voluto che la Commissione d'inchiesta fosse estesa anche alle Regioni. Proprio perché non abbiamo paura della verità, vogliamo capire fino in fondo quello che non ha funzionato nella gestione del Covid-19, a tutti i livelli istituzionali. Quindi, con questo emendamento, chiediamo di estendere anche alle Regioni la Commissione d'inchiesta.

per dire che comunque la maggioranza ultimamente si è abituata a far politica usando una propaganda un po' scadente per coprire le proprie mancanze e le proprie lacune.

con la seguente: «svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire, ridurre e mitigare la diffusione e l'impatto dell'epidemia da abbiamo sentite di tutti i colori oggi. Ho sentito che noi non vogliamo assumerci le nostre responsabilità, ho sentito addirittura colleghi del Veneto che rivendicano una commissione che, è vero, è stata istituita in quella Regione, ma al collega Speranzon, che vedo distratto in Aula adesso, voglio dire che in Veneto succedono tante cose, come ad esempio avere un osservatorio osservatorio sui fenomeni criminali e mafiosi che non pubblica annualmente le sue relazioni sul sito della Regione. Una cosa che invece avviene ad esempio in

le motivazioni per cui si va ad indagare anche sulle Regioni, a mio avviso è un grande errore perché in questo modo non facciamo emergere

che non rientrano più in un sistema che gli permette di assistere nel migliore dei modi i nostri anziani. Le RSA oggi non sono più strutture assistenziali, ma sanitarie e probabilmente, raccogliendo dei dati e facendo delle indagini,

avrebbero potuto agevolare e fare il bene dei cittadini.

momento un passo indietro sulle motivazioni per cui è nata la volontà di istituire una Commissione di inchiesta sull'emergenza Covid. Vorrei che si facesse tutti un passo indietro perché temo che al Paese, sulla cui pelle è passata questa pandemia che ha lasciato dei segni per chi non c'è più, per chi abbiamo pianto, per i bambini che hanno vissuto in un periodo surreale e che oggi vivono un disagio da isolamento... *(Brusìo)*. Continuo a sentire brusìo brusìo dalla maggioranza e quindi capisco che probabilmente l'importanza che potrebbe avere questa Commissione di inchiesta in realtà è solo propaganda.

un'eventuale epidemia, che mi auguro non capiti mai in futuro. Lo dovremmo alle vittime della pandemia; lo dovremmo al tessuto sociale dell'Italia; lo dovremmo ai giovani che erano prima seduti sulle tribune e che, secondo me, molto straniti, poiché hanno assistito ad un dibattito in cui sembrava che il ping pong fosse su chi ha responsabilità, chi ha paura di chi, chi ha paura di che cosa. Allora l'invito che farei a tutti è fare un passo indietro e capire che, se veramente da questa Commissione di inchiesta vogliamo ottenere dei dati, delle informazioni che permetteranno in futuro di non commettere gli errori che sicuramente saranno stati commessi a livello nazionale, regionale, delle Province autonome e nei territori, l'occasione è proprio quella di rendere ampio il perimetro della valutazione e dei poteri di questa Commissione. Vorrei veramente un momento di riflessione da parte di tutti per capire che, se dobbiamo utilizzare uno strumento nel rispetto del valore che questo ha nella nostra Costituzione e soprattutto nei confronti dei cittadini italiani, sarebbe il momento di far approvare questo tipo di emendamenti.

Ho sentito alcune cose francamente surreali, come ad esempio dire che a livello regionale si indaga sulle Regioni e a livello nazionale sullo Stato. La tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è materia concorrente e l'indagine deve essere congiunta. Come ho dichiarato durante il mio intervento in discussione generale e a dimostrazione che noi non abbiamo paura di queste indagini, ribadisco che, se questo emendamento passa, noi voteremo a favore del provvedimento. l'approvazione di questo emendamento determina il fatto che voteremmo a favore del provvedimento. Chiedo quindi, per il tramite della Presidenza, posto che questo emendamento ha già avuto il parere contrario del relatore e del Governo: chi è che ha paura di qualcosa?

questo emendamento assume rilevanza particolare soprattutto alla luce dell'andamento delle votazioni sugli articoli precedenti, che chiedevano l'estensione dell'indagine anche alle Regioni. Parto ottimisticamente dal presupposto che questa indagine sia volta a fare chiarezza e a raccogliere dati utili al fine di fare un piano anti-pandemico che tragga beneficio dalle esperienze pregresse. Da lombarda io sinceramente mi chiedo per quale ragione nella mia Regione le persone cadessero morte o malate in misura dieci volte superiore a quello che accadeva nelle altre Regioni. Voglio sapere perché e, come lo voglio sapere io, lo vogliono sapere gli altri lombardi e i residenti delle altre Regioni, che sono stati colpiti dalla pandemia in modo più grave degli altri. Qual è la ragione? E come si fa a fare questa indagine, se non mettiamo a confronto le Regioni, non per andare a cercare un colpevole, ma per imparare dal pregresso e fare meglio nel futuro? Purtroppo questa idea non è stata accolta, forse per paura di un giudizio che in realtà non era previsto. A questo punto il mio emendamento va in un'altra direzione: valutare e verificare se l'inquinamento dell'aria, presente per esempio in Lombardia, sia un fattore che abbia reso la circolazione del virus più veloce, condizionandone quindi la diffusione, e se l'inquinamento dell'aria abbia creato una malattia più seria e più letale nelle Regioni dove c'è questo grado di inquinamento. La mia domanda è: forse si ha paura anche di fare questa verifica? Forse perché la Regione Lombardia è sotto procedura di infrazione UE ed è stata condannata perché non ha fatto nulla per ridurre le emissioni nocive nell'aria? Insisto affinché questo emendamento venga accolto, per fare chiarezza nell'interesse di tutti.

proprio nel bacino padano, che è uno dei territori più inquinati. Non c'è la volontà di non fare quel tipo di intervento, ci mancherebbe altro; possiamo benissimo fare questo approfondimento anche senza approvare questo emendamento. Lo possiamo fare perché nei compiti... quando si vuole, in una Commissione di inchiesta, discutere, valutare e approfondire quello che è avvenuto, nulla vieta che si possano chiamare degli esperti, che hanno magari verificato e fatto degli studi che dicono che il fattore inquinante può essere anche stato un veicolo di trasmissione. Guardi, è anche nostro interesse, perché, se fosse come dice lei, poi non si potrebbe sostenere che siamo stati brutti e cattivi e che abbiamo governato male la Regione, essendoci stato magari un fattore differente. È interessante, è una cosa che si può benissimo fare anche senza approvare questo emendamento, su cui siamo d'accordo, perché, se ci sono degli studi o un approfondimento che possono andare in questa direzione, ciò può essere un motivo valido per farci preparare meglio e soprattutto per chiedere all'Europa maggiori risorse destinate proprio al bacino padano, cosa che l'Europa non prevede, nonostante si sappia che il bacino padano ha delle caratteristiche, di carattere di carattere geografico e quant'altro, che costituiscono un punto debole del nostro territorio proprio sulla questione dell'inquinamento.

No, dico semplicemente che si può fare questo tipo di verifica senza bisogno di votare un emendamento; possiamo benissimo farlo all'interno del contesto. È un tema sensibile, su cui diamo

Solo per sottoscrivere questo emendamento e per dire per suo tramite al senatore Romeo di far pace con sé stesso. Se è favorevole all'emendamento, lo approvi e non lo bocci, altrimenti non torna. Se è favorevole,

Presidente, intervengo anche per permettere a coloro che assistono ai nostri lavori di comprendere quello che stiamo facendo.

Signor Presidente, intervengo a proposito dell'emendamento 3.40, con riferimento poi anche all'emendamento 3.44. Lo sottolineo perché centrali fra quelle che sono state proposte dalla maggioranza per avviare l'indagine, cioè la necessità di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti, quindi delle decisioni che sono state prese rispetto alla pandemia. È evidente che per fare un'effettiva valutazione di tutto questo è necessario capire se ciò che veniva determinato dai DPCM e dalle decisioni del Governo avesse coerenza poi nelle Regioni e altrettanto tempestiva applicazione, perché se poi lì creava il problema, è evidente che non avremmo una relazione effettiva. Credo quindi che sia utile valutare questi due emendamenti per per dare il significato che qualcuno della maggioranza oggi ha cercato di sostenere che l'obiettivo sia davvero quello di comprendere cosa è successo e non costruire un processo.

**Il Senato non approva**.

«a verificare con attento monitoraggio nelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali quali siano state le attività di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni

un aiuto. Abbiamo assistito a un intervento molto importante del Sottosegretario alla salute, che ci ha spiegato il mondo dei sogni dalla legge di bilancio in avanti. E, quindi, sostanzialmente avremo la possibilità attraverso la Commissione di inchiesta di verificare tutti quei potenziamenti che, grazie alla prossima legge di bilancio, ci saranno. Avremo altresì la possibilità di verificare quali mancanze ci sono state nei diversi sistemi sanitari regionali. Mi chiedo perché il relatore e il Governo sono contrari a impegnarsi a fare una cosa che emergerà dalla Commissione. Per quale motivo?

lei mi ha chiesto aiuto, ma il mio parere non è previsto dal Regolamento. Quello dei relatori e del Governo resta contrario. Trovo le sue parole ragionevoli, ma è una mia opinione personale che non ha alcuna valenza.

"andrà tutto bene" era il *refrain* che tutti ricordiamo caratterizzare le scuole, gli ospedali, le finestre e i balconi del nostro Paese in quei drammatici mesi del 2020, nei quali siamo stati sorpresi dalla pandemia da SARS-Covid 2019. Trattavasi probabilmente di una sorta di *training* autogeno inventato ad arte, di autosuggestione e di speranza che le cose non peggiorassero. Ma - come tutti drammaticamente sappiamo - non è andata affatto bene: *in primis,* perché lo stato di emergenza fu emanato dal Governo in sordina già il 27 gennaio 2020, conscio che dalla Cina l'epidemia si stava espandendo in Italia, ma scoperto dalla politica solo molto dopo e solo grazie all'incubo nel quale siamo piombati dopo che a Codogno, da un'eccellenza della nostra medicina e della nostra sanità, fu individuato il famoso paziente zero; *in secundis*, perché sono indelebili nel nostro cuore e nella nostra mente il batticuore e la tachicardia che ci caratterizzava innanzi al *countdown* quotidiano dei contagi e dei morti, che solo nel 2020-2021 ammontavano a 160.000 anime. Chi può dimenticare la sfilata delle bare di Bergamo scortate dai nostri encomiabili militari che, insieme a medici e infermieri, sono stati la colonna vertebrale *(Applausi)* di un Paese piombato nell'ora più buia, come ammise lo stesso *Premier* di allora. un grazie non è stato nulla innanzi al loro impegno, alla vita che in molti hanno consacrato alla causa per garantire la nostra vita: un esempio di moralità e di abnegazione che ad oggi aspetta ancora un riconoscimento concreto dalla politica e del quale tutto il Parlamento si deve sentire responsabile. Innanzi a tutto questo patrimonio di dolore, ma anche di resilienza di un Paese straordinario, e l'abbiamo detto in molti oggi; innanzi al venir meno delle garanzie costituzionali e della salute pubblica, all'evidente necessità dell'allora Governo di commissariare le libertà costituzionali, per quale motivo - mi chiedo - non cercare di capire le cause, gli errori, se ci sono state illegalità o magari anche virtuosismi - certo, perché ci sono stati anche virtuosismi - sconosciuti però in quei mesi invernali? Perché qualcuno non vuole questa doverosa Commissione d'inchiesta che dobbiamo a quei morti, ma anche ai tanti vivi che ancora stanno pagando quell'enorme esborso di denaro pubblico? Perché qualcuno ha paura della verità, come titolava oggi un noto quotidiano, forse non a caso? Capire cosa è successo durante la pandemia è un servizio che la politica deve al Paese, deve agli italiani, anche perché troppo spesso capita che nel nostro Paese, *ad usum Delphini*, la memoria storica sia molto breve. Noi, al contrario e per fortuna degli italiani, abbiamo la memoria lunga. Da quando il Governo Conte ha ammesso di non essere affatto pronto - come dichiarato viceversa qualche giorno prima in TV - e ha debuttato con il sistema delle solenni e un po' inquietanti conferenze stampa di emergenza nazionale, è iniziato il periodo tra i più tristi della storia della nostra Nazione. Non è colpa di nessuno, è colpa di quello che è accaduto nel mondo. Lo staremo a vedere, ma non dobbiamo nasconderci. Ce li ricordiamo bene quei momenti, quei giorni di silenzio per le strade, interrotti solo dal rumore delle sirene e dei mezzi di soccorso; così come ricordiamo la sofferenza e il dolore di quei momenti, specie di quelle famiglie che addirittura non hanno potuto salutare i loro cari, morti da soli, senza la *pietas* necessaria al defunto, perché le regole lo impedivano e in tanti, troppi, non hanno avuto questa opportunità. Quel dolore, Presidente, ancora oggi non si cancella e mai si cancellerà. *Last, but not least* - come direbbero gli inglesi - come non ricordare le centinaia di imprese che hanno lavorato garantendoci la sussistenza innanzitutto alimentare, nonostante i rischi per la loro salute, e quelle purtroppo costrette, viceversa, a chiudere e i danni economici e sociali incalcolabili incalcolabili avutisi, i suicidi relativi all'impossibilità di proseguire il proprio lavoro? Come dimenticare questa drammatica situazione, questo bollettino di guerra, nonostante l'Italia sia lo Stato che ha applicato le misure più restrittive di tutte le Nazioni? Rivolgo quindi una doverosa domanda a tutti noi, Presidente, che poi è il motivo dell'istituzione di questa Commissione: siete e siamo davvero sicuri, in coscienza, che sia andato tutto come doveva andare, che sia andato, appunto, tutto bene? Allora, colleghi, ai futuri commissari spetterà il compito non certo facile di verificare ogni aspetto della pandemia, come i motivi motivi per cui il Piano pandemico del 2006 non fosse mai stato aggiornato dai vari Governi, e i motivi per cui, una volta aggiornato, non sia stato attivato. Si poteva magari guadagnare tempo e salvare vite umane. Ai commissari spetterà il compito di indagare, ad esempio, la relazione dell'Italia con l'OMS e i motivi per cui sia stato ritirato il rapporto pubblicato, con cui si diceva che l'Italia non era pronta. Così come sarà doveroso verificare perché, mentre scoppiava la pandemia, l'Italia regalava milioni di mascherine alla Cina - è stato detto più volte, ma è bene ripeterlo - mandando i nostri medici a combattere contro il *virus* a mani nude. Alla Commissione spetterà poi verificare il perché della presenza dell'esercito russo nel nostro Paese, visto quello che è accaduto dopo, vista la guerra che oggi caratterizza l'Europa a mano della Russia. Spetterà inoltre verificare doverosamente i contratti di appalto, i soldi spesi per i vaccini, per i centri vaccinali, le famose primule del Commissario straordinario, l'app Immuni, i banchi a rotelle, che forse possono dar fastidio a qualcuno, ma francamente nelle scuole io non li ho mai visti e vengo dall'Alto Adige, dove c'è una grande spesa economica in merito e sono sempre all'avanguardia. Occorrerà verificare tutto, anche gli eventuali effetti avversi da vaccino. Lo dice una che si è vaccinata e lo rifarebbe perché crede nella scienza, ma qualcuno vorrebbe che restassero un tabù. Dobbiamo istituire questa Commissione, perché lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che hanno perso un loro caro e lo dobbiamo a tutti gli italiani, non certamente ai colleghi per utilizzare la Commissione d'inchiesta come un tribunale, come avete voluto far credere voi dell'opposizione, o come un plotone di esecuzione, come la clava politica da utilizzare contro qualcuno o contro l'attuale opposizione, come dalla stessa, appunto, denunciato. Sulla Commissione di inchiesta vogliamo infatti il rispetto delle persone, il rispetto del lavoro dei sanitari, che sempre tutti noi abbiamo chiamato eroi, come persone in prima linea che hanno fatto più di quello che competeva loro da un punto di vista professionale. Non solo hanno seguito i malati, ma hanno cercato umanamente di dare loro vicinanza e conforto, ancora una volta senza gli strumenti, in una sorta di preistoria sanitaria inconcepibile per un Paese civile e moderno. Abbiamo il dovere, colleghi, di ricordare che cosa è avvenuto e le ragioni per cui è avvenuto. Ecco perché è di fondamentale importanza - anzi si è già in colpevole ritardo - istituire la Commissione, soprattutto per evitare che tutto possa accadere di nuovo; per riuscire a intervenire adeguatamente in futuro e rispondere prontamente alle esigenze che si potranno manifestare. Farlo attraverso una Commissione vuol dire peraltro far tornare protagonista il Parlamento e la politica, cioè la nostra democrazia, che appunto è parlamentare e ogni tanto dovremmo ricordarcelo. L'istituzione della Commissione, quindi, è un atto di giustizia, di ripristino delle libertà costituzionali. È un atto di verità con la "V" maiuscola. Concludo e chiedo, Presidente, cosa c'è mai da temere se da sempre è stato assicurato che tutta l'azione del Governo dell'epoca, e anche di quello successivo - non era solo il Governo Conte, ricordiamolo, ma anche il Governo Draghi - appoggiato per lo più da tutti noi, è stata compiuta in assoluta trasparenza? Male non fare, paura non avere, recita un famoso proverbio. Come mai, dunque, improvvisamente questa trasparenza non la si vorrebbe più, e proprio dalla democrazia parlamentare? Crediamo quindi che sia importante istituire la Commissione d'inchiesta, con le precise finalità elencate e con l'obiettivo alto e nobile di crescere come Paese. Tutti insieme dovremmo volerla, come coscienza collettiva di crescere come istituzioni. Con il Governo Meloni è finita quell'Italia in cui uno fa una scelta, ma non se ne assume la responsabilità politica. È finito quel tempo: lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dai banchi del Governo, il 25 ottobre, quando ha preso l'impegno solenne con gli italiani di costituire questa Commissione. Noi Civici d'Italia, Noi Moderati, UDC, Coraggio Italia, MAIE, insieme a tutta la coalizione unita del centrodestra di Governo, vogliamo arrivare alla verità,

Signor Presidente, Governo, colleghi, innanzitutto una premessa che fa il Gruppo Per le Autonomie: noi ci riconosciamo pienamente nell'intervento che il senatore Casini ha fatto all'inizio di questo pomeriggio. Ringrazio la senatrice Pirovano per il suo intervento accorato e appassionato, da sindaco, di cui approvo i contenuti, ma non le conclusioni. Spiego perché. Il Senato e la Camera dei deputati hanno il compito di tracciare la via per l'Italia del futuro, fondata su quanto di buono è stato fatto e sulla rielaborazione degli errori commessi. Cosa ci ha lasciato di buono l'esperienza Covid? Certamente l'abnegazione dei sanitari e la disponibilità dell'intera popolazione a sacrificarsi collettivamente per un interesse superiore: la salute di tutti. due mattoni importanti, su cui costruire l'Italia del futuro. La Commissione proposta saprà tenerne conto e valorizzarli? Ho dei dubbi, grossi dubbi. Premessa: è evidente che, in quella situazione concitata e complessa, siano stati commessi degli errori. La giustizia è stata coinvolta e farà il suo corso, per accertare eventuali reati e responsabilità. Ma ho il dubbio che questa Commissione finirà soprattutto per sollevare molta polvere su chi ha salvato l'Italia. Ho il dubbio che, attraverso questa Commissione, qualcuno intenda riscrivere a posteriori la storia. Ho il dubbio che questa Commissione finisca per essere un tribunale politico per mettere sul banco degli imputati i precedenti Governi e le forze politiche che ne hanno fatto parte. Ho il dubbio che questa Commissione vada a calpestare anche solamente l'idea di una memoria condivisa, per lasciare spazio, secondo un malcostume diffuso in Italia, a due memorie contrapposte. Ho il dubbio che questa Commissione faccia carta straccia dello spirito di unità nazionale che animò quelle settimane, soprattutto le prime settimane, per trasformare la memoria della pandemia in un elemento di battaglia politica, la più infima, perché fatta su una vicenda che ha generato lutti, dolori e immani sacrifici. Presidente, se si vuole davvero onorare la memoria di quello che è stato, bisognerebbe dimostrare di avere capito la lezione e remare tutti quanti per alzare le risorse a favore della scienza, della ricerca e della sanità pubblica. Invece - si noti bene - la legge di bilancio che fra qualche tempo approderà in quest'Aula mette mano alle pensioni dei medici (e non solo), che sono coloro che hanno, in alcune circostanze e in quella Se fossimo davvero capaci di guardare avanti e con un approccio obiettivo, forse andremo anche a vedere a chi

Paese, grazie alle enormi doti del suo sistema produttivo, è quello che ha saputo reagire di più alle ripercussioni economiche, diventando quello con la maggior crescita in Europa al momento delle riaperture.

Per concludere, signor Presidente, la pervicacia con cui l'attuale maggioranza di Governo continua a ripetere che chi c'era prima ha sbagliato tutto inquieta perché non porta a nulla, se non a costruire un consenso elettorale farlocco. Tutti i Governi hanno contribuito, quale più quale meno, a far crescere il Paese e tutti avevano le migliori intenzioni di migliorarlo. Sarà la storia, e non certo il Governo successivo, a stabilire chi ha fatto bene e chi ha fatto meno bene. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto contrario alla nascita di questa Commissione

devo dirlo con grande franchezza - anche con una certa animosità da un certo punto di vista, anche perché è un problema che mi tocca molto da vicino.

aveva mai provato nella propria esperienza di vita. Penso che non dovremmo avere timori a fare una discussione a 360 gradi su cosa è accaduto

rispetto all'insieme del Paese? Intendo dire che probabilmente per il livello di industrializzazione, di inquinamento, di concentrazione, di consumo di suolo, per l'aria che respiriamo la malattia

Il problema è la natura della Commissione, è il modo in cui viene fatta che - secondo noi - è anticostituzionale. Ed è per questo che non siamo d'accordo e abbiamo presentato una questione pregiudiziale.

è chiaro che è già scritto come andrà a finire. Se invece volete smentirci, comportatevi, come si usa dire, in modo corretto e fate un'indagine, perché poi

chi ha ascoltato il dibattito di ieri e di oggi è sicuramente felice, nonostante gli scontri, perché abbiamo avuto modo di entrare nel merito di uno dei punti più qualificanti l'accaduto degli ultimi anni. La pandemia non è stato un evento come gli altri: ci ha profondamente cambiato. Chiedere di conoscere la verità non è andare contro la Costituzione o contro l'altra parte politica, ma il tentativo di imparare per il futuro. Certo, cosa sia la verità è tema complesso (Ponzio Pilato se lo domanda nell'interrogatorio a Gesù: «*Quid est veritas*?») e nell'era in cui stiamo vivendo, quella della post-verità, è molto difficile poterne individuare i paletti. Noi del nostro Gruppo abbiamo chiesto la Commissione d'inchiesta nella primavera del 2020, abbiamo fatto una petizione nel gennaio del 2021 con migliaia di firme, abbiamo posto questo tema nella campagna elettorale del 2022 e abbiamo coerentemente votato a favore alla Camera dei deputati nel 2023, quindi ovviamente votiamo a favore. Vorremmo però tentare di fare un ultimo sforzo ascoltando le ragioni degli altri. Ringrazio, tra gli altri, il senatore Magni, da cui mi dividono tante cose, ma di cui apprezzo la sincera *verve* democratica e la passione civile. Proviamo a capire perché abbiamo questa opinione: credo infatti che sia utile ascoltarsi, per cercare di andare fino in fondo a capire le ragioni. Parto dal primo tema, la scuola: se n'è parlato poco nel dibattito. L'OMS dice che il nostro Paese è quello che ha chiuso le scuole più di tutti gli altri. La pandemia c'è stata dappertutto: da noi, 341 giorni di chiusura, dice l'OMS; 138 giorni in media dalle altre parti. E a questo fa da contraltare - sarà un caso, per carità di Dio

Vogliamo prenderne atto o vogliamo far finta di niente? Il Covid c'entra qualcosa o no? Ci basta la battaglia che ha fatto, tra gli altri, il collega Sensi sul *bonus* psicologo o possiamo capire che forse la chiusura delle scuole ha inciso sulla depressione dei nostri ragazzi? Vogliamo parlarne in modo serio o bisogna buttarla tutta in politica contro Conte, Speranza, Fontana e Zaia?

è una delle conseguenze della pandemia e delle chiusure scolastiche. Lo dico perché nel marzo del 2020 chiesi di riaprire le scuole e tanti di quelli che sono qui - di sinistra, ma anche di destra - mi insultarono, dicendo che ero pazzo. Alcuni presunti esponenti tecnici del comitato tecnico scientifico fecero uscire una velina il giorno dopo, dicendo che, se si fossero riaperte le scuole, si sarebbero avute 151.000 persone in terapia intensiva a giugno, una baggianata del tutto non scientifica. Signor Presidente, votiamo a favore della Commissione perché si faccia tesoro degli errori e dell'utilizzo propagandistico che qualcuno ha fatto del comitato tecnico scientifico e del fatto che un Paese che non pensa alle scuole e ai danni sui suoi ragazzi è miope. Vengo al secondo punto di discussione: i ristori. Onorevoli colleghi, visto che il clima si è rasserenato in Aula, come forse qualcuno di voi si è accorto, mi capita talvolta di fare qualche conferenza all'estero, con grande entusiasmo delle altre forze politiche. Perché vi dico questo? Perché io ho ricevuto l'invito a recuperare dai ristori, nel pieno della pandemia, 21.000 euro.

ma con quale criterio lo Stato dà i soldi a Matteo Renzi? O, perlomeno, permette a Matteo Renzi di chiedere 21.000 euro, quando ci sono ristoranti, botteghe artigiane, aziendine, che non hanno visto un centesimo o che hanno avuto necessità di restituire i soldi con dei tempi sbagliati? Vogliamo dire che sulla gestione dei ristori altri Paesi hanno gestito la vicenda meglio di noi? O pensate che sia un'offesa? Terzo punto: gli acquisti. È mai possibile che un ex Presidente del Consiglio dei ministri (non scelto di essere il garante della vendita dei ventilatori cinesi, per di più malfunzionanti (ogni riferimento a Massimo D'Alema è voluto), che lo abbia fatto senza alcun ruolo istituzionale? È mai possibile che ci fosse un unico soggetto, il commissario Arcuri, il cui mandato andava dalla gestione di Invitalia, fino alla gestione delle mascherine e a quella delle primule, sui vaccini? È un sistema che funziona questo, sì o no? *(Applausi)*. Per me non funzionava; tanto è vero che poi è arrivato Draghi, hanno cambiato il sistema, al posto di Arcuri è arrivato Figliuolo e le cose, secondo me, sono migliorate. Poi qualcuno può dire di no. È legittimo, ma lo capite che, su un tema del genere, non fare chiarezza non significa difendere una parte politica? Non fare chiarezza significa offendere il nostro futuro. Arrivo

Qualcuno di noi c'è stato, sa che è una cosa seria. Qualcuno ci ha scritto libri. Ma vi sembra normale che la comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi, nel momento di massima tensione, quando tutta Italia era chiusa in casa, quando si annunciavano le dirette e poi si stava un'ora e mezzo ad aspettare che la diretta partisse, passasse dalla pagina personale del *leader* politico e non dai canali istituzionali? Che sottigliezze, mi si risponderà. Invece no! Perché da questo modo proprietario di concepire la comunicazione istituzionale, qualcuno ha tratto un vantaggio politico e ha lucrato un vantaggio politico che continua ancora adesso. *(Applausi)*. Dare delle regole di decenza istituzionale nella comunicazione politica, che sono mancate all'atteggiamento del presidente Conte e del portavoce Casalino, è un fatto di etica delle istituzioni. Quando arriva il vaccino, non si fa la diretta col camioncino che arriva al Brennero per poi dimenticarsi di fare il piano vaccinale! Perché il piano vaccinale, quando il Governo se n'è andato, era rimasto fermo. Ancora, potrei continuare. È mai possibile che questo Parlamento non discuta delle azioni di un Presidente del Consiglio?

È mai possibile che il Presidente del Consiglio parli con Putin e, per gestire una epidemia che diventa pandemia, chiami i soldati dell'esercito russo? Ma chiama i medici, se vuoi gestire una pandemia. *(Applausi)*. Io non ho mai visto una pandemia gestita dai soldati russi. E potremmo continuare a lungo, sul tema dei vaccini, sul comitato tecnico. Io ho fatto una battaglia, contro parte della destra e contro tutto il MoVimento 5 Stelle, che in quest'Aula, con la senatrice Taverna, urlava contro i vaccini e contro di noi. Io sono sempre stato dalla parte dei virologi e della scienza. Proprio per questo non ho paura a confrontarmi, perché chi crede nella scienza non ha alcun problema a guardare i dati sui vaccini e a verificare come questi abbiano contribuito a sconfiggere malattie. C'è un ultimo punto e poi vado alla conclusione; in quest'Aula si parla di deriva autoritaria. Tutte le volte che c'è una riforma costituzionale c'è una deriva autoritaria. Io non ci credo. È mai possibile che si sia derogato alle norme costituzionali più importanti e ai diritti fondamentali con un DPCM? *(Applausi)*. Io ero d'accordo. Io ero d'accordo. Ma vi rendete conto che c'è un sistema istituzionale in cui basta un DPCM? Oggi c'è un motivo solido e nobile. È normale che basti un DPCM per derogare la prima parte della Costituzione? Su questi temi, signor Presidente del Senato, bisogna fare chiarezza e siccome bisogna fare chiarezza, noi votiamo convintamente a favore, ma vi diciamo in conclusione due cose. La prima, con tutto l'affetto per il presidente Casini: questa Commissione si può non fare come le altre si possono non fare. Allora si abbia il coraggio di cancellare l'articolo 82 della Costituzione e si dica che il Parlamento, per le considerazioni che Casini ha espresso, deve essere privato del diritto di fare Commissioni. Se però c'è l'articolo 82, se c'è un punto sul quale il Paese ha diritto di conoscere come sono andate le cose per il futuro, quello è il Covid. Lo sta facendo tutto il mondo, non lo sta facendo Bolsonaro che non c'è più. La Commissione europea ha fatto e sta facendo una commissione di inchiesta sul Covid, la cui relatrice per il Partito socialista europeo è l'onorevole Moretti. Non raccontiamo allora che soltanto qui si fanno queste cose. una battuta: siccome ho ascoltato il dibattito e mi è piaciuto molto, quando ha parlato molto bene la senatrice Sbrollini, il mio amico senatore Patuanelli ha fatto polemica contro di lei dicendo che noi abbiamo un'ossessione nei confronti di Giuseppe Conte. Non dirò Patuanelli di stare sereno per evidenti ragioni, ma vorrei rassicurarlo sul fatto che questa ossessione noi l'abbiamo curata quando abbiamo mandato a casa Conte per portare Draghi. *(Applausi)*. Abbiamo un'altra ossessione: dire la verità al popolo italiano su quello che è accaduto. L'abbiamo promesso nel 2020, lo abbiamo detto agli elettori, lo abbiamo votato alla Camera, lo facciamo anche al Senato, a testa alta e viso aperto. Presidente, ci sono momenti come questo in cui tutti dovremmo chinare il capo davanti a chi oggi non c'è più; per loro, per le loro famiglie abbiamo il dovere e la responsabilità di rivisitare il percorso dal quale non possiamo e non vogliamo deviare senza dimenticare che il subdolo aggressore che ci ha colti impreparati, resi impotenti e piegato ha un solo nome ed è Covid. Ci sono tuttavia svariate strategie per affrontare un avversario. Come si è introdotto l'avversario nelle nostre vite? Eravamo preparati? Abbiamo agito con tempestività? Abbiamo preso alla leggera l'assalto? Quali strumenti abbiamo impiegato per contrastarlo? Sono queste le domande alle quali vogliamo e dobbiamo dare delle risposte attraverso l'istituzione di questa Commissione parlamentare di inchiesta, che non vuole essere uno strumento per sostituirsi alla magistratura, come ci ha ricordato anche giustamente il Presidente della Repubblica, e perché i ruoli non vanno confusi. Non vuole essere neppure un plotone di esecuzione o un'inquisizione politica, come ha detto Giuseppe Conte, perché, vedete, per noi di Forza Italia, mai processi politici è un principio che vale sempre, non solo quando fa comodo. *(Applausi)*. Presidente, lo dico a chi, anche qui in Aula, è abituato a fare i processi di piazza o che ha fatto politica sempre e solo con i processi di piazza. Ecco, questa Commissione non dovrà seguire il loro esempio. Possiamo però interrogarci sul perché in Italia ci sono stati più morti che nel resto d'Europa senza che questo diventi un terreno di scontro politico? Dare risposte ai cittadini per noi è un atto di onestà e di responsabilità perché molte pagine sono poco chiare, sono piene di *omissis*, molti comportamenti lasciano più di qualche dubbio e molti interrogativi sono rimasti inevasi. Voler insabbiare tutto, lasciar segreto ciò che segreto non doveva essere, vuol dire al contrario offendere la memoria dei morti e il diritto di sapere dei vivi. C'è una cosa sola che deve guidare tutti noi: la ricerca della verità. Sostenete di aver agito nel massimo rispetto delle regole, senza commettere errori e che tutte le scelte erano giuste, in buona fede. Non abbiamo motivo di non credervi, ma allora cosa cosa temete? Gli emendamenti che avete presentato sono purtroppo rivelatori, perché tentate di tenere la polvere ben nascosta sotto il tappeto; anzi, peggio, di scaricare le responsabilità sulle Regioni, assolvendo il Governo di allora; quelle Regioni che per mesi avete lasciato a combattere mani nude, perché chi era al Governo non decideva *(Applausi)* e quando lo faceva era sempre troppo tardi. Erano le Regioni a chiedere con forza l'istituzione delle zone rosse. Era il Governo Conte II - tutto il Governo, senatore Renzi - a non decidere o, peggio, a negare, in un *mix* di responsabilità politica, ottusità burocratica e anche contabile. Questo ce lo dobbiamo dire. Nel frattempo, mentre a Roma andavano in scena le conferenze e si andava avanti a colpi di DPCM, nel resto del Paese a lavorare erano i sindaci, lasciati da soli in trincea ad affrontare la crisi sanitaria, a preoccuparsi della popolazione, a rassicurarla, anche utilizzando creatività e fantasia: si sono improvvisati tante cose, anche volontari e psicologi. Eppure tutti, anche tra le vostre fila, dovrebbero avere interesse a fare chiarezza su una pagina, la più drammatica forse dal dopoguerra ad oggi: perché la mancanza dell'aggiornamento del piano pandemico, la sua mancata attuazione dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica da parte dell'OMS, non è stata oggetto di valutazione da parte della *task force* istituita dal Ministero della salute? Perché il presidente del Consiglio Conte alla fine di gennaio 2020 parlava di situazione sotto controllo e sosteneva di aver attivato tutti i protocolli di prevenzione? È giusto sapere quali informazioni fossero alla base della sicumera, supportata dall'allora segretario del PD Zingaretti, che ostentava sprezzante serenità bevendo spritz in compagnia, al grido di "Milano non si ferma"? Ecco, è corretto per noi e non c'è bisogno di chiederci se sia giusto o meno. Secondo noi, non è soltanto lecito, ma è doveroso indagare su eventuali abusi, sprechi, speculazioni e comportamenti illeciti. Questi diventano ancora più gravi quando sono commessi alle spalle degli

risultati difettosi - quando si riuscivano ovviamente a trovare - pagati a caro prezzo dallo Stato italiano e dai cittadini ovviamente; la nomina del commissario straordinario per l'emergenza Arcuri; i verbali secretati; i banchi a rotelle - mi spiace dirlo - per garantire il distanziamento sociale nelle classi. Mi rendo conto che avete un nervo scoperto, colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma

(100 milioni per la gestione del sistema di allerta per i contagi), scaricata solo dal 2 per cento, con pochissime notifiche, a fronte di migliaia di casi riportati dai bollettini ufficiali giornalieri. il piano vaccinale - che mancava - mentre avevamo i cartonati a forma di primule, costate ben 345 milioni. *(Applausi)*. Per non parlare infine dei nostri figli, che hanno pagato un prezzo altissimo per la schizofrenia del Governo del tempo. Quando tutta l'Italia era ancora aperta, le scuole sono state le prime a chiudere, anche se efficienti sotto il profilo della della sicurezza. Quando il Paese ha ricominciato a vivere una parvenza di normalità, questa è stata negata agli studenti, rimasti con la didattica a distanza: è stata una scelta che ha provocato danni enormi ai nostri ragazzi, soprattutto dal profilo psicologico.

condividere. Non può essere un comodo lavacro, perché criticare senza far nulla significa essere complici. Nessuno in quest'Aula e nel Paese può credere che il senatore Renzi non esercitasse un'importante ruolo decisionale in quel Governo e aver contribuito all'arrivo di Draghi - sicuramente lui si vanta di averne il merito può lavare la coscienza, ma non toglie la responsabilità di aver fatto parte di quella maggioranza che lui aveva voluto e che ha preso quelle decisioni. Voglio essere molto chiara anche su un altro punto: nessuno provi a usare questa Commissione in modo strumentale contro quella che fu la svolta che ci ha permesso di uscire dal tunnel e di sopravvivere. Forza Italia non mette, né metterà mai in discussione la scienza e la decisione di rendere obbligatori i vaccini che ci hanno salvato la vita *(Applausi)*, impedendo molte più vittime e contagi e scongiurando conseguenze peggiori. Ma certo qui si vuol far chiarezza anche su come è stata gestita la campagna vaccinale, con particolare attenzione, ovviamente, per i soggetti più fragili, perché con la scoperta dei vaccini a tempo di record era fondamentale che l'immunizzazione degli italiani fosse la più rapida ed estesa possibile. L'arrivo del generale Figliuolo, per fortuna e solo grazie a lui, ha dimostrato quanta improvvisazione e incompetenza ci fosse stata prima. In definitiva, questa Commissione d'inchiesta cerca risposte, vuole squarciare il velo del silenzio, vuole capire come siano stati gestiti gli enormi poteri garantiti dallo stato di emergenza, ma soprattutto dobbiamo capire cosa non ha funzionato, perché bisogna fare in modo che se dovesse un'altra pandemia, speriamo mai, questo Paese non ricada negli stessi errori. *(Applausi)*. Lo dobbiamo alle nostre vittime, a quelle bare di Bergamo portate via dai camion militari, ai tanti che hanno perso i loro cari senza neanche poter dare loro l'ultimo saluto. Lo dobbiamo al personale sanitario, ai medici che hanno sacrificato la loro vita per salvare la nostra. Lo dobbiamo a tutti noi, perché tutti abbiamo sofferto in un modo o nell'altro i colpi del Covid. Lo dobbiamo all'Italia e lo dobbiamo al diritto di verità. Per questo motivo annuncio il voto favorevole alla Commissione d'inchiesta da parte del Gruppo Forza Italia.

per due anni il nostro Paese ha combattuto una guerra, una guerra contro un nemico invisibile, ma un nemico spietato. Lo ricordava chi mi ha preceduto: un nemico che ha fatto nel mondo 7 milioni di morti, 770 milioni di contagiati. Una guerra che noi abbiamo combattuto in trincea: noi come istituzioni, come Parlamento che non si è fermato un solo giorno, il Governo. L'hanno combattuta in trincea, gli operatori sanitari e tutti gli operatori dei servizi essenziali, che hanno combattuto soprattutto nei primi tempi a mani nude, affrontando la morte con coraggio questa trincea l'hanno occupata soprattutto i malati, i malati delle terapie intensive, i malati che aspettavano insieme agli operatori sanitari per ore nelle ambulanze per accedere ai pronto soccorso. Noi questa guerra però l'abbiamo dovuta affrontare con poche armi, con armi spuntate, a causa dei tagli che erano stati perpetrati per dieci anni, dal 2008 al 2018, al nostro Servizio sanitario nazionale. Erano stati sottratti al Fondo sanitario nazionale ben 37 miliardi di euro. Avevamo perso 71.000 posti letto: infatti, in terapia intensiva c'erano solo 5.000 posti ad inizio pandemia, che abbiamo dovuto raddoppiare in pochissimo tempo; 46.000 medici e infermieri già allora avevano lasciato il Servizio sanitario nazionale pubblico per andare a lavorare nel privato e non avevamo armi, anche perché c'era stata una riforma nel 2001 che aveva trasferito la gestione della sanità alle Regioni e quindi avevamo venti sistemi sanitari regionali che lavoravano in modo diverso. Allora in questa guerra in trincea, senza armi, noi abbiamo scelto il faro più luminoso che ci fosse, che era la scienza. Per la prima volta la politica ha preso delle decisioni seguendo un metodo scientifico, leggendo i dati, guardando i risultati degli studi, interpellando la comunità scientifica. Io sono orgogliosa e sarò riconoscente a vita a tutti i membri del comitato tecnico-scientifico, che gratuitamente con generosità hanno lavorato per due anni a disposizione delle istituzioni. Sono riconoscente al Consiglio superiore di sanità e al suo presidente Locatelli, così come sono riconoscente all'Istituto superiore di sanità e al suo presidente Brusaferro, che per la prima volta davvero ringrazio in quest'Aula per il lavoro che hanno fatto. *(Applausi)*. Così come chiaramente ringrazio il Governo di allora, il ministro Speranza e anche le Commissioni sanità, di cui molti di noi facevano parte. Senatore Zaffini, lei sicuramente lo ricorda. Grazie a quel lavoro, che abbiamo fatto seguendo la scienza, siamo riusciti a diventare un modello per gli altri Paesi europei che hanno affrontato dopo di noi la pandemia e per la comunità internazionale. L'ha riconosciuto l'Organizzazione mondiale della sanità. In quei mesi, in cui noi prendevamo quelle decisioni e leggevamo quei dati, le debolezze del nostro Servizio sanitario nazionale sono apparse da subito chiarissime. chiarissime. Queste debolezze erano il definanziamento (ma evidentemente questa lezione non l'avete imparata, perché tornate a tagliare in sanità), il blocco delle assunzioni, per cui c'era carenza di personale (quel tetto è ancora vigente e non lo state superando), e un filtro territoriale totalmente inesistente. Infatti abbiamo scritto un PNRR che aveva, nella Missione 6, proprio la rete territoriale che voi state depotenziando, togliendo ben 700 milioni alle case di comunità e agli ospedali di comunità. Soprattutto a voi non è chiaro che la disomogeneità nella gestione della sanità è un danno. Non è chiaro perché state ulteriormente potenziando questa gestione regionale, con l'autonomia differenziata che, nostro malgrado, ci troveremo a brevissimo addirittura a discutere in quest'Aula. Vi chiedo quindi perché continuate a voler cancellare la storia, perché questa deve essere l'ennesima occasione mancata in cui, anziché fare un lavoro a beneficio del Paese, utilizzate, come siete bravi a fare, la politica e queste Aule solo per fini elettorali o per attaccare chi c'era prima di voi. Siete bravi a speculare sulle tragedie; quelle piazze che voi usavate come palchi, quelle piazze affollate di negazionisti e complottisti, che gridavano alla dittatura sanitaria. Mi ricordo i vostri interventi in queste Aule di Parlamento, che usavate come teatri, nonostante purtroppo i teatri fossero chiusi, per trasfigurarvi quando inveivate contro il Presidente del Consiglio e lo chiamavate criminale. Ma, a memoria di quello che avete fatto, restano i video e restano anche i video delle famose conferenze stampa di alcuni Presidenti di Regione, che in maniera esilarante mostravano come indossare le mascherine o cercavano di spiegare cosa era l'indice RT. Oggi continuate ad esercitare questa arte teatrale con una vera e propria farsa, perché state mettendo su un tribunale politico. L'avete ammesso in Commissione alla Camera, ma l'ha ammesso oggi anche il sottosegretario Gemmato, che nel suo discorso discorso questo ha detto. Questo tribunale ha una sentenza già scritta; questo tribunale rischia di generare un conflitto tra poteri dello Stato, perché decidere se una legge approvata dal Parlamento è o no conforme alla Costituzione non è potere nostro, ma è un potere della Corte costituzionale. Rischiate di far confliggere i poteri dello Stato, tanto che il Capo dello Stato ha dovuto ricordarvi che non esiste un contropotere giudiziario. Vi voglio chiedere: state processando solo Conte e il Governo Conte o pensate di dover processare anche gli operatori sanitari, valutando i protocolli che sono stati messi in campo? Che abbiate la volontà di punire il personale sanitario lo vediamo dal fatto che gli state anche tagliando le pensioni. *(Applausi)*. Oppure state processando gli scienziati? Magari voi siete più bravi a capire se quei vaccini funzionavano o non funzionavano. Noi siamo orgogliosi e siamo grati del lavoro

ci entriamo e lo facciamo sempre a testa alta, così come siamo entrati a testa alta nel Copasir da subito a chiarire quello che era successo. Io invece mi chiedo perché volete tener fuori le Regioni da questa Commissione d'inchiesta. Vi ricordo che nella scorsa legislatura questa Commissione d'inchiesta l'avevamo chiesta noi, portava la nostra firma il disegno di legge in cui si chiedeva di fare luce sulla gestione della sanità a 360 gradi: Regioni, struttura centrale, enti locali.

i malati Covid nelle RSA, che poi sono diventate dei focolai, dei *lager* in cui centinaia di anziani sono morti, le hanno emanate i Presidenti di Regione: come facciamo a non discutere di questo? *(Applausi)*. Io credo che l'Italia non abbia davvero bisogno dei patrioti da poltrona o da telecamera. L'Italia è un grande Paese ed è stato un grande Paese anche nel superare la più grande emergenza sociale e sanitaria dal dopoguerra ad oggi. Io di quei tempi certamente ricorderò i commoventi esempi di solidarietà degli imprenditori che hanno sacrificato il lavoro di una vita riconvertendo le loro aziende per produrre macchinari, attrezzature medicali e dispositivi di protezione; ricorderò l'esempio dei giovani che andavano a fare la spesa per gli anziani che non potevano uscire, degli operatori del 118 che non avendo i dispositivi utilizzavano le buste della spazzatura. Ascoltate un consiglio, ve lo voglio dare. Liberatevi dei fantasmi del passato e cominciate a guardare al futuro e a soprattutto al presente, perché c'è un Paese allo stremo, se non lo vedete! C'è un'emergenza liste d'attesa: quella sì richiede una Commissione d'inchiesta per trovare soluzioni. *(Applausi)*. Come affrontiamo il tema delle liste d'attesa? Come vogliamo intervenire sull'emergenza lavoro, sulle politiche attive del lavoro, sui mutui che le famiglie non riescono più a pagare? A noi piace molto il teatro, ma a questa farsa non vogliamo e non possiamo partecipare, pertanto voteremo contro l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Signor Presidente, senatrici e senatori, i momenti vissuti durante il periodo Covid rimarranno indelebili nella nostra mente. Io sono di Piacenza, una delle prime città colpite dopo Codogno, e ricordo ancora le telefonate, le corse a raccogliere i dispositivi medici e gli strumenti per proteggere il nostro personale sanitario e i nostri pazienti. Ricordo le consegne a qualsiasi ora con le strade vuote, il solo rumore delle ambulanze. io c'ero a supporto di chi ha continuato a lavorare con determinazione e non l'ho fatto per me, ma per senso civico, senza nascondere la paura nell'entrare quelle volte anche solo nella portineria dell'ospedale. Tutti noi abbiamo fatto qualcosa nel nostro territorio: gli imprenditori che hanno sacrificato e riconvertito le loro aziende, i giovani. Dobbiamo però essere obiettivi e dare una spiegazione a tutti quei pazienti, infermieri e medici che i loro figli non li rivedranno mai più. Lo dobbiamo a quei nonni chiusi nelle RSA, alla memoria storica del Paese che tanti sacrifici ha fatto per renderlo il più bello del mondo e che abbiamo perso. La democrazia nasce nell'analisi dei nostri errori, ma bisogna saperli correggere e non ripeterli. Non possiamo ricordarci solo la frase «va tutto bene» o «andrà tutto bene», perché con il numero dei morti che c'è stato non è andato tutto bene. Non c'era il piano pandemico, non c'erano dispositivi di protezione e se c'erano non erano a norma, non arrivavano i respiratori, non c'erano certezze, se non la restrizione della libertà personale. Per tutti questi morti, per tutto il personale sanitario, dobbiamo interrogarci sul perché del mancato aggiornamento del piano pandemico e della mancata sorveglianza. Per tutti loro ci dobbiamo interrogare sul perché dall'inizio dell'emergenza non siano stati adeguatamente acquistati materiali e dispositivi di protezione individuale, ci dobbiamo interrogare sulla mancata definizione della preallerta e dell'allerta, ci dobbiamo interrogare sul perché, da quando è stato dichiarato lo stato d'emergenza, siano passati quaranta lunghissimi giorni prima che si facesse qualcosa. Lo chiediamo anche per Giuseppe De Donno e Lucio Marrocco, due suicidi che la dicono lunga su come sia stato gestito il Covid. Lo chiediamo anche perché dopo il Covid i problemi di salute mentale sono aumentati del 25 per cento, soprattutto nei giovani, a fronte dell'isolamento e della solitudine.

La mancanza di *leadership* e di preparazione richiede invece un panorama ampio di responsabilità ministeriali e istituzionali che vanno corrette e sistemate per rinnovare il nostro sistema anche nell'emergenza-urgenza. Avete parlato e sparlato della Lombardia, ebbene in Lombardia c'erano 900.000 mascherine ferme che non abbiamo potuto utilizzare, lo stesso nel Lazio. Nelle Marche avete sequestrato i materiali per costruire i dispositivi, anche quelli che arrivavano in dogana a fronte di donazioni. In Calabria si moriva perché mancava l'ossigeno. Tutti - e dico tutti - i governatori regionali hanno segnalato inefficienza, ritardi e inadeguatezze, ma soprattutto quelli del centrodestra non si sono tirati indietro quando i consiglieri regionali gli hanno chiesto le Commissioni Covid. Avete comprato banchi a rotelle che non sono serviti se non a essere accantonati da quella parte. Quanto ci sono costati? Nell'esprimere il voto favorevole, naturalmente, della Lega, devo ribadire che noi vogliamo questa Commissione d'inchiesta perché non abbiamo paura della verità, perché vogliamo non dover perdere altri pezzi della nostra storia, perché ce lo chiede il popolo che ci ha mandati a governare, ce lo chiede il Paese, ma soprattutto ce lo chiede il nostro senso di responsabilità verso il nostro Paese che ha perso tanto. Non ci sono colpevoli, non è un processo. Soprattutto, bisogna ammettere che non c'è nulla da nascondere, a meno che abbiate qualcosa da nascondere voi, come quando i Cinque Stelle cambiavano i membri della Commissione sanità alla Camera perché non erano in linea con le restrizioni del Governo Conte II. Ma state sereni, la Commissione d'inchiesta non è un processo. L'unica persona a processo per aver difeso i confini e per le scelte che oggi sono state fatte e che risultano corrette è Matteo Salvini. Sulla base di quanto è già stato detto, per dissipare ogni dubbio sulla trasparenza di chi ha gestito la sanità in quel periodo anche nell'interesse di chi ne aveva la responsabilità istituzionale, siamo a esprimere il voto favorevole al disegno di legge. Auspichiamo che dal lavoro della Commissione d'inchiesta emergano elementi informativi utili anche per il rafforzamento dei processi di valutazione e il controllo istituzionale, nel contesto di una strategia più ampia che vada a coniugare la programmazione del Servizio sanitario nazionale con una effettiva dinamica dei bisogni da tutelare e con la necessità di una riprogettazione, di un rinnovamento complessivo anche dei professionisti sanitari. Tutto questo per contrastare gli sprechi, le inefficienze, le disfunzioni, le inappropriatezze, percorrendo la strada di una oculata razionalizzazione prima di continuare a generare del debito. Il 18 marzo, Giornata per le vittime Covid che abbiamo istituito nella scorsa legislatura, non deve rimanere una data, ma deve avere risposte che la Commissione d'inchiesta sicuramente saprà dare.

dalle conclusioni del ministro Speranza a Montecitorio, quando, in una giornata non semplice certamente per il Partito Democratico, ma per tutti i partiti che hanno assunto la responsabilità di Governo, sia nel Governo Conte II, sia nel Governo Draghi - era evidente l'amarezza del Ministro della salute.

non solo con questo voto, ma soprattutto dopo: faremo di tutto per farvi cambiare idea in questi minuti, ma temo che sarà difficile far cambiare idea a chi pensava che

Molte persone erano amici, alcuni parenti, altri conoscenti, altri ancora collaboratori. Non ci sono più persone che hanno servito lo Stato e non ci sono più persone che hanno servito la sanità, senza sapere cosa stesse accadendo in quei giorni.

Sì, ma lei si preoccupava del fatto che suo figlio non abbia potuto partecipare agli allenamenti di *basket* e non era quella la priorità per il Paese in quelle settimane. Noi l'abbiamo ascoltata, ora ascolti: si faccia rappresentare dai suoi amici no vax. Il 23 febbraio 2020 per me è il giorno in cui inizia un altro pezzo di storia per il nostro Paese: ognuno di noi ha negli occhi il giorno in cui ha capito che c'era il Covid e per me è il 23 febbraio del 2020, il giorno in cui il Governo Conte II varò il primo decreto-legge con il quale intervenne pesantemente nell'organizzazione sanitaria e attraverso il centro dell'organizzazione sanitaria delle Regioni. Il 23 febbraio è una data che ho particolarmente nel cuore: mio padre compiva ottant'anni, eravamo casualmente insieme - è una coincidenza storica - a sentire Papa Francesco che era a Bari, in un grande piazzale, con un sole straordinario, c'era anche il Presidente Mattarella,

Prima ci hanno dato degli untori, molti Paesi in Europa e nel mondo; poi han capito che non eravamo gli untori, ma che eravamo stati i primi in Europa,

ai colleghi della maggioranza, che pensano di utilizzare come una clava una Commissione bicamerale d'inchiesta, e qui mi associo alle parole del presidente Casini sull'utilizzo improprio delle Commissioni d'inchiesta. Vorrei lasciare nella loro memoria, per non ripeterle, le parole del collega Franceschini su quanto dobbiamo essere legati alla difesa della credibilità dell'istituzione che rappresentiamo. Ma vorrei ricordare, ai colleghi Lega e Fratelli d'Italia, che, dal 23 febbraio del 2020, ci sono stati quattordici decreti-legge fatti in emergenza, in emergenza vera, che hanno toccato, quasi tutti, l'emergenza epidemiologica e, molti di essi, hanno riguardato interventi per le imprese. Avete votato contro la liquidità alle imprese, avete votato contro gli ammortizzatori straordinari per tutte le imprese. Per la prima volta la Repubblica italiana ha avuto ammortizzatori sociali straordinari. Susanna Camusso e Annamaria Furlan sono state protagoniste di quelle mediazioni. Anche un bar con un solo dipendente aveva la possibilità di ottenere un ammortizzatore sociale. Non era mai successo nella storia delle relazioni industriali italiane. *(Applausi).* Avete votato contro i ristori. Sì, contro i ristori. Mi dispiace che il senatore Renzi non sia in Aula. Se il senatore Renzi è stato diretto destinatario di una comunicazione fatta dagli organi dello Stato, è perché, probabilmente, a partita IVA un'impresa fa *business*, a differenza di chi non lo fa. Ha fatto bene a dir di no, ma lì c'era l'emergenza, rispetto alla quale tutti coloro che avevano una partita IVA ed un'impresa si sono ritrovati la comunicazione dello Stato. Lo Stato doveva preoccuparsi di tutti: dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, di chi viveva sotto la soglia di povertà. E ci hanno pensato i sindaci a portare la busta della spesa a casa, e ripeto i sindaci. *(Applausi)*. Parliamo delle Regioni. Certo, parliamo delle Regioni. Ho avuto la responsabilità di coordinarle in quei momenti drammatici. Eviterò, per rispetto istituzionale verso quei Presidenti, di fare i nomi di chi ci ha supplicato, dall'8 e 9 marzo in poi e certamente fino alla riapertura del 4 giugno - non ho dimenticato

affannati nel dirci come funziona la sanità, salvo poi smontarla. La cosa che ci fa più male, infatti, è che non avete capito

che si è sottoposto volontariamente alla fallimentare - lo aggiungo con rispetto - Commissione d'inchiesta della regione Lombardia. Io ci sono andato, mi sono sottoposto a tutte le domande. Ad un certo punto, non c'erano più domande,

non da un uomo solo al comando, non da Giuseppe Conte, non da un Ministro, Speranza, Boccia o Franceschini, ma dal Dipartimento per la protezione civile, che ogni giorno si riuniva due volte al giorno, alle 9 del mattino, con tutti i tecnici delle Regioni, e alle 15, puntualmente, attraverso il Ministro, con tutti i Presidenti di Regione. Noi abbiamo vissuto così per tre mesi e mezzo. Forse a qualcuno è sfuggito, forse qualcuno ha perso la memoria. Mentre voi dicevate: aprite, noi dicevamo: chiudiamo. Mentre voi dicevate: il Covid-19 non esiste, noi dicevamo: andiamo avanti e difendiamo - come ha ricordato opportunamente il presidente Franceschini - il diritto alla salute

e su quelle storie. E non venga in mente a nessuno di pensare che strumentalizzare il dolore di una parte dei parenti può diventare azione politica, perché è sciacallaggio e anche di basso livello.

tema sarà molto, ma molto più sentito anche in Commissione bicamerale. Lo voglio anticipare. Stiamo cercando di farvi capire che state facendo un errore gravissimo, ma nella Commissione queste saranno la puntualità e la passione con le quali affronteremo questi temi. di quanti pazienti sono stati portati con gli elicotteri di notte, da quali ospedali a quali ospedali. PRESIDENTE.Senatore Boccia, siamo al quinto minuto oltre il tempo. Ho grande rispetto e capisco l'importanza della discussione, ma lei non mi metta in difficoltà. BOCCIA Signor presidente, dietro la Protezione civile, dietro l'Esercito italiano, non ci sono i nomi di chi guida quei dipartimenti o quelle parti dello Stato: ci sono migliaia di donne e di uomini che li servono con disciplina e onore. Aver messo in discussione, sia ai fini politici sia ai fini di propaganda che sono tutti dentro l'idea di questa Commissione, alcune personalità che hanno guidato la Protezione civile e gli apparati dello Stato è stata un'operazione che ha minato la credibilità di quelle istituzioni,

Presidente, mi ero ripromesso, nell'essere presente in Aula il più possibile in questa giornata, di tentare di fare un intervento Non è proprio nelle mie corde, non è proprio quello che mi riesce più facile, non è proprio la mia aspirazione nel fare politica, ma mi ero ripromesso in questo dibattito di fare un intervento pacato in linea anche con il lavoro che abbiamo svolto. Dopo aver ascoltato l'intervento del presidente Boccia e di qualche altro senatore, confesso che la mia difficoltà è elevata. Cerco, però di restare sull'auspicio. Presidente, abbiamo adottato un approccio molto aperto nel discutere il testo in esame; lo abbiamo affrontato in Commissione, abbiamo fatto due letture vere sia alla Camera che al Senato. In Commissione abbiamo anche operato un'attività emendativa importante, abbiamo corretto alcuni passaggi del testo che anche a noi suscitavano perplessità. Devo dire che di questo io sono personalmente molto soddisfatto come Presidente della 10a Commissione decima che ha affrontato il lavoro. È stato un lavoro puntuale e preciso, e a tal proposito ringrazio il relatore Gianni Berrino, ma anche tutti i componenti della Commissione. quello che è successo in Commissione paradossalmente non trova riscontro nel dibattito che si è svolto invece in Aula. Credo che noi abbiamo il dovere di fare questa Commissione. Colleghi dell'opposizione, lasciatevi dire quanto segue

entrare nella Commissione e nei suoi lavori deve mettere tutta quell'energia qui espressa - e, a mio avviso, anche un po' mal riposta - per tentare di fare un lavoro serio in quella sede. Verificato che questo non sarà possibile, verificato che tutti i processi alle intenzioni che voi avete declamato nel dibattito d'Aula si saranno realizzati, farete sempre in tempo eventualmente ad adottare un altro atteggiamento. Ma non si può partire fin dall'inizio negando la necessità di fare e poi, collega Patuanelli, dire che, se votiamo l'emendamento, voi la votate; non si può negare la necessità di farla davanti a quella che è stata una vera e propria notte della Repubblica. Noi in quel periodo abbiamo vissuto una notte della Repubblica e abbiamo pagato un tributo pesantissimo. Collega Boccia, sinceramente, ma di che cosa ci dobbiamo vantare? Abbiamo realizzato il maggior numero di decessi tra i Paesi europei e il maggiore abbattimento di prodotto interno lordo nel primo anno di pandemia, proprio in virtù delle chiusure che abbiamo fatto,

Abbiamo approvato 180 miliardi di scostamento di bilancio, complessivamente. Quindi, come si fa a dire che noi ci siamo chiamati fuori? Come si fa a dire che noi stavamo dalla parte dei no vax e dei negazionisti?

Abbiamo vaccinato 50 milioni di italiani e abbiamo pagato un tributo di 192.406 morti, che risultano dal censimento. Abbiamo pagato un tributo di decessi economici per le chiusure, a cui siamo stati obbligati più o meno d'accordo. Su qualcosa eravamo d'accordo, mentre su qualcosa avremmo agito con dettagli diversi, ma generalmente noi siamo stati sempre d'accordo che bisognava intervenire seriamente per impedire la la vicinanza tra il portatore di Covid e gli altri sani. Io ricordo le discussioni in Aula con il ministro Speranza, quando dicevo che dovevamo fare 500.000 tamponi al giorno, perché era l'unico modo per verificare dove stavano i cosiddetti portatori senza sintomi del Covid. Tutte queste vicende noi le abbiamo vissute, ma mai ci saremmo sognati

ricordate? Allora, è ovvio che sui dettagli ci possiamo dividere. È del tutto evidente che possiamo avere dei punti di riferimento diversi, ma sul farla o non farla non è possibile dividersi. Non è possibile che il Parlamento italiano dica che quello che è successo nei due anni di Covid al Parlamento italiano non interessa: non è possibile. Poi è ovvio che i dettagli fanno parte del gioco e noi li accettiamo tutti. Io voglio sperare che alla fine un sussulto di obiettività sopravvenga Credo che quello che dobbiamo fare adesso, Presidente, è votare rapidamente questa Commissione, istituirla facendo in modo che sia una delle tante Commissioni esistenti, ma anche che le vengano dati i mezzi e gli strumenti e soprattutto l'attenzione che è stata promessa dall'opposizione. Io sono convinto che la stessa energia ci sarà - attenzione - anche da parte della maggioranza. Occorre fare in modo che questa Commissione rapidamente ci dica che cosa è successo: ci dica quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e faccia in modo che, qualora dovesse succedere una nuova emergenza pandemica, uguale o simile a quella che noi abbiamo subito, gli errori commessi non vengano ripetuti. Guardate che di errori fatti ce ne sono stati tantissimi.

non c'è un protocollo per affrontare un'eventuale nuova epidemia, uguale o simile a quella del SARS-CoV-2. È ovvio che ci sono state lacune pesanti. Quindi, colleghi, do tutto il mio contributo di esperto di opposizione, ma fateci fare la Commissione. Mettete in chiaro quello che voi intendete realizzare, attraverso un lavoro serio di questa Commissione, fate parte della Commissione e, al verificarsi del lavoro serio, portiamo avanti la Commissione tutti insieme. Se noi dovessimo fare tutto quello che voi avete sospettato, cioè il plotone d'esecuzione e chi più ne ha più ne metta, fate sempre in tempo a denunciare che un simile atteggiamento

che senso ha questo atteggiamento? Spiegatemi che senso ha questo atteggiamento. Io glielo do un senso. Ho finito, Presidente. Non voglio fare il processo alle intenzioni, perché francamente io accuso sempre gli altri, e quindi figuriamoci. Ma sembra proprio che fate come i tacchini col Natale,

Se secondo voi è andata bene, con il *record* di decessi e con il più grosso abbattimento di prodotto interno lordo, fate voi. Io credo che gli italiani, che ci ascoltano e ci giudicano, sapranno anche giudicare chi è coerente con quello che ha fatto e ha detto in tutti questi anni e chi invece è totalmente incoerente.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso dal Gruppo, dissenso mio personale, ma che è anche espressione del dissenso del Gruppo in Senato di Azione. Le Commissioni di inchiesta servono per cercare la verità e avere strumenti di approfondimento e conoscenza. Qui nessuno ha paura della ricerca della verità. Il Paese, le famiglie italiane colpite da lutti durante la pandemia pretendono che si faccia luce sulla verità. Ma il testo che stiamo approvando oggi in Aula, diversamente dalle intenzioni, costituirà un ostacolo alla ricerca della verità dei fatti e non contribuirà a creare una memoria condivisa su una ferita aperta nel Paese. La verità non può e non deve essere piegata sulla base della convenienza politica. Voglio essere molto chiaro: Azione nasce come partito in dissenso rispetto ai partiti che avevano dato vita al Governo Conte II. Nessuno più di noi di Azione avrebbe il titolo e la libertà per attaccare le scelte di quel Governo. Ma usare una Commissione Covid per vendetta politica è un errore che chiunque si definisce garantista non dovrebbe mai commettere. Oggi è facile dire cosa avremmo fatto o cosa avremmo dovuto fare, con gli occhi di dopo. Oggi è comodo dire che il ministro Speranza avrebbe dovuto fare questo o quello. Ma bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che, come Paese, eravamo tutti impreparati davanti a una pandemia sanitaria. *(Applausi)*. Troppo comodo dire oggi cosa avremmo dovuto fare ieri. Se l'idea è avere elementi di conoscenza perché questo non si possa più ripetere, allora non c'è bisogno di una Commissione parlamentare d'inchiesta per il Covid. C'è bisogno della fatica di leggere gli atti delle istituzioni europee, che stanno dicendo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Se vogliamo chiederci perché le forze armate russe sono entrate nel nostro territorio, non c'è bisogno di una Commissione Covid: c'è bisogno di raccogliere l'allarme delle istituzioni europee sul rischio di ingerenza dei Paesi stranieri sulle prossime elezioni democratiche. Istituire una Commissione senza entrare nella competenza delle Regioni, senza poter valutare gli atti dei Comuni, delle ASL, delle aziende sanitarie, delle RSA per anziani non restituirà la verità per i morti di Covid a Bergamo e in tutto il resto d'Italia, ma rischia di restituirci solo una manipolazione della ricerca della verità per fini politici, per valutare gli atti compiuti dal Governo Conte II e dal Governo Draghi. Con quale coerenza e credibilità le forze politiche che erano in maggioranza di quei Governi ora possono rimettere in discussione... Concludo in un minuto, Presidente. C'è un tema che non è solo politico, ma è anche giuridico. Questi atti aventi forza di legge sono stati in alcuni casi promulgati dal Presidente della Repubblica, che, nel discorso alla cerimonia del Ventaglio, ha usato parole molto precise: esiste un organo che valuta la legittimità costituzionale e questo organo si chiama Corte costituzionale. *(Applausi)*. Non è una Commissione parlamentare. Ci sono degli organi precisi che hanno i ruoli e i compiti per affermare queste cose. Chi oggi dà voce ai no vax contro la ricerca scientifica e il procedimento di validazione non sta dalla nostra parte, dalla parte di Azione. Per questo noi voteremo contro l'istituzione di questa Commissione.

"Il link apre una nuova finestra"). Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio di oggi, l'ordine del giorno della seduta di domani, con inizio alle ore 10, prevede la discussione dei seguenti argomenti: dalla sede redigente, disegno di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge in materia di associazioni sindacali militari e delega revisione strumento militare; decreto-legge in materia di politica di coesione e immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati, in ordine al quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia; decreto-legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali; legge annuale per il mercato e la concorrenza. È un programma ottimistico. È stato altresì stabilito che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge concernenti la Commissione d'inchiesta e la delega al Governo saranno di cinque minuti.

Signor Presidente, parlo di calcio e forse interessa a qualcuno. Non so se sapete che le vicende dello stadio di San Siro di Milano si sono fermate sul vincolo giustamente apposto. La squadra del Milan sta quindi cercando una soluzione alternativa: ha puntato gli occhi su un'area dell'*hinterland* di Milano, in città metropolitana, nel Comune di San Donato Milanese, nella zona Sud-Est di Milano, e ha recentemente depositato il progetto presso il Comune e chiesto una variante al piano urbanistico. Peccato che non abbiamo una legge sul consumo di suolo in Italia. Visti i recenti avvenimenti sul dissesto idrogeologico, questo progetto sarebbe da bocciare *a priori,* per i gravi danni che andrebbe a causare al territorio. Dal punto di vista ambientale andrà costruita una piattaforma di cemento spessa sette metri e larga 106.000 metri quadri, che andrà a galleggiare sulla falda acquifera del Sud-Est di Milano. il danno ulteriore e gravissimo è quello culturale, perché quest'area è inserita nel parco agricolo Sud, dove insistono l'abbazia cistercense di Chiaravalle (quindi medievale) e il borgo medievale di Chiaravalle.

Questo intervento andrebbe a far sì che la ciribiciaccola dell'abbazia di Chiaravalle, ovvero il campanile, avrebbe come sfondo il cemento di un mega stadio alto 50 metri, con tutto quello che comporta un'edificazione del genere: chiaramente rumori.

C'è tanto da recuperare di già edificato e non si può pensare di costruire sul terreno libero con una piattaforma di 106.000 metri quadri di cemento al posto del verde, con buona pace del dissesto idrogeologico e della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.